Comunico che in data 28 luglio 2023 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali* «Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento» finestra"). Comunico altresì che in data 31 luglio 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» (829). **Sulla grazia concessa all'ex presidente Signor Presidente, intervengo per esprimere, a nome di tutti i colleghi dell'Interparlamentare, la nostra soddisfazione per la grazia

Questo atto che si estende al Presidente della Repubblica e ad alcuni esponenti del Governo legittimamente eletto e indebitamente destituito dai generali, è un primo passo - noi speriamo - verso la normalizzazione. Vorrei anche ricordare che pochi anni fa la *leader* birmana è stata qui, in un'Aula del Senato ed ha avuto la possibilità di un incontro con tanti di noi. Voglio dirvi che questo atto ovviamente non modifica il nostro giudizio su un regime illiberale, che ha creato ogni sorta di lutto per il popolo birmano, costretto all'esilio migliaia di esponenti della società civile e che continua a praticare uccisioni di massa assolutamente intollerabili. Ci auguriamo

un abbraccio ideale di quest'Aula va a San Suu Kyi, che ha tanto sofferto nella sua vita e che in questo momento, non dico abbia risolto i problemi suoi o del proprio popolo, ma vede un minimo di speranza in fondo a un *tunnel* di lutto e di disgrazia. Grazie a tutti Restano fermi gli argomenti all'ordine del giorno della seduta di oggi: informativa del Ministro per la protezione civile sulle emergenze derivanti da eventi calamitosi eccezionali e comunicazioni del Ministro per gli affari europei sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nella seduta di domani saranno discussi il disegno di legge delega fiscale, collegato alla manovra di finanza pubblica, e il decreto-legge concernente organizzazione della pubblica amministrazione, sport e Giubileo. Poiché il Governo ha preannunciato che, al termine della discussione generale, porrà la questione di fiducia sul predetto decreto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, la Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del relativo dibattito. Si è stabilito che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. La chiama è prevista nella mattina di giovedì 3 agosto. Sempre giovedì 3, alle ore 15,30, in luogo del *question time*, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali terrà un'informativa sul reddito di cittadinanza. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti. Il calendario dei lavori della settimana prevede, inoltre, con sedute fino a venerdì 4 agosto, se necessario, la discussione del decreto-legge concernente la tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. La prossima settimana l'Assemblea si riunirà per l'eventuale seguito di argomenti non conclusi, lunedì 7 agosto, alle ore 12. agosto | h. 15 | - Informativa del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare sulle recenti emergenze derivanti da eventi calamitosi

l'informativa di questo pomeriggio al Senato consente di riferire, come mio dovere, elementi spero utili per comprendere e apprezzare l'eccezionale sforzo operativo che il servizio nazionale della Protezione civile ha svolto e sta ancora svolgendo assicurando sia livello centrale di coordinamento, sia a livello territoriale operativo il massimo sforzo per mitigare l'impatto e le conseguenze dei fenomeni estremi che si sono verificati in Italia al Nord e al Sud dal 19 luglio in poi. Terrei distinti per maggiore chiarezza gli eventi del Nord Italia, anche per la loro specificità, rispetto alla situazione calamitosa nelle Regioni del Sud della Nazione. A partire dal 19 luglio è stato emanato un avviso nazionale di condizioni meteorologiche avverse per precipitazioni a prevalente carattere temporalesco accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento a partire dal pomeriggio dello stesso 19 luglio e per la notte a seguire su Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Trento e Bolzano. La previsione ha indotto quelle Regioni e le due Province autonome ad una valutazione della criticità idrogeologica per temporali e all'emissione di conseguenti allerte gialle e arancioni per diversi giorni. L'evoluzione della situazione è stata monitorata, come sempre accade in questi casi, anche a livello centrale dal Dipartimento della protezione civile ventiquattro. Il primo dato triste che mi sento di riferire è che nel Comune di Lissone si è verificato, purtroppo, il decesso di una donna che camminava a piedi in località di Corteno Golgi una ragazza, mentre dormiva in una tenda in un campo *scout,* è stata raggiunta dalla caduta degli alberi. Il nostro pensiero va a queste vittime e alle tre che si sono registrate

il Consiglio dei ministri, su proposta del sottoscritto, delibera lo stato di emergenza di rilievo nazionale, fissandone di volta in volta la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di Protezione civile, individuando altresì le prime risorse finanziarie da rendere disponibili a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Tale deliberazione viene adottata sulla base di un'istruttoria tecnica che consenta di inquadrare gli elementi di base richiesti dalla norma. La deliberazione avviene su proposta della Regione o della Provincia autonoma interessata in relazione agli eventi occorsi e poi si procede con le determinazioni del Governo.

Il Dipartimento sta coordinando, insieme alle strutture tecniche regionali, la raccolta uniforme dei dati e delle informazioni di base, comprensiva di una prima stima dei principali danni rilevati al fine di addivenire, anche all'esito di opportuni sopralluoghi effettuati con i tecnici dei due dipartimenti (nazionale e regionale), alla predisposizione delle proposte di deliberazione di stato di emergenza che, non appena disponibili, valuteremo e sottoporremo alla condivisione del Governo. In questo momento non è possibile fornire una ipotesi di quantificazione delle esigenze, data la vastità del territorio e la specificità dei fenomeni che hanno avuto impatti così rilevanti. Le Regioni interessate, con il supporto dei sistemi territoriali di Protezione civile e il Dipartimento nazionale, sono impegnati al massimo per completare le valutazioni tecniche necessarie nel più breve tempo possibile, al fine di consentire, con ogni possibile urgenza, al Consiglio dei ministri di adottare tempestivamente le necessarie determinazioni. Dopo che il Consiglio dei ministri avrà eventualmente dichiarato lo stato di emergenza nazionale, con ordinanze di protezione civile si potrà provvedere alle varie tipologie di interventi e azioni. Ne sintetizzo alcuni: interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale, interventi anche strutturali per la riduzione del rischio residuo. È chiaro che per quanto riguarda la valutazione dell'impatto, se volete, io potrei entrare nei particolari

puntualmente questa fase dell'informativa per rispetto del successivo punto all'ordine del giorno mi induce a chiedervi clemenza se non entro troppo nei particolari. Le ordinanze di protezione civile potranno regolare, quindi, le azioni di cui ho appena parlato prevedendo specifiche e circostanziate deroghe alle normative ordinarie, allo scopo di semplificare e velocizzare l'attuazione degli interventi. Mentre sulle Regioni settentrionali venivano fronteggiati gli eventi cui ho appena accennato, eventi gravi e per alcuni versi anche inediti, sulle Regioni meridionali la massa d'aria in risalita dall'entroterra nordafricano apportava un'ondata di calore a carattere di assoluta eccezionalità, sia nell'intensità che nella persistenza, facendo registrare temperature superiori ai 40 gradi, con punte fino a 46-48 gradi, cioè valori superiori ad ogni precedente *record* storico. Al Centro-Sud e nelle isole si è assistito ad una predisposizione graduale, quindi, della vegetazione al passaggio del fuoco, con conseguente aumento delle condizioni di pericolosità, che in giornate particolarmente ventose e calde - soffiava un impetuoso vento di scirocco vento di scirocco - come quella del 25 luglio, hanno favorito lo sviluppo e la propagazione degli incendi boschivi. In conseguenza delle condizioni particolarmente severe, il dipartimento della Protezione civile ha assicurato l'azione di propria competenza per il coordinamento degli assetti aerei, composti sostanzialmente da *canadair* e da elicotteri della flotta aerea dello Stato a supporto delle operazioni svolte a terra dalle squadre specializzate. Le azioni specifiche e mirate presso l'unità di crisi dipartimentale hanno coinvolto anche il centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comando operativo di vertice interforze delle Forze armate, le Regioni Sicilia e Calabria e le prefetture interessate. Com'è a tutti noto, per la legge quadro in materia di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, la n. 353 del 2000, la competenza primaria per lo svolgimento delle attività di prevenzione e lotta attiva al fenomeno degli incendi boschivi è delle Regioni e delle Province autonome. L'intervento da terra è rinforzato dalle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, anche a seguito dello scioglimento del Corpo forestale dello Stato, hanno acquisito risorse e competenze specializzate. In questo dispositivo si integra la flotta aerea di Stato, composta da apparecchi ad ala fissa e rotante resi disponibili dalle diverse amministrazioni centrali e coordinate, sul piano tattico e operativo, dal centro operativo aereo unificato del dipartimento della Protezione civile. Oltre alla gestione del concorso della flotta aerea dello Stato, il dipartimento ha monitorato l'evolversi delle criticità connesse agli incendi che hanno interessato diversi territori italiani, tra cui, in particolar modo, quelli delle province di Messina, Catania, Trapani, Siracusa e Palermo, determinando l'evacuazione precauzionale di numerose abitazioni, provocando l'interruzione dei servizi di fornitura di energia elettrica e delle comunicazioni e gravi problemi alle infrastrutture di mobilità stradale e ferroviaria. Si rileva, inoltre, il decesso di due persone, come ho accennato all'inizio, nel Comune di Cinisi e di una nel Comune di Cardeto, in provincia di Reggio Calabria. Nello stesso Comune si sono registrate due persone gravemente ustionate a causa delle fiamme.

Nella stessa giornata si sono verificate diverse criticità nella gestione operativa delle richieste di concorso aereo. In particolare, a causa delle forti correnti d'aria ascendenti e discendenti, la flotta aerea della Regione Siciliana non ha potuto effettuare, nella provincia di Trapani e in quella di Palermo, per mancanza delle condizioni di sicurezza necessarie, alcuni interventi per parte della giornata del 25 luglio. In Calabria, a causa delle temperature elevatissime, sulla pista dell'aeroporto di Lamezia Terme per alcune ore non è stato possibile il decollo di alcuni mezzi. Si è provveduto a distaccare, sempre nelle giornate del 25 e 26 luglio, un velivolo *canadair* della flotta di Stato sotto la gestione dei Vigili del fuoco per l'incendio che ha interessato la vasta discarica di Bellolampo poco distante da Palermo. Nella giornata del 26 luglio le richieste di concorso aereo per gli incendi boschivi risultano essere state ventiquattro: otto in Sicilia, sette in Calabria, quattro in Sardegna, tre in Puglia, una in Abruzzo e una nel Lazio. è stato possibile a seguito della disponibilità di una flotta sulla quale se mi consentite - più avanti mi permetterò di intervenire brevemente. Vorrei riportare l'elenco, trasmessoci dalla direzione generale dell'Enel, delle interruzioni in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna registratesi fra il 13 luglio e il 25 luglio. L'infrastruttura elettrica ha subito diverse interruzioni dovute principalmente a fulminazione e forte vento, che hanno causato la caduta sulle linee aeree di media tensione di numerosi alberi posti al di fuori delle fasce di rispetto. Nella maggior parte dei casi, il servizio elettrico è stato interamente ripreso da manovre eseguite da remoto e in campo, grazie alla selezione del tratto che ha registrato il guasto e alla rialimentazione di altra linea. Si tratta di fenomeni che hanno portato numerosi danni anche all'infrastruttura stradale, rendendo spesso difficoltose le operazioni in campo. Le Regioni maggiormente interessate nel Sud Italia, a partire dal 12 luglio, dall'interruzione dell'erogazione di energia elettrica sono state la Campania, l'Abruzzo, la Puglia e soprattutto la Sicilia. Nell'isola il fenomeno di ondata di calore si è particolarmente concentrato nelle Province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Catania, costringendo in alcuni momenti alla disalimentazione di oltre 100.000 utenti, il che naturalmente ha creato difficoltà facilmente comprensibili, se si tiene conto che la temperatura all'esterno lambiva i 46 gradi.

ricorrere, in tempi ragionevolmente brevi, alla riparazione dei guasti. Non sono aduso a fare riferimenti personali e di questo vi chiedo scusa, lasciatemi dire, parlando della Sicilia, che nei giorni scorsi mentre la mia isola, assieme ad altre Regioni italiane, faceva i conti con incendi devastanti, alcuni giornali - non certo di area governativa - e membri di questo Senato si attardavano nella ricerca di archivio di inadempienze legate al mio trascorso ruolo di Presidente di quella Regione per una legislatura. Preferirei in verità essere contestato per le attività di Ministro, ma essendo stato per tanti anni all'opposizione - come si si suol dire - conosco il mestiere. Quando si indicano percorsi e possibili obiettivi da questo banco di Governo, occorre essere sempre credibili; non immuni da errori naturalmente, ma credibili. Nel mio non breve percorso politico, ovunque chiamato dal voto popolare credo di aver attraversato le paludi senza mai prendere la malaria e lo dico con assoluta umiltà, senza superbia, ma con la serena consapevolezza di aver fatto sempre il mio dovere. Se diciamo che la tutela del territorio costituisce una priorità, alle parole dobbiamo far seguire i fatti. Non ho diritto a repliche, come vuole il Regolamento in caso di informativa, ma credo non sia di cattivo gusto capire come la Sicilia sia arrivata a questa particolare, intensa, grave e drammatica stagione di incendi senza comprendere quello che è stato fatto negli ultimi anni per quell'isola.

realizzate in Sicilia e dopo cinquant'anni mai collaudate, con il risultato che non possono essere utilizzate appieno perché costituiscono un serio e costante pericolo. C'è stata la pulitura dei fiumi; quasi 500 milioni contro il dissesto idrogeologico, l'acquisto di 150 *pick-up* antincendio e di altri 122 mezzi antincendio. Dico questo e vi chiedo scusa per il riferimento, che non è personale, ma alla Sicilia - perché è ovvio che, quando si tratta di dovere valutare le cose fatte, fatte male o non fatte, diventa assolutamente facile ricorrere alle ricerche di archivio. Abbiamo il dovere di comprendere e di capire che cosa fare, altrimenti questa informativa diventa uno sterile e triste rito di elencazioni, che finisce anche con il dovere lambire qualche sentimento di larvata ipocrisia. Cosa fare?

Il tema è il riproporsi di eventi calamitosi, che impone al Governo una riflessione davvero seria e profonda. Quando il Presidente del Consiglio dice che la tutela e la difesa del territorio diventano una priorità nell'agenda di Governo, credo che faccia un'ammissione assolutamente responsabile. Il tema è la programmazione della prevenzione, la prevenzione strutturale. Abbiamo avviato verso il varo il disegno di legge sulla ricostruzione, con un modello unico di ricostruzione.

La cultura del rischio non pare essere particolarmente diffusa. Come dicevo l'altro giorno alla Camera - e non ho difficoltà a ripeterlo qui in Senato

affinché le esercitazioni di protezione civile coinvolgano tutto il mondo scolastico, a cominciare dalle scuole elementari perché le esercitazioni servono a creare una coscienza e una cultura del rischio. Poi dobbiamo accelerare con l'adozione dei piani di adattamento al cambiamento climatico. Se ne parla dal 2016

sono i piani comunali di Protezione civile che molto spesso non vengono adottati e quando avviene non vengono sottoposti alla revisione. C'è un grave problema nella politica di prevenzione, repressione e neutralizzazione degli incendi ed è quello legato alla flotta aerea dello Stato, tema a cui più volte ho fatto cenno. Come Come sanno gli onorevoli senatori e l'onorevole Presidente, la previsione, la prevenzione e il contrasto attivo agli ingenti boschivi, in un'epoca come la nostra contraddistinta dal cambiamento climatico (e qui non ci sono negazionisti, lo voglio ribadire), rappresentano un impegno centrale per il Servizio nazionale di Protezione civile, anche nell'ambito del più ampio quadro europeo di gestione delle emergenze. La possibilità di far fronte a tale impegno in maniera efficace, purtroppo, incontra un limite oggettivo nell'attuale indisponibilità a livello europeo di una flotta antincendio adeguatamente dimensionata e moderna, che sia in grado di garantire un intervento tempestivo e simultaneo anche in più scenari operativi. Per rispondere a questa esigenza, la Commissione europea ha avviato nel 2021 interlocuzioni con le principali industrie aeronautiche europee, al fine di verificare la possibilità di sviluppare e produrre un nuovo velivolo, cosiddetto anfibio, in grado di sostituire gli attuali Canadair, che vengono realizzati in regime, purtroppo, di monopolio in tutto il mondo. Noi abbiamo avviato con la società per azioni Leonardo

di produrre e fornire, non soltanto all'Italia, ma anche alla flotta dell'Unione europea, questo tipo di velivolo, del quale purtroppo si avverte il dramma del numero limitato nei momenti drammatici della gestione delle crisi. Ed è quanto avvenuto purtroppo anche quest'anno. Non credo sia marginale ricordare che gran parte degli incendi sviluppatesi nelle Regioni del Sud sia di origine dolosa; non sappiamo ancora se piromani o incendiari per la sottile differenza che bisogna necessariamente fare, ma in Sicilia, in Puglia e in Calabria sono tanti gli incendi originati dal dolo e quindi dalla volontà criminale dell'uomo. dell'uomo. Al di là dell'inasprimento della pena, che è stato disposto con una norma del 2021, credo che sia giusto esaminare l'opportunità di un'aggravante per chi commette tale reato nell'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. È un tema che sto affrontando col collega Nordio e del quale naturalmente il Parlamento sarà reso edotto. Appare estremamente importante procedere ad un nuovo intervento normativo con l'introduzione di ulteriori strumenti funzionali all'attività di contrasto al fenomeno, in grado cioè di favorire l'azione sia preventiva che repressiva, spezzando quel circuito vizioso che connette gli incendi boschivi a lucrose occasioni di guadagno per soggetti privi di scrupolo. L'obiettivo è rafforzare il sistema di protezione dei nostri boschi estromettere dal circuito operativo i soggetti che hanno volutamente cagionato, per biechi interessi economici, gli incendi che hanno devastato migliaia e migliaia di ettari. Il cambiamento climatico c'è e non da oggi. C'è da almeno quindici ormai non può più essere un alibi. Ecco perché il cambiamento climatico non può essere un alibi per quanti fanno finta di non capire che serve un cambio di passo!

Quando dico che la cultura del rischio non pare sufficientemente diffusa, lo dico a ragion veduta, per i numerosissimi casi di incendio che si sono verificati nelle campagne a causa delle mancate misure preventive, che peraltro le norme vigenti pongono a carico dei proprietari

interventi strutturali, che devono passare attraverso strumenti di pianificazione e di programmazione.

e di obiettivi, legato alla gerarchia degli interventi che ogni forza politica e ogni Governo ritengono di dover redigere (a volte anche sbagliando, per carità, perché nessuno è depositario di certezze). Per questo Governo, però, il tempo degli interventi a pioggia per metterci non al sicuro, ma per mitigare i rischi legati al cambiamento climatico, è finito: servono strumenti di programmazione che coinvolgano i Governi locali, regionali e nazionali.

di dire una cosa e farne un'altra a proposito dei fondi del PNRR legati alle misure di prevenzione. È fin troppo noto ed è accessibile a tutti come alcuni studi elaborati assai di recente, non ultimo quello della Banca d'Italia,

Se l'opera pubblica supera l'importo di cento milioni, servono quindici anni e sei mesi. È chiaro che questo potrebbe anche riguardare qualsiasi opera pubblica, ma non è così.

le infrastrutture fluviali sono quelle che richiedono la maggiore quantità di tempo:

i fondi destinati alla lotta al dissesto idrogeologico non avrebbero mai potuto trovare alimento nel PNRR *(Applausi)*, visto che la scadenza è a giugno 2026 fine avremmo dovuto spiegare a Bruxelles perché gran parte di quei fondi sarebbe rimasta assolutamente inutilizzata. Abbiamo invece il dovere - questo sì

che invece hanno una scadenza molto più ampia rispetto ai fondi del PNRR. L'ultimo tema che vorrei affrontare con quest'Assemblea così attenta e silenziosa *(Applausi.

Con la fornitura tempestiva di fondi per la ricostruzione, infatti, come ricorda uno studio recente, le assicurazioni consentono alle attività economiche di tornare più rapidamente ai livelli precedenti alla calamità. Tassi di copertura elevati e pagamenti rapidi possono quindi attenuare notevolmente i danni economici e possono inoltre ridurre i rischi per la stabilità finanziaria e diminuire il costo per i contribuenti degli aiuti pubblici per coprire le perdite non assicurate. Nonostante tutto questo, l'Unione europea ha dovuto dichiarare come la cultura assicurativa contro il clima sia assai poco diffusa:

i crescenti effetti del cambiamento climatico fanno sì che la copertura sia destinata a ridursi a causa dell'aumento dei premi, che soffoca la domanda, e dal ritiro degli assicuratori da aree particolarmente esposte. Tutto questo rende ancora più difficile un approccio al metodo assicurativo. Il tema naturalmente è al centro dell'attenzione del Governo, che intende promuovere un confronto anche con l'Unione europea, per trovare una soluzione rapida e accessibile a quanti, non solo in Italia, vivono in aree esposte al rischio. Alla fine di questa informativa assai sintetica - e naturalmente, se richiesto, possiamo produrre una relazione analitica - interpretando il pensiero di tutti, lasciatemi rivolgere un sincero apprezzamento alle migliaia di Vigili del fuoco

ai sindaci, ai Presidenti di Regione, agli amministratori e a quanti, in qualsiasi ruolo, si sono dovuti confrontare nelle scorse settimane con una delle stagioni più difficili che, purtroppo, abbia mai registrato la nostra Nazione.

Ho letto gli atti di quella struttura, che ho trovato particolarmente attiva e interessante; molte di quelle competenze,

Sono convinto che un lavoro ancora più analitico consenta di non disperdere quel patrimonio di competenze e anche di capacità e innovazioni normative, ma ogni altra iniziativa che dovesse emergere dal Parlamento non può che dal Governo essere tenuta nella grande e dovuta considerazione, perché il tema riguarda tutti, nessuno escluso. Non è una gara per capire ciò che non è stato fatto nel passato e gli errori che si compiono oggi; sarebbe troppo facile. La gara è volta a comprendere quanto e quando si riuscirà a rendere più sicura questa Nazione di fronte al flagello che il clima, ma non solo, ci ci sottopone giorno dopo giorno. Grazie per l'attenzione. Grazie Presidente, colleghi, ringrazio il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, oggi in Aula per questa informativa puntuale e chiara sui recenti eventi calamitosi accaduti in Italia dal 19 luglio in poi. In apertura vorrei rivolgere il mio più profondo cordoglio per le vittime del maltempo in Lombardia e degli incendi in Sicilia *(Applausi)* ed esprimere affettuosa e sentita vicinanza ai loro familiari. Vorrei altresì rivolgere un ringraziamento di cuore agli uomini e alle donne della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, delle Forze dell'ordine, ai volontari, sempre presenti negli ultimi anni nei luoghi delle calamità, e alle Forze armate, pronti sempre ad affrontare l'emergenza con uno spirito di servizio, una dedizione e un amor di Patria che sono e devono essere per noi in quest'Aula un monito e un esempio di senso di responsabilità. Il Ministro nella sua relazione ha suddiviso il suo intervento in due parti: la prima, sulle tempeste di vento e grandine al Nord; la seconda, sugli incendi che hanno colpito il Sud e, *in primis*, la Sicilia. Il maltempo al Nord, com'è noto, ha provocato anche danni economici importanti a cittadini, famiglie e imprese.

Ho chiesto al Governo, come prima sottolineato dal Ministro, il riconoscimento dello stato di emergenza per i Comuni colpiti dal maltempo al Nord, tra cui il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, il il Trentino-Alto Adige e i primi sostegni economici per cittadini, famiglie e imprese, oltre al riconoscimento dello stato di calamità per il mondo dell'agricoltura, visti gli ingenti danni subiti dalle imprese agricole in quei territori. Al Sud abbiamo registrato una situazione speculare, che ha destato molta preoccupazione con gli aumenti *record* delle temperature e, di conseguenza, degli incendi. Su questo fronte bisogna fare un altro ragionamento: gli incendi purtroppo non sono stati spontanei, ma per la maggior parte dolosi. A mio avviso, dobbiamo, A mio avviso, dobbiamo, da un lato, rendere più severe le sanzioni contro chi provoca danni all'ambiente e al nostro patrimonio naturalistico e, dall'altro, investire di più sulla prevenzione, sulle risorse umane, oltre che sulle nuove tecnologie applicate alla alla prevenzione, tipo i droni, le telecamere e i sensori. Il mese di giugno 2023 è stato a livello mondiale il più caldo di sempre. Lo scorso anno in Europa a causa delle alte temperature ci sono state 60.000 vittime, di cui 18.000 solo in Italia, il Paese più colpito del vecchio Continente. Grazie a tutti di maltempo, ma di cambiamento climatico, come appunto abbiamo detto. La tropicalizzazione è un fenomeno globale che è arrivato circa dieci anni fa e che riguarda tutto il pianeta. Il cambiamento climatico è una minaccia per la salute pubblica, ma aggiungo anche per il tessuto economico e sociale, visti gli effetti dirompenti che le calamità naturali hanno su famiglie e imprese. Per noi la linea della scienza è l'unica che si può e si deve perseguire. Non può e non deve esserci alcun negazionismo, perché, come ha detto il presidente Mattarella pochi giorni fa, discutere di certi temi non ha senso ed è surreale. Questo Governo e questa maggioranza si sono sempre contraddistinti per il fare: le parole chiave sono «programmazione» e «*governance*». Serve programmare, realizzare le vasche di laminazione, la messa in sicurezza dei fiumi e gli invasi per raccogliere l'acqua piovana (di cui riusciamo a trattenere solo il 10 per cento) e fare manutenzione alla rete idrica (perdiamo il 40 per cento dell'acqua dei nostri acquedotti), così come serve una regia coordinata e integrata, ovvero un sistema di *governance* nazionale, che deve indicare le priorità di intervento in ciascun ambito territoriale. È urgente oggi una *road map* di azioni contro il cambiamento climatico e non è solo un problema di risorse: l'Italia sconta un ritardo, come ha evidenziato ancora una volta il Capo dello Stato qualche giorno fa. Contro i cambiamenti climatici... …in una sostenibilità ambientale a 360 gradi, ma anche economica e sociale. È il momento di fare, che è il verbo che conoscono questo Governo e questa maggioranza. Per queste ragioni, come Gruppo UDC-Civici d'Italia-Coraggio Italia-MAIE, valutiamo positivamente l'informativa del ministro Musumeci.

ai ringraziamenti, in particolare ai Vigili del fuoco, ma anche - come ha ricordato anche lei - a tutti i volontari che combattono contro quelli che in tutta evidenza non sono più fenomeni eccezionali, eccezionali, ma la diretta conseguenza però di una gigantesca rimozione o perlomeno di una gigantesca sottovalutazione. Purtroppo, questo è il punto: ci ritroviamo qui sempre più spesso a esprimere cordoglio, contare i danni e manifestare una solidarietà che spesso è tardiva, se non ipocrita. Questo disastro con il quale ci confrontiamo, fatto di alluvioni, frane, smottamenti, siccità e incendi, non si è certamente determinato per caso. Lei dice che qui non ci sono negazionisti, ma, Ministro. glielo voglio dire con nettezza: la maggioranza politica di cui lei è espressione - e con essa, purtroppo, anche una parte significativa del sistema di informazione nel nostro Paese per lungo tempo ha per lo meno ridimensionato, se non apertamente negato, che fosse in atto una drammatica emergenza legata ai cambiamenti climatici e continua a farlo ancora oggi. Ancora oggi, invece di riconoscere questa clamorosa sottovalutazione del pericolo e quindi di cambiare radicalmente e urgentemente rotta, la sua maggioranza punta il dito non

che fa caldo come sempre in estate. Lei capisce, Ministro, che queste dichiarazioni sono totalmente imbarazzanti e irresponsabili? *(Applausi)*. State costruendo una narrazione strumentale e propagandistica, secondo la quale la transizione ecologica sarebbe impossibile perché socialmente ingestibile, quando è vero esattamente il contrario, cioè che, senza un impegno straordinario in quella direzione, anche le conseguenze sociali dei cambiamenti climatici diventeranno sempre più drammatiche. Lei stesso ha detto recentemente (anche oggi) di accelerare sul piano nazionale di adattamento ai

inderogabilità di due provvedimenti che sono fermi al palo da un sacco di tempo: la legge sul clima e la legge contro il consumo di suolo. Inoltre, non credo sia più rinviabile una presa d'atto

che non sia più rinviabile la tassazione degli extraprofitti delle società energetiche e anche questo noi di AVS lo chiediamo in vano da mesi. Il punto è che, senza una visione organica improntata effettivamente all'adeguamento del Paese agli effetti del cambiamento climatico, davvero non si farà nessun passo in avanti. Occorrerebbe invece un piano unico, capace da una parte di contrastare gli impatti causati dagli incendi, dalle alluvioni, dalle frane e, dall'altra, di costruire un'ottica di prevenzione capace di ridurre le emissioni, che sono evidentemente la causa principale

In dieci anni, dal 2010 al 2020, in Sicilia sono andati a fuoco 237.000 ettari,

Lei dovrebbe conoscere perfettamente la situazione: siamo dinanzi a un vero e proprio cataclisma infrastrutturale, dovuto non soltanto purtroppo alla crisi climatica, ma anche ad anni e anni di errori, di sottovalutazioni e di scelte completamente insufficienti. Qui nessuno minimizza le mani criminali che certamente ci sono, in particolare sui roghi, ma queste emergenze si dovevano in qualche modo prevedere, anche per mettere le squadre operative nella condizione di affrontare nel modo più efficace il disastro. Concludo davvero il ricordandole che purtroppo in questi anni è mancata una programmazione, in particolare sulla prevenzione, ma sono stati fatti anche errori di carattere politico generale...

vi pare possibile - lo chiedo al Parlamento e anche al Paese - che in questo contesto e in questo disastro si possa davvero parlare del Ponte sullo Stretto di Messina?

non può vestire i panni del rappresentante del Governo che tenta di scaricare sull'amministrazione regionale le responsabilità delle azioni di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi *(Applausi)*, perché questa responsabilità, Ministro, è stata sua fino a settembre 2022, cioè fino a meno di un anno fa. I dati, quelli che lei ovviamente non cita, parlano chiaro: la Sicilia è maglia nera in Italia sia per numero di reati accertati - ben mille nel 2021 relativi agli incendi boschivi - sia per gli ettari attraversati dalle fiamme, 81.000, che costituiscono quasi il 51 per cento delle nonché per aggressione delle aree protette, anche qui il 51 per cento delle aree nazionali. La matrice criminale e criminogena di questi fenomeni, che sfrutta i periodi estivi per aggredire porzioni del territorio, è ormai un fatto noto, acclarato, innanzi al quale, però, non ricordo un solo intervento da parte del suo Governo regionale negli anni passati e per il quale oggi, francamente, non possiamo accettare la sua mestizia, che ci appare come una mera espressione di circostanza alla quale non ha fatto seguito alcun impegno concreto. Attribuire la responsabilità degli incendi in Sicilia al cambiamento climatico e alle alte temperature, che superando i 46 gradi seccano la vegetazione e l'avviano verso la combustione, come dice nella sua informativa, è un modo per nascondere le gravi carenze politiche e la mancanza delle risorse necessarie a contrastare i fenomeni incendiari. Cinque giorni di incendi in Sicilia hanno causato 60 milioni di danni diretti e 200 milioni di danni alla filiera agricola, senza parlare dei *blackout* di intere aree rimaste senza luce e senza acqua, compresa la sua Catania e compreso anche Palazzo d'Orléans, la sede della Presidenza della Regione Siciliana, che per un'intera giornata è rimasto isolato e senza luce perché non c'erano neanche i gruppi elettrogeni che potessero sopperire alla mancanza Sul suo tavolo, Ministro, il Presidente della Regione Siciliana ha già presentato la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza, per il quale mi auguro che il Governo si adoperi prontamente e seriamente, però i danni subiti non sono certamente soltanto quelli economici, perché, quando bruciano un intero villaggio e un'intera porzione di territorio, non bruciano soltanto le cose, ma i ricordi delle persone, i beni, le attività economiche e i sacrifici fatti per costruirle e questi sono danni che nessuna nessuna risorsa e nessun ristoro economico potrà riparare. In questo frangente, così drammatico, mi chiedo con quali mezzi la Protezione civile abbia affrontato l'emergenza. Al di là di quello che lei ci ha raccontato,

una sola industria che li realizza, come se il monopolio impedisse l'acquisto dei mezzi per l'implementazione della flotta, una teoria nuovissima che non avevo mai sentito da nessuna parte). *(Applausi)* Perché? Dov'erano Perché? Dov'erano i mezzi di terra? Dov'erano le autobotti che avrebbero dovuto raggiungere i posti dove c'era l'incendio prima che il vento propagasse le fiamme, prima che il fuoco avvolgesse i locali, gli immobili e le case e prima che tre persone, nel palermitano, morissero nel fuoco delle loro abitazioni, dato che i Vigili del fuoco non sono riusciti a

di cui era stato programmato l'acquisto, forse prossimamente ne verranno consegnate 12, a seguito di una gara lunghissima, pubblicata nel 2020, e con un contratto che è stato siglato soltanto il 29 dicembre 2022. Impieghiamo due anni soltanto per comprare le autobotti e parliamo di affrontare l'emergenza. Non parliamo poi dei droni: pare che li abbiamo acquistati con una tecnologia non adeguata e quindi non possono essere utilizzati. La Regione Calabria, però, fa una bella campagna di informazione e ci dimostra che con i droni sono riusciti anche a individuare due inneschi dolosi e a prevenire il fuoco prima che si propagasse, ma in Sicilia questa questa cosa non può funzionare. Presidente, mi avvio a chiudere, però una cosa la voglio dire: il ministro Musumeci ci parla di cultura del rischio e ci dice che non siamo abituati... finisco davvero, ma è una cosa brevissima. Non siamo abituati alla cultura del rischio; facciamo le esercitazioni, ma forse le facciamo più per coreografia che non per il fatto che ci crediamo davvero. Forse non tutta l'Assemblea ricorda che, appena un mese fa, in Sicilia avete lanciato la campagna IT-Alert, ossia è stato diffuso un messaggio di testo dalla Protezione civile con un avviso sonoro che serviva da esercitazione per dimostrare che, a fronte di un grande evento calamitoso, la Protezione civile sarebbe in grado di avvisare in tempo reale tutta la popolazione. Questo *test* l'avete lanciato il 5 luglio in tutta la Sicilia e all'esito della sua dimostrazione pratica il direttore generale del Dipartimento di protezione civile della Sicilia, ingegner Cocina, ha dichiarato: «Possiamo affermare che il *test* di IT-Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale di Protezione civile,

che sistema di Protezione civile è quello nel quale si dispone di una tecnologia del genere, che dite che ha funzionato, però poi nel villaggio delle Masse a Messina il parroco alle due di notte ha dovuto dare l'allarme con le campane della chiesa per far fuggire la popolazione dalle case? *(Applausi)*. Questo è il vostro sistema!

su una cosa, signor Ministro, noi siamo d'accordo con lei: sullo stringerci intorno alle famiglie delle vittime di questi ultimi eventi intorno alla fatica, rappresentata in quella immagine evocativa pubblicata sui giornali, dei Vigili del fuoco, della Protezione civile, che è un fiore all'occhiello del nostro Paese, e dei sindaci, che spesso soli, solissimi, affrontano situazioni gravissime.

E nel cercare di riempire questo vuoto, al Ministro quella che evidentemente per questo Governo non è una funzione centrale e cioè la Protezione civile. Signor Ministro, siamo il Paese della Protezione civile di Zamberletti,

Vedere che un Governo, per riempire di significato qualcosa che non lo ha, utilizza una delle funzioni che dovrebbero essere più trasversali e più guidate

oggi ha faticato ad argomentare come il nostro Paese deve affrontare il tema del cambiamento climatico. Insieme a questo, c'è una cultura imperante imperante dentro la destra ed è inutile negarlo: è la cultura di chi nega che i cambiamenti climatici siano obiettivamente un problema. Lei non è tra questi ed io ovviamente le do atto di tutto ciò, però il problema esiste all'interno di questo Governo. Siamo un Paese a forte rischio, a forte rischio, non soltanto per l'aumento del caldo: pensate a quello che sta avvenendo nel nostro mare; ci sono studi che indicano - e credo che per lei ieri fosse il giorno limite per presentare il piano sul mare piano sul mare - un innalzamento del mare di 40 centimetri, in alcuni casi anche di un metro. Sono proprio i mari i luoghi dove si formano, a causa del surriscaldamento, le celle cosiddette autorigeneranti, le celle temporalesche che spesso determinano problemi nelle nostre città. A questo ovviamente dobbiamo porre rimedio, cercando di avere sul tema dell'ambiente una strategia più convincente, seria e di lungo periodo. Bisogna però anche dire con grande franchezza, signor Ministro, che ci sono problemi non risolvibili, se non attraverso la realizzazione di infrastrutture e di opere che siano in grado di mettere in sicurezza il nostro entroterra e le nostre città. Sono gli argini, sono le briglie, sono gli scolmatori, sono le casse di espansione. In questo Paese - lei lo ha ricordato, ma ancora una volta senza andare a fondo delle questioni - c'è stato un solo momento in cui si è pensato a una strategia complessiva per per dotare le nostre città e il nostro territorio di un piano serio e duraturo sulla questione del cambiamento climatico e del dissesto idrogeologico. Sto parlando del piano Italia sicura. *(Applausi)*. Che cos'era il piano Italia sicura? Una strategia 1.445 cantieri aperti, 500 milioni a Genova (dove le opere sono ancora in corso, per cui il Bisagno finalmente sarà in sicurezza tra pochi anni), 120 milioni in Toscana per quattro casse di espansione sull'Arno e poi tanti altri interventi in città metropolitane. Il piano Italia sicura non doveva essere cancellato *(Applausi)* ed è una grande responsabilità che portano in carico gli esponenti del MoVimento 5 Stelle e della Lega, che lei non ha citato. Quel piano doveva essere ancora oggi in corso e dare compiutezza alle necessità del Paese.

a firma Renzi-Paita; chiamatela come ritenete, ma date a questo Paese una

è come intende affrontare il tema della deforestazione e il problema che abbiamo nell'entroterra. Signor Ministro, sappiamo che su questa partita - e chiudo davvero - c'è bisogno di un'azione unitaria...

chiesto la deliberazione dello stato di calamità e di emergenza anche per la Sicilia. Gliel'ho detto lo stesso giorno e mi sento in dovere di ripeterglielo oggi per il suo impegno e per il suo lavoro sempre certosino. L'informativa odierna - lo sappiamo - è la fotografia di un Paese fragile. Il nostro, uno dei territori più belli al mondo, sembra oggi essere soggetto ai capricci delle stagioni e degli eventi meteorologici.

cui è fondamentale organizzare gli interventi contro il dissesto idrogeologico e per una più puntuale gestione delle acque. Al Sud invece il problema principale dagli incendi boschivi estivi: una maggiore prevenzione può evitare che gli incendi vengano appiccati e si propaghino con estrema facilità. Nessuno - e lei poc'anzi lo ha ribadito - può convincerci che gli incendi di questi giorni in Sicilia siano stati per autocombustione o per incuria dell'uomo. Non è così. Sono incendi accesi, Ministro, o fatti accendere da chi ha un interesse. Siamo d'accordo con lei: si tratta di interessi di chi pensa di recuperare qualche ettaro di pascolo in più, altre volte quei roghi sottendono più sofisticate idee di speculazione edilizia. Il danno, però, non solo ambientale che un incendio boschivo causa al territorio è davvero enorme. Ci sono zone montuose in cui gli incendi sono raggiungibili solo dagli aerei e dai 6.000 litri di acqua scaricata dai loro serbatoi. È vero serve aumentare il numero dei Canadair, ma è anche vero che un Canadair costa circa 25 milioni di euro e un'ora di volo circa 6.000 euro. Bisogna organizzare, oltre alla flotta aerea, gli equipaggi, le basi operative, la copertura delle operazioni di volo su tutto il territorio. Ma è anche vero che il resto del territorio costa molto meno, perché si può adottare una puntuale opera di prevenzione.

vicini a tutte quelle famiglie, soprattutto della mia Provincia, Siracusa, Ministro, che lei conosce benissimo. A Melilli, oltre a perdere ettari di terreni agricoli, hanno perso bestiame e foraggio; intere famiglie sono senza casa. I danni, quindi, subiti sono economici e ambientali. A Siracusa un'azienda vinicola è andata in fumo; a Marzamemi case completamente distrutte e gente che si è ritrovata senza nulla in mano in un nanosecondo. Ministro, sono certa del suo impegno. Per evitare danni futuri bisogna adottare le più innovative tecniche di osservazione satellitare che danno un monitoraggio molto puntuale. Intervenire per spegnere un incendio dopo quindici minuti è molto più semplice che spegnere un incendio che già ha bruciato ettari. Signor Ministro, lei è a capo del Ministero delle emergenze e della Protezione civile e conosce molto meglio di chiunque noi qui dentro questi temi. Pensiamo che ci sia un grande lavoro da fare per passare dalla fase dell'emergenza a quella della protezione del territorio e poi della programmazione. Noi la ringraziamo per l'impegno che ci sta mettendo e le auguriamo buon lavoro.

Ministro, l'ultima volta che le ho dedicato un mio intervento eravamo in Parlamento siciliano, io deputata regionale e lei Presidente della Regione. Dico questo per dire che io e i siciliani la conosciamo bene, Ministro. Conosciamo bene il suo modo di fare politica, anzi di non fare politica, di non governare i processi che attengono alla politica. E conosciamo bene anche la sua storia politica, di come abbia barattato la Sicilia per un posto qui in Parlamento.

sul buon governo della Regione, sull'opportunità, anzi la necessità di avere lui l'opportunità di essere ricandidato a Presidente della Regione per raccogliere i frutti del suo Governo. Il suo stesso partito, però, gli ha detto che nessuno lo voleva e che quindi non poteva ricandidarsi a Presidente della Regione. Allora, per eliminare l'imbarazzo,

Presidente, ho letto nelle dichiarazioni del ministro Musumeci una rassegnata presa d'atto di cosa manca in Sicilia; di cosa non si è fatto in Sicilia; di cosa bisognerebbe fare in Sicilia. Signor Presidente, è come se il ministro Musumeci non fosse stato Presidente dei siciliani. Invece lo è stato, fino all'altro ieri: Presidente da novembre 2017 a ottobre 2022. Cinque anni! Cinque anni per non fare nulla: zero prevenzione contro gli incendi, zero politiche di sviluppo aeroportuali, zero politiche ambientali. E che dire poi del fatto che nel 2018 egli è stato nominato Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti. Tra le sue responsabilità c'era anche la discarica di Bellolampo. L'allora Presidente doveva completare la settima vasca, assolutamente necessario perché la quarta, quella che oggi brucia e regala diossina ai residenti della Sicilia e ai palermitani, era già esausta.

Il ministro Calderoli diceva l'altro giorno in Commissione bilancio - i commissari presenti lo ricorderanno - che, se i Presidenti delle Regioni non riescono a spendere le risorse per realizzare le opere e le infrastrutture necessarie per i territori, devono prendersene la responsabilità. È cambiato registro:

sulla quale è legittimo avere opinioni controverse, ma non è legittimo parlarne ora.

Ebbene, che dire anche dei soldi non spesi? Ma andiamo avanti. Signor Presidente, è un Ministro che si è permesso anche di offendere gli amministratori delle zone alluvionate, asserendo che lo Stato non può essere considerato come un bancomat e che le responsabilità - come qualcuno di Fratelli d'Italia diceva l'altro giorno in quest'Aula

che è facilissimo risolvere il problema. Bene: perché non l'ha fatto quando era Presidente della Regione? Colleghi, il ministro Musumeci prima è stato nominato Ministro per il Sud, poi delle politiche del mare, ma senza le deleghe ai porti e poi, alla fine, della protezione civile: quasi che si cercasse di ricompensarlo per qualche servigio, cercando però anche di dargli una delega che non facesse tanti danni. Ma i danni li ha fatti. Li ha fatti quando era Presidente della Regione

La senatrice Damante ha potuto esprimere fino in fondo, senza disturbo, il suo intervento.

non interviene un senatore siciliano, ma interviene un senatore lombardo per ricordare ai colleghi senatori, e soprattutto ai cittadini che ci stanno ascoltando, che il problema del cambiamento climatico non è solo della Sicilia, cari colleghi, ma riguarda tutto il Paese, dal Brennero a Lampedusa.

prima di entrare nel merito del mio intervento, voglio ringraziare senza retorica, ma con vero animo grato, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, la Guardia costiera, i militari e le Forze di polizia *(Applausi)*, per il lavoro che li vede impegnati da Nord a Sud del Paese, per fronteggiare le emergenze, soccorrere e mettere in sicurezza i cittadini. Sono loro che rappresentano in prima linea lo Stato e a loro dobbiamo assicurare tutto il nostro sostegno. Così come abbiamo il dovere di garantire la vicinanza e la collaborazione di Governo e Parlamento ai sindaci e ai Presidenti di Regione, di tutti i colori politici, che vedono colpiti sempre più spesso i relativi territori dalle calamità e dall'azione degli incendiari. Signor Ministro, il Governo faccia tutto il possibile per assicurare il ripristino dei servizi ai cittadini, la riparazione dei danni e il ristoro alle attività economiche e ai lavoratori colpiti. Fin qui, però, si tratta ancora una volta di gestire l'emergenza. È un'attività nella quale il nostro Paese si è spesso distinto e anche stavolta dobbiamo svolgerla al meglio, ma non possiamo abituarci a questo. Siamo bravi a gestire l'emergenza, ma non possiamo solo gestire l'emergenza. Signor Ministro, vedo che annuisce e, quindi, è d'accordo con me. Che si tratti di siccità, bombe d'acqua, grandine, incendi, terremoti, che c'entri il cambiamento climatico o l'azione di criminali e piromani - vanno trovati e puniti, per dare un esempio *(Applausi)* e per far capire agli italiani che certe cose non si fanno o che siano sciagure imprevedibili, nessuno di noi può sentirsi incolpevole, perché arriviamo tardi, tutti: la politica, la società, la stampa e le imprese. Arriviamo tardi nel mettere al centro dell'attenzione della nostra azione la cura del territorio. Il territorio italiano è fragile, troppo fragile, e non l'abbiamo saputo gestire guardando al futuro. Abbiamo sempre guardato al presente, a risolvere i problemi, ma non abbiamo mai guardato a quello che può succedere in futuro. È questo il cambio di passo che dobbiamo fare e che - va dato atto al Governo - abbiamo iniziato a fare, ma non basta. È tempo finalmente di realizzare le opere necessarie per limitare i disastri e i danni del dissesto idrogeologico, per migliorare la raccolta e l'approvvigionamento dell'acqua, per migliorare la resistenza degli edifici ai terremoti, per difendere i boschi dagli incendi. Fare e non fermare. Abbiamo rinviato troppo a lungo, anche per dare retta agli ambientalisti del solo e del semplice no. Per anni abbiamo sentito gente dire di no, che non si può fare, non si può fare, e non si può fare. Adesso ci vengono a dire che forse bisognava fare qualcosa, oppure ci dicono che adesso dobbiamo fare qualcosa. Per settanta anni, sentiti dire che non si potevano fare certe cose. *(Applausi)*. Ora, signor Ministro e signor Presidente, deve farsi avanti l'Italia del sì, quella che investe nel potenziamento delle infrastrutture idriche - la siccità dell'anno scorso ce la ricordiamo ancora - nel rafforzamento del Mose, nella diga di Genova; quella quella che, anche grazie al nuovo codice degli appalti, può accelerare le opere di cura del territorio; quella che mette mano al PNRR, per far sì che gli interventi contro il dissesto idrogeologico possano essere realizzati sul serio, anche rimodulandoli, per evitare che restino solo sulla carta. Ma ne parleremo dopo, con il ministro Fitto. Signor Presidente, prima di concludere, voglio rivolgere al Governo un ultimo invito: fra i tanti a pagare le conseguenze e i danni di questi fenomeni estremi, c'è la categoria degli agricoltori, degli agricoltori, che sono la prima avanguardia nella cura del territorio. Questa Assemblea ha votato il riconoscimento dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, forse all'unanimità. Sono anche, sul piano economico, le prime vittime dei disastri provocati dall'emergenza climatica. Aiutiamoli a proteggersi e a proteggerci. Le polizze assicurative in questo settore sono ancora troppo poco diffuse e, grazie anche ai vincoli europei, quando ci sono coprono solo i danni provocati da fenomeni estremi. estremi. Noi pensiamo che dobbiamo valutare una forma di agevolazione che li aiuti a stipulare polizze con una copertura più ampia, perché ormai i fenomeni climatici fuori controllo sono diventati la normalità. Signor Presidente, nella nostra azione di Governo dobbiamo anche garantire a tutti i Comuni il sostegno pieno per la ricostruzione e il mantenimento dei servizi. Pensiamo solo alle scuole di tutti i Comuni delle Regioni interessate da fenomeni drammatici, in particolare al Nord del nostro Paese: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Regioni che non ho ancora sentito nominare. eventi calamitosi di pochi minuti che però rischiano di bloccare servizi essenziali che spesso sono sulle spalle di sindaci e amministratori locali, che troppe volte si sono ritrovati da soli. Monitori e aiuti il Governo coloro che sono davvero in difficoltà. Concludo, Presidente, con la speranza che tutto il Parlamento si ritrovi in queste parole. Nei prossimi anni la sfida della sicurezza del territorio deve essere una priorità, perché certamente non possiamo controllare gli effetti immediati del cambiamento climatico, ma altrettanto certamente possiamo fare molto di più per proteggere i cittadini e le imprese. Se questa è una sfida di tutti, mettiamo da parte le ideologie e gli integralismi. Portiamo avanti le opere che servono tutti insieme perché, se il Governo ha un colore politico, Presidenti di Regione e sindaci e sindaci possono averne un altro e loro sanno cosa c'è da fare. Mi auguro che anche i loro compagni di partito a Roma sappiano ascoltarli e non vogliano agitare la bandierina del clima solo per racimolare qualche voto tra chi imbratta monumenti o blocca il traffico per protesta.

credo nella separazione dei poteri, credo nel valore del potere esecutivo, ma altrettanto nel valore del potere legislativo. E penso che lei, come Presidente del Senato, debba tutelare i senatori e un po' meno gli interventi che fa il Governo.

di utilizzare forse il lessico più appropriato. Non siamo infatti di fronte al maltempo o - lo dico anche ai colleghi - al cambiamento climatico: è una crisi climatica e dovremmo imparare a utilizzare i termini giusti.

ci ha detto che non dovremmo preoccuparci, perché abbiamo una *Premier* che ha deciso di mettere la lotta contro il cambiamento climatico al primo posto dell'agenda. L'ha detto qui, ma evidentemente quando fa i comizi in Spagna se ne dimentica e urla e strepita rispetto a provare a fermare - cito - il fanatismo ultraecologista. *(Applausi)*. Poi ci spiegherà che cosa è il fanatismo ultraecologista. Come capirà dal mio accento, come il collega Centinaio non sono siciliana, sono lombarda. E le dico che mi dispiace che, mentre noi del Partito Democratico ci vogliamo occupare

in quei giorni - e ci ha fatto un elenco di quali sono stati gli eventi climatici estremi. Il suo compito dovrebbe essere un altro, e se lo aspettano anche gli italiani: quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, ma quello che a noi interessa è sapere cosa intendete fare ora - cosa che lei non ha detto - restando abbastanza vago. D'altra parte, sappiamo che siete abituati a fare questo. Ci chiedete l'unità e di affrontare i problemi in maniera unitaria - cosa che noi vogliamo fare - ma poi voi ne approfittate sempre per fare battaglia politica. È fresca quella che avete fatto, purtroppo, sulla pelle degli emiliano-romagnoli, che ancora stanno aspettando i sette miliardi che mancano. *(Applausi)*. Avete fatto perdere tantissimo tempo per la nomina del commissario, perché eravate interessati a una battaglia politica e anche a fini elettorali, ma parleremo anche di questo. Torniamo al tema del lessico e delle parole da utilizzare. Lei parla di messa in sicurezza del territorio, ma glielo diamo un nome? Parliamo di un piano e di un quadro vero sul clima. Parliamo di un piano di manutenzione straordinaria del territorio. Vogliamo parlare di una cabina di regia nazionale che funzioni, che coinvolga enti locali e Regioni, di una legge sul consumo di suolo zero? No, Ministro, non ne parliamo, perché per ora sappiamo solo che il vostro interesse, rispetto alla tutela del territorio, è quello che avete manifestato tagliando 16 miliardi dai progetti del PNRR destinati alla gestione dei rischi. *(Applausi)*. Ne parleremo dopo con il ministro e speriamo che possa essere meno vago e che abbia, almeno lui, rispetto del Parlamento. Il Parlamento anche in questo caso è arrivato dopo. Vogliamo sapere cosa farete per il Friuli-Venezia

giorni per accogliere una mozione per destinare risorse agli aiuti rispetto ai danni registrati. Siete capaci di fare ostruzionismo anche su quello, proprio perché non avete assolutamente volontà di lavorare insieme. Rispetto alla Sicilia, a cui lei

che nelle ultime settimane hanno attraversato l'intera Nazione. Paradossalmente mi sono trovato in Friuli sotto le grandinate e poi sono arrivato in Sicilia e ho visto gli incendi nella mia amata Palermo,

che ha cercato di delineare lo stato dei fatti in quei tragici giorni in cui si sono accavallate due emergenze diverse ma altrettanto drammatiche: quella del maltempo al Nord, su cui il Ministro è ampiamente intervenuto, e quella altrettanto drammatica ma differente degli incendi al Sud.

acquistare un assetto aereo significa investire su qualcosa che si produce nell'arco di quattro anni; se qualcuno studiasse - come penso che tutti noi facciamo - sicuramente saprebbe che la Canadair non produce gli aerei CL-415 da qualche anno;

a fare un processo a un Ministro per il ruolo da lui ricoperto in un'altra fase della sua vita, laddove non mi sembra che nessuno in questa sede

quando c'è un incendio, non discutono, ma si uniscono e vanno a spegnerlo. Quando la casa brucia non si discute: si spegne l'incendio; quando c'è un'alluvione, si corre a salvare le colture, le auto e le strade.

intendiamo lavorare per il futuro. Signor Ministro, lei ha parlato di una gara. Noi non partecipiamo alla gara di chi è stato più bravo prima o dopo. Amiamo partecipare tutti assieme alla gara per portare avanti l'Italia e sono sicuro che insieme a lei la vinceremo.

del Senato stigmatizzi le parole del ministro Crosetto per proteggere le fondamentali prerogative del Parlamento.

nell'ambito di un proposta approvata dalla cabina di regia la scorsa settimana e già inviata in Parlamento, che affronta le questioni collegate alla rimodulazione e alle modifiche del Piano nazionale di ripresa e resilienza e a una indicazione precisa delle proposte di modifica relative alla quarta rata. Preliminarmente penso sia importante fare una considerazione sulla terza rata per poter avere un quadro d'insieme del lavoro fatto e soprattutto per poter illustrare i contenuti del lavoro che il Governo sta portando avanti rispetto alla questione al nostro esame. È necessario e importante farlo partendo da una considerazione, che in altre circostanze ho avuto modo di sottolineare, relativa al fatto che, dalla terza rata in poi, il percorso e l'approccio sul tema dell'avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza cambiano per due ragioni: innanzi tutto per una ragione collegata al numero degli obiettivi che aumentano rispetto alle rate e, in secondo luogo, perché per la prima volta, dopo le prime due rate, si interviene sulla valutazione della fisicità degli interventi, e quindi si inizia a verificare quello che accade realmente rispetto al tema degli investimenti e della spesa. Questo ha comportato un lavoro molto complesso - com'è noto - rispetto alla valutazione e al raggiungimento degli obiettivi relativi alla terza rata,

hanno previsto, anche alla luce dell'insediamento del Governo ad ottobre dello scorso anno, la possibilità di intervenire successivamente in fase di verifica (il cosiddetto *assessment*); il che è avvenuto dal mese di gennaio in poi. In questa direzione abbiamo avuto modo di intervenire per raggiungere questo risultato, anche alla luce delle difficoltà oggettive che sono emerse rispetto al tema della valutazione e dei criteri che, proprio perché sono intervenuti gli elementi relativi alla fisicità degli interventi, hanno portato

un gruppo di interventi dentro una misura e verificarne lo stato di avanzamento e attuazione. Questo chiaramente ha reso molto articolati il lavoro e il confronto, a tal punto che il Governo è è dovuto intervenire con 47 modifiche legislative e amministrative rispetto ai vari obiettivi della terza rata. È importante sottolineare ciò, perché dentro tali modifiche ci sono sicuramente degli interventi di carattere legislativo che hanno visto il Governo dover modificare, correggere, integrare, nel confronto con la Commissione europea, alcune delle indicazioni previste all'interno dei cinquantacinque obiettivi, per quanto riguarda sia i trenta obiettivi che che ci siamo trovati di fronte all'insediamento del Governo, sia i venticinque obiettivi che si consideravano raggiunti ma che invece hanno avuto la necessità di alcuni elementi di integrazione. Farò degli esempi specifici anche su questo per poter individuare in modo puntuale le questioni di cui ci occupiamo. È evidente che, in tale contesto, c'è un'altra valutazione da fare rispetto all'avanzamento delle rate. Se per la prima rata ci troviamo di fronte a due *target* e 49 *milestone*, per la seconda rata un *target* e 44 *milestone*, per quanto riguarda sono diventati 16 e le *milestone* sono 39. Questo dato indica in modo molto chiaro anche le modalità di approccio ed è alla base dell'analisi relativa non solo alla terza e alla quarta rata, ma anche e soprattutto alle proposte di modifica complessive che il Governo ha approvato in cabina di regia e che saranno oggetto di una proposta, come ho sottolineato in più circostanze. È utile ricordare che si tratta di una proposta sulla quale aprire il perché è necessario sottolineare che all'interno di tale proposta emerge una serie di valutazioni che guardano non alla scadenza immediata, ma complessivamente alla scadenza finale del Piano. È quindi evidente che il nostro obiettivo è individuare delle soluzioni che facciano emergere e superino delle criticità di vario genere del lavoro che ci porterà dalla valutazione degli obiettivi della quinta rata fino alla decima rata, cioè fino a giugno 2026. è l'obiettivo che il Governo ha messo in campo per avere un quadro d'insieme sul quale fare riferimento e soprattutto per individuare anche gli obiettivi che vanno di pari passo, collegati non solamente agli investimenti ma anche alle riforme. Questo penso sia importante importante sottolinearlo, perché diverse riforme sono state e sono oggetto di interventi molto complessi. Ne cito una solamente perché penso che sia la più complessa e la più importante: mi riferisco in modo particolare alla legge annuale per il mercato della concorrenza, che anche a livello europeo è stata definita la più complessa fra tutte le riforme degli Stati membri. Questo penso rappresenti anche una dimensione alta rispetto alla sfida che abbiamo di fronte. Così come penso che sia altrettanto importante citare alcuni degli aspetti collegati: dalle concessioni portuali alla riforma dell'energia elettrica, agli oneri di sistema in bolletta elettrica, ai servizi idrici integrati, al teleriscaldamento, ai piani urbani integrati. Questo solo per citare alcuni degli obiettivi sui quali il Governo è intervenuto rispetto al raggiungimento della terza terza rata. Da questo confronto che si è sviluppato con la Commissione europea è emersa - come è noto - in modo particolare una criticità. Anche qui, questa mattina alla Camera ed in generale si è discusso molto al riguardo. Il Governo ha individuato, nel confronto positivo con la Commissione europea, una soluzione al problema. Lo voglio dire perché il tema degli studentati e dei posti letto per gli studenti non riguarda non riguarda in modo specifico l'azione immediata del Governo, visto che è concentrato nella terza rata. Ma ha visto il Governo lavorare d'intesa con la Commissione europea per evitare quello che più volte abbiamo letto sui giornali e che qualcuno immaginava qualcuno immaginava o individuava come un elemento di polemica politica. Mi riferisco al non raggiungimento dell'obiettivo e, quindi, dei pagamenti parziali delle rate. Per evitare questo, il Governo ha aperto, sulla base dell'esperienza della terza rata, un lavoro e un confronto con la Commissione europea che ha portato allo spostamento obiettivo, esattamente quello degli studentati. Abbiamo definito - e mi fa piacere che oggi sia qui con me proprio il ministro Bernini, che ha lavorato in modo assolutamente

della terza rata, una modifica preliminare, condivisa con la Commissione europea a livello tecnico, che ha individuato i dieci obiettivi da modificare, a cui si è aggiunto aggiunto l'obiettivo degli studentati e dei posti letto. Questo ha consentito di presentare, previ una valutazione e un confronto di carattere tecnico, una modifica complessiva della quarta rata che ci ha consentito di poter avviare preliminarmente un confronto che evitasse quanto è accaduto nella fase di verifica sulla terza rata. Quindi, l'esperienza della terza rata è stata utile per individuare un percorso nuovo nuovo rispetto alla quarta rata ed è fondamentale per tutto ciò che dirò successivamente rispetto all'intero complesso delle modifiche che presentiamo su tutto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, come ho ricordato. È molto positivo - ed esprimo soddisfazione su questo - il fatto che questi obiettivi, che sono stati individuati

corretto alcuni aspetti. Il primo riguarda il fatto che i bandi per gli asili nido sono stati prorogati in diverse circostanze, non consentendo quindi di raggiungere l'obiettivo del giugno del 2023, che era quello dell'assegnazione dell'intera quota di lavori relativi proprio alla realizzazione degli asili nido. Allo stesso modo il Governo si è trovato di fronte a un'interpretazione - e l'interpretazione tornerà molto nel lavoro che stiamo facendo - rispetto alla lettura di quanto previsto all'interno dei bandi. L'interpretazione sugli asili nido, per esempio, ha portato la Commissione europea valutare come nuovi posti quelli relativi a interventi di demolizione e ricostruzione dell'asilo; i nuovi posti sono esclusivamente quelli previsti

per non raggiungere l'obiettivo, ma ha modificato un obiettivo intermedio e, in modo coerente e coordinato, presenta oggi nella proposta di revisione un aumento di risorse, pari a 900 milioni di euro, per mantenere il *target* finale della realizzazione dell'obiettivo del numero dei posti di asili nido. *(Applausi)*. È molto importante chiarire questo, perché ci consente di avere il giusto approccio rispetto alle questioni di cui oggi ci siamo occupando e voglio sottolinearlo anche relativamente a una serie di altri misure sulle quali siamo intervenuti: penso alle infrastrutture sulla ricarica elettrica e alla tecnologia satellitare e all'economia spaziale; penso al progetto di Cinecittà e alla sperimentazione dell'idrogeno per la mobilità delle ferrovie. Potrei fare altri esempi sui quali il lavoro preventivo di intesa ci ha portato a una proposta, che abbiamo in cabina di regia e inviato alla Commissione europea. Così com'è accaduto sulla terza rata, è accaduto anche rispetto alle modifiche della quarta rata, se è vero come è vero che venerdì scorso la Commissione europea ha approvato la nostra proposta di terza rata e le nostre modifiche relativamente alla quarta rata, a condividere l'impostazione per la quale non si perde nemmeno un euro, ma, spostando l'obiettivo (il 55°) dalla terza alla quarta rata,

complessivi della terza e della quarta rata senza alcun ritardo. Credo che questo sia un risultato molto positivo e importante, soprattutto perché sia la terza che la quarta rata non appartengono più propriamente all'azione del nostro

raccontare, ci ha consentito di avere un approccio rispetto al tema della revisione complessiva del Piano che fa di necessità virtù e che

L'approccio che vi è sul PNRR non è quello della rendicontazione ordinaria che abbiamo conosciuto sulle altre risorse europee o sulle risorse nazionali: è un approccio completamente differente, così com'è molto differente il tema dell'ammissibilità dei progetti. C'è un C'è un caso sul quale poi tornerò, che è quello relativo agli stadi di Firenze e di Venezia all'interno dei Piani urbani integrati, che testimoniano concretamente qual è la difficoltà relativa all'ammissibilità degli interventi. Poi c'è il tema del DSNH (*do not significant harm*), che è un aspetto molto importante e rilevante rispetto alla valutazione preliminare degli interventi. questo si inserisce all'interno di una valutazione più generale che è collegata alle modalità di formazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, se è vero - com'è vero - che all'interno del Piano ci sono 67 miliardi di euro di progetti in essere. Da qui dobbiamo partire, perché 67 miliardi di euro di progetti in essere vuol dire che ci sono 67 miliardi di progetti che esistevano già prima della nascita del PNRR, che sono stati ipotizzati e immaginati con logiche e regole completamente differenti e che non hanno in alcun modo fatto i conti con il meccanismo e con il percorso che noi abbiamo conosciuto, ad esempio già sulla terza rata, che è quello di rendicontazione, di ammissibilità e soprattutto - mi dispiace che questo tema spesso nelle dichiarazioni e nelle critiche venga omesso o non considerato - della tempistica. Non dimentichiamo che tutti i progetti, oggetto della rimodulazione che noi proponiamo, hanno una

30 giugno 2026. Per queste ragioni è evidente che la proposta di modifica si imposta su diversi aspetti, il primo dei quali è collegato al numero delle misure che proponiamo di modificare: sono 144 che modifichiamo, rispetto ad una previsione complessiva di 298 misure (63 riforme e 235 tra investimenti e sub-investimenti). Proponiamo di modificare 144 misure con l'obiettivo di mettere in campo delle risoluzioni su diversi aspetti. Il primo aspetto è quello interpretativo e correttivo:

è il motivo per il quale noi abbiamo dovuto recuperare i 900 milioni di euro per fare un nuovo bando e per dare una risposta complessiva e finale rispetto ai numeri e ai dati relativi al raggiungimento dell'obiettivo in questo senso. Questa valutazione ci deve portare a dire che

l'interpretazione e la modifica formale della misura, per evitare di passare nei prossimi mesi o nei prossimi anni ad un confronto non chiaro rispetto a differenti interpretazioni. Questo è un primo aspetto molto importante. La seconda questione relativa alle modifiche riguarda la possibilità, a parità di risorse all'interno della stessa missione, di spostarle su differenti progetti ed è un tema che sarà oggetto del confronto con la Commissione europea. La terza questione riguarda le modalità alternative per raggiungere gli obiettivi, in modo particolare su alcune misure, spostando sempre parte dei progetti, rispetto alla possibilità di avere progetti in grado di mantenere la data del giugno del 2026. La quarta questione, che attiene a nove misure in particolare che sono oggetto del grande dibattito politico che si è nel nostro Paese, riguarda interventi previsti che sono stati finanziati all'interno del PNRR. Da una valutazione specifica (entrerò poi nel merito, illustrando i contenuti delle principali misure oggetto di questa discussione)

poter fare questo ragionamento, anche mettere in campo una riflessione collegata alle priorità di revisione, rispetto al fatto che - lo voglio dire in modo molto chiaro e lo sto ribadendo da giorni - il definanziamento degli interventi si concretizzerà al termine del confronto con la Commissione europea. Sarà quello il momento nel quale andremo a riarticolare il finanziamento di questi interventi con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione,

auspicato e sollecitato dalla Commissione europea nelle sue recenti raccomandazioni, laddove indica agli Stati membri la necessità di rendere complementari le risorse della coesione, insieme alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È importante chiarire tutto ciò perché lo dico in modo chiaro - tutto questo non comporta alcun problema per gli interventi in corso, che proseguiranno regolarmente, così come previsto. Quando sarà terminato il lavoro di verifica, andremo a fare la valutazione e la ricollocazione rispetto agli altri programmi. Qui voglio esprimere alcune parole di chiarezza, perché anche su questo c'è la polemica che accompagna queste scelte.

quello nazionale e quello regionale. Quindi è evidente che stiamo definendo un percorso con le Regioni, in questo periodo - ci tengo a sottolinearlo - che chiarirà questi aspetti, soprattutto su un dato, che cito spesso, ma che spesso viene dimenticato ed omesso. Il dato è relativo allo studio e al lavoro che abbiamo fatto, all'inizio della legislatura, sull'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, risorse europee e nazionali, relativamente alla programmazione 2014-2020, che torneranno nell'analisi delle misure per le quali proporremo lo spostamento del finanziamento. Questo studio e questa verifica ci dimostrano che, a due mesi

che ci troviamo di fronte non al rischio, che viene più volte rappresentato, di intervenire su progetti già finanziati che non possono trovare altra copertura. Ci troviamo invece di fronte ad una valutazione che ci porta a dire che, tanto per le amministrazioni centrali, quanto per le Regioni, esiste la necessità di andare a fare una verifica puntuale sulla percentuale di risorse che sono realmente utilizzate, perché dentro queste risorse e dentro i programmi di intervento, regionali e nazionali, troveremo alcuni interventi - non voglio dire molti: spero che siano alcuni, ma temo che siano molti - che ritroveremo all'interno delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi è necessario andare a fare questo lavoro, per evitare queste sovrapposizioni, per evitare - lo dico anche con riferimento al dibattito precedente, che ho ascoltato nella sua fase conclusiva - di avere, per esempio sul dissesto idrogeologico, una serie di progetti che sempre gli stessi, che vanno in tutte le programmazioni, ma che puntualmente non vengono realizzati. Vorremmo dunque provare a mettere un punto fermo e capire con quali fondi, finalmente, questi interventi verranno realizzati. *(Applausi)*. Questo è il punto dal quale partiamo. Prendo come esempio proprio il tema del dissesto, non prima di aver fatto una valutazione rispetto al tema dei 67 miliardi di euro dei progetti in essere, in essere, siccome in queste ore c'è un grande dibattito sulla necessità di tutelare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nella loro ripartizione, per citare due elementi:

e la coesione e sono stati inseriti all'interno del Piano nazionale di ripresa di resilienza *(Applausi)*. E non ho ascoltato nemmeno alcuna reazione quando il Fondo opere indifferibili, che è stato costituito fino a sei miliardi di euro, è stato preso dal Fondo di sviluppo e coesione e messo per finanziare le opere dell'intero dell'intero Paese. Lo voglio ricordare perché penso che la logica dei due pesi e delle due misure non aiuti la discussione e lo voglio ribadire perché la posizione del Governo è quella di garantire il mantenimento delle percentuali previste all'interno del riparto del Fondo di sviluppo e coesione. Voglio anche ricordare che quando noi parliamo del Fondo di sviluppo e coesione, parliamo dei 49 miliardi da dividere e da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato e le Regioni, per poi parlare dei 43 miliardi di risorse europee della coesione più quelle del cofinanziamento (risorse europee 2021-2027), che sono a loro volta ripartite tra risorse nazionali e risorse regionali. È quindi evidente che che il margine al quale noi facciamo riferimento è ampio, all'interno del quale non mi sembra che ci sia, così come talvolta viene indicato, una copertura totale dei progetti se è vero, come è vero, che noi abbiamo una programmazione

C'è un problema di capacità di spesa che è oggettivo, che i numeri ci consegnano e che nulla ha a che fare con i rischi che vengono oggi immaginati e rilanciati in questa direzione. Faccio questo riferimento perché è utile proprio dall'esperienza maturata avere un approccio collegato alle questioni relative alle modifiche che noi stiamo presentando relativamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza e lo voglio individuare in modo specifico rispetto ai singoli temi oggetto delle proposte di modifica, avendo chiarito, come ho detto, che questo percorso si completerà alla fine del confronto con la Commissione europea e avendo detto con chiarezza che la verifica di queste misure deve fare i conti con alcune criticità. Entriamo nel merito di queste criticità perché penso che sia opportuno parlare con i fatti e non con valutazioni di carattere generale. Passiamo al tema del dissesto idrogeologico; vorrei qui fare alcune riflessioni importanti. è collegata all'elenco degli interventi che compongono la misura del dissesto idrogeologico, sulla quale noi proponiamo la rimodulazione. Perché la proponiamo? La proponiamo perché all'interno di questa misura ci sono gli interventi del Piano stralcio del 2019 per 175 milioni di euro, del 2020 per 164 milioni di euro, del 2021 per 191 milioni di euro, del piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019 per 266 milioni di euro, per il piano delle aree metropolitane per 14 milioni di euro,

Ora, stiamo definanziando qualcosa in modo irresponsabile o ci stiamo ponendo il problema che questi interventi per ragioni oggettive oggi si pongono e ci pongono di fronte a un problema serio? Questi sono i progetti in essere, i progetti in essere, progetti che erano nei cassetti da molti anni e che difficilmente, per usare anche qui un eufemismo, possono superare le valutazioni previste nel PNRR sul tema della rendicontabilità, dell'ammissibilità e della capacità di spesa di questi interventi entro giugno

che qualcuno possa, tra un anno o due, venire a rimproverare noi per non essere stati capaci di spendere risorse di progetti che oggi possiamo modificare, ma che domani non possiamo in alcun modo modificare. *(Applausi)*. Questo riguarda il tema del dissesto idrogeologico,

strutture previste e delle modalità di spesa più rapide, la possibilità di valutare come parte di questi interventi possano essere finalizzati per un intervento diretto rispetto alle necessità dell'Emilia-Romagna, cosa che valuteremo nei prossimi giorni e nei prossimi mesi.

andando a leggere l'elenco di questi interventi, ci rendiamo conto delle situazioni reali e di quanto questi interventi non solo dal nostro punto di vista abbiano forse molto poco a che fare con il PNRR, ma sicuramente avranno e avrebbero una difficoltà quasi insormontabile rispetto ai temi collegati alla rendicontazione, all'ammissibilità e alla capacità di spesa, anche se in alcuni casi questi interventi - ed è il motivo per il quale noi garantiamo la copertura

Si parte da progetti di 900 o 1.200 euro per avere il 75 per cento dei progetti che sono sotto i 100.000 euro e per avere circa un miliardo di euro per investimenti e interventi sulla viabilità che, come è noto, non è ammissibile. Vogliamo porlo oggi questo tema o aspettiamo di porlo quando non sarà più possibile fare nulla? *(Applausi)*. È responsabile affrontare oggi questa questione o è irresponsabile? È corretto affrontare oggi la soluzione di questo problema e avere preventivamente un confronto con la Commissione europea che ci ci può consentire di capire se i temi dell'ammissibilità e della rendicontabilità sono compatibili con le previsioni europee o dobbiamo farlo dopo, quando non sarà più possibile trovare delle soluzioni o delle correzioni? Così possiamo fare valutazioni anche rispetto ad altri temi, come i piani urbani integrati, che sicuramente sono interventi che vanno garantiti e finanziati come tutti gli altri, perché non è in discussione in alcun modo la possibilità di finanziarli. Vogliamo dimenticare l'esperienza del Piano urbano integrato di Firenze e del Piano urbano integrato di Venezia? possiamo dimenticare che all'interno dei piani urbani integrati, dopo aver approvato un decreto interministeriale ad aprile dello scorso anno che prevedeva il finanziamento di tutti i piani urbani integrati e dopo aver previsto, nell'ambito della relazione semestrale depositata in Parlamento, con chiarezza quali sono gli aspetti collegati all'approvazione dei piani urbani integrati, la Commissione europea ha sollevato la questione di inammissibilità degli stadi che ci ha portato a trovare una soluzione con il Comune di Venezia che si è caricato sul suo bilancio la parte relativa allo stadio e un confronto complesso con il Comune di Firenze. sono due piani urbani integrati che facevano parte di questo progetto: vogliamo essere certi che nella verifica con la Commissione europea i piani urbani integrati abbiano tutti gli elementi di ammissibilità? Vogliamo essere certi che non ci troviamo di fronte a delle difficoltà di rendicontazione e, soprattutto, che i tempi collegati alla realizzazione

abbastanza delicato dal punto di vista del rischio di strumentalizzazione, perché è un tema per il quale questo Governo, a partire dal Presidente del Consiglio, ha da sempre manifestato con chiarezza e con forza assoluta attenzione e sensibilità. Mi riferisco al tema relativo all'investimento 1.2, cioè alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie. Ebbene, anche qui il nostro obiettivo è quello di salvaguardare questi interventi, interventi, che sono sempre stati finanziati con la politica di coesione e che per la prima volta vengono spostati all'interno del PNRR. Ed è opportuno ricordare anche a questo

Ad oggi, il 31 luglio 2023 (il giorno in cui ci è stato comunicato), lo stato di attuazione dei progetti vede circa il 60 per cento dei progetti non avviato. Nessuna amministrazione ha chiesto l'anticipazione, evidenziando forte criticità. Noi vogliamo

tuttavia immaginabile ignorare le considerazioni, i numeri, la situazione alla quale ho fatto riferimento adesso dal punto di vista della rappresentazione reale e oggettiva dello stato dell'arte.

sinceramente non corrispondono - mettiamola così - alla realtà dei fatti. Mi riferisco alla missione 6 salute, dove nessuno rifinanzia nulla: c'è una valutazione collegata ad un dato oggettivo

garantendo l'unitarietà della missione, non spostando risorse da questa missione, quindi aggiungendone altre sugli interventi del bilancio dello Stato relativamente all'edilizia

ai progetti di rigenerazione urbana. Anche a questo riguardo leggo tante agenzie e tante dichiarazioni. A fronte di un importo di 3,3 miliardi di euro

il termine era stato fissato al 30 luglio del 2023; su questo basta vedere i numeri e le percentuali, sulle quali io non desidero intervenire in modo dettagliato, perché non è un mio intento aprire un confronto

quindi evidentemente ci sono dei dati oggettivi sui quali è necessario intervenire oggi, perché così possiamo mettere in campo delle soluzioni. Questo vale anche per il finanziamento delle aree interne (725 milioni di euro), anticipazioni di pagamento sono solo di 18 milioni di euro. Sono le misure che noi abbiamo individuato per trovare una soluzione per questo tipo di interventi e per garantire la possibilità che essi vengano mantenuti, perché nessuno è impazzito e siamo consapevoli del fatto che gli interventi finanziati abbiano, in molti casi, costituito delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Pertanto non c'è da parte di nessuno l'idea di definanziare tali progetti e basta; c'è l'idea di comprendere quanto questi interventi non siano compatibili con le previsioni normative, di misura, di rendicontazione, di ammissibilità e di tempistica previste all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Quindi salvaguardiamo l'intervento per tempo, avviando un confronto serio con la Commissione europea ed intervenendo in un'analisi dettagliata sui tempi di attuazione. Questo è il quadro relativo alle misure di modifica che noi abbiamo individuato, cioè alle nove misure. Questo è il quadro che ci consente

spiegarne la logica e il lavoro che si sta mettendo in campo, non solamente indicare il lavoro preventivo che si è fatto con la Commissione europea sul fronte dell'ammissibilità dei progetti; penso però che sia anche l'occasione per dare alcune risposte anche rispetto a delle criticità che ho ascoltato e che non corrispondono alla verità. Innanzitutto, quando parliamo dei progetti con i principali *stakeholder* di questo Paese (ENI, Enel, Snam e Terna), parliamo di 3 miliardi complessivi all'interno del Piano e lo stiamo facendo con un obiettivo ben preciso, perché nella filosofia REPower EU ci sono tre misure di investimento e sei importanti riforme. Cito la più importante, quella del testo unico delle rinnovabili, molto atteso a livello europeo, sul quale ci stiamo

e delle imprese. In questa dimensione si apre un confronto per articolare le soluzioni e le proposte che sono state individuate, che fa parte - piaccia o meno, anche su questo sono state fatte molte polemiche - di una strategia complessiva che il Governo ha messo in campo relativamente all'obiettivo del piano Mattei, cioè di un ruolo strategico del nostro Paese e del nostro Governo all'interno del contesto del Mediterraneo, come il presidente del Consiglio Meloni Meloni ha sin dal primo momento indicato. Così come ha segnato in modo molto chiaro, nella dimensione internazionale, non solo il confronto e gli incontri che portano con sé non solamente la grande questione energetica e il riposizionamento geopolitico delle opportunità del nostro Paese nel contesto del Mediterraneo, rispetto alle opportunità infrastrutturali nel contesto europeo, ma anche una riflessione di protagonismo assoluto che ha visto la soluzione anche di altri aspetti. Cito, e non entro nel merito, l'accordo sottoscritto dal presidente del Consiglio Meloni, dalla presidente von der Leyen e dal Presidente tunisino che rappresenta

Mi sfugge la ragione per la quale dovremmo proporre la revoca dei finanziamenti per il dissesto idrogeologico o per i beni confiscati alla mafia. L'idea, abbastanza ridicola, di definirci insensibili a queste tematiche semplicemente non regge, perché è paradossale. Noi stiamo provando a trovare le soluzioni per poter utilizzare bene e al meglio le risorse previste sia all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia all'interno della dinamica degli altri programmi di intervento. Questo lo voglio sottolineare, perché è un lavoro che stiamo portando avanti soprattutto perché anche quando parliamo di politica della coesione, cioè delle risorse europee, mi piace sottolineare che l'accordo di programma quadro che ha stabilito l'assegnazione di queste risorse fu definito su valori e dati di contesto socioeconomico pre-Covid. Oggi lo stiamo adeguando, utilizzando anche un altro grande risultato che ci tengo a sottolineare, raggiunto nel Consiglio europeo di febbraio, allorquando, su proposta italiana, proprio del presidente del Consiglio Meloni, si è ottenuta la possibilità di avere flessibilità nell'utilizzo delle risorse del del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle risorse della coesione. Questo ci consente di essere competitivi con gli altri Paesi, perché modificare le regole sul regime di aiuti di Stato, così come è stato fatto, rischia di essere un favore ai Paesi che hanno una capacità fiscale propria come la Germania, e rischia di essere un elemento di totale mancanza di competitività per un Paese che non ha capacità fiscale, vista la situazione generale, come il nostro. Aver ottenuto questa flessibilità, collegandola in questo contesto, apre il fronte ad una grande opportunità, quella di poter utilizzare bene e al meglio queste risorse. Ecco l'approccio che abbiamo avuto rispetto al lavoro portato avanti in questo periodo. Lo abbiamo fatto in modo serio e responsabile. Voglio anche ribadire il livello molto intenso e positivo di collaborazione, sia a livello tecnico che istituzionale, con la Commissione europea. Le dichiarazioni di venerdì scorso, della presidente della Commissione von der Leyen, del commissario Dombrovskis e del commissario Gentiloni ne sono una autorevolissima conferma, che indica non un risultato raggiunto, ma uno *step* importante di un percorso molto lungo che con serietà e credibilità vogliamo portare avanti.

Signor Presidente, voglio cominciare proprio dal ringraziare il Ministro. un ringraziamento sincero e privo di retorica per il suo lavoro, per la chiarezza che ha portato anche oggi in quest'Aula, per la precisione che mette in ogni intervento sui progetti che riguardano il PNRR,

ha continuamente coinvolto le istituzioni parlamentari, le Commissioni del Parlamento, questa Assemblea come anche quella della Camera dei deputati. Mi lasci dire che se ci fosse stata la stessa sensibilità la stessa costanza da parte di Ministri di altri Governi, probabilmente alcuni problemi su cui abbiamo lavorato in questi mesi non ci sarebbero stati. Lo dico perché ancora oggi abbiamo ascoltato la segretaria del Partito Democratico che chiedeva, prendendo la parola alla Camera dopo il suo intervento, una maggiore partecipazione del Parlamento nelle attività che il Governo sta portando avanti e in particolare su tutto il *dossier* del PNRR. Voglio fare una brevissima cronistoria per rimettere alcuni puntini sulle come il PNRR è approdato nella sua storia in quest'Aula e in genere nelle Aule del Parlamento. Il PNRR è stato approvato il 12 gennaio 2021 in Consiglio dei ministri in quell'approvazione non c'era nessun dettaglio sulla *governance* del PNRR. Oggi sappiamo che abbiamo dovuto mettere in piedi una cabina di regia di un certo tipo; sappiamo che, chiunque chieda notizie, possiamo rispondere su chi e come governa questo *dossier*. Non c'era nulla sul cronoprogramma; oggi si chiede che cosa deve succedere e il Ministro è qui e in Commissione a rispondere. Soprattutto non c'era nulla sui progetti, nel senso che le schede dei progetti non sono mai state incardinate nella discussione parlamentare. Il PNRR è stato inviato il 25 aprile in Parlamento per essere approvato il 26 e il 27 aprile nelle due Camere: ore per leggersi 273 pagine piene di schede e di numeri; in realtà nessuno ha mai saputo quello che ha votato, perché nessuno si è mai potuto leggere quel Piano nazionale di ripresa e resilienza. anche perché il Governo del tempo era stato molto chiaro. Non c'erano modifiche da fare, era un pacchetto chiuso: prendere o lasciare. Questo a dispetto di chi oggi chiede interventi del Parlamento, trasparenza e partecipazione. Lo si vede che quello era un pacchetto chiuso, perché chi ha scritto quel PNRR forse non conosceva bene come funziona il sistema italiano e forse anche quello europeo. Prima il Ministro ha citato forse l'esempio più clamoroso, quello degli asili nido, un obiettivo importante e imponente; un obiettivo che poneva la realizzazione di 264.480 posti entro il dicembre 2025. Sapete, in una città come Roma, quanto serve per aprire un asilo nido? Cinque anni, da quando si comincia a progettarlo nella delibera comunale fino a quando si taglia il nastro. E qualcuno ha pensato, con le risorse che erano state messe a disposizione in quel caso, di poter aprire 264.480 posti entro il dicembre 2025. È dovuto intervenire il Governo, ci abbiamo messo altre 900.000 euro, abbiamo dovuto fare delle modifiche. Un altro elemento per cui chi ha scritto quel PNRR non stava su questa terra sta anche nel fatto che esisteva una tale parcellizzazione degli interventi che diventava impossibile realizzare gli obiettivi.

che ha determinato il fatto che questo Governo abbia dovuto cominciare a mettere in campo delle modifiche di quel Piano. Non è un caso, forse, che dei 55 obiettivi che dovevano essere realizzati al 31 dicembre scorso, quando questo Governo è entrato in carica, ad ottobre, ne erano stati realizzati solamente 25: gli altri 30 in due mesi li ha fatti l'attuale Governo e anche questo va raccontato e va detto. Nella famosa quarta rata - ce lo diceva poc'anzi il Ministro - abbiamo dovuto cambiare 10 dei 27

perché qui c'è in gioco l'Italia: sono soldi che ci dà l'Europa - a debito o a credito, poi, anche di questo bisognerebbe parlare - ma il ministro Fitto e tutto il Governo, insieme alle forze di maggioranza, si sono rimboccati le maniche per dire che, anche se c'è qualcosa che non va - e molto non andava, abbiamo sentito gli esempi di Firenze, di Verona e così così via - lavoriamo perché questo lavoro significa il benessere e il futuro dell'Italia. Sulle rate si è fatta tanta polemica. Nessun Paese in Europa ha chiesto le rate che abbiamo chiesto noi, a parte Spagna e Grecia. L'Italia sta facendo il suo dovere e ha fatto il suo lavoro.

Presidente della Commissione europea e così sarà anche per la quarta rata. Volevo semplicemente sottolineare questo aspetto. Ci sono tanti modi per fare opposizione: chi vi parla ha nell'opposizione la sua storia. Siamo stati opposizione per lungo tempo in questo Paese e anche in questo Parlamento. Sappiamo benissimo quali sono le regole del fare opposizione, sappiamo quali sono i criteri. Si può fare di tutto, però, quando eravamo all'opposizione, c'era un limite che non si oltrepassava mai: l'abbiamo chiamata opposizione patriottica, per cui si può fare opposizione tranne che negli interessi del Paese; quando c'è in gioco il Paese, non si fa opposizione strumentale. la quale ci possiamo confrontare e dividere su tante cose: ci confrontiamo e ci divideremo sulla riforma della giustizia; ci siamo confrontati e ci siamo divisi sul reddito di cittadinanza. Non facciamoci però la guerra sul destino dell'Italia, perché, attraverso il PNRR, passa questo, passa un futuro diverso del nostro Paese, un modo nuovo di immaginare il Paese che verrà. Puntiamo magari a migliorare ancora; puntiamo a superare gli aspetti burocratici che spesso rischiano di bloccare anche la volontà di cambiamento che poniamo in essere; dare ai Comuni, agli enti locali e ai territori gli esperti che servono per dare una mano a chi non ha la capacità di progettazione e di progettualità che il Piano richiede.

proprio sul PNRR si manifesta talvolta la diversità tra una visione conservatrice della politica e quella della sinistra. La prima è quella del piano di realtà; la seconda è quella dell'utopia.

In realtà non stiamo sognando nulla; stiamo costruendo un'Italia diversa, un'Italia che c'è, che cresce, che cambia, anche grazie a quello che sarà fatto e sarà realizzato con gli obiettivi del PNRR che il Governo raggiungerà.

buona fede o il suo impegno, ma in ragione della maggioranza che sostiene questo Governo. Come sappiamo, il PNRR è la risposta che l'Europa cerca di dare a una situazione di emergenza che si è preventivata e che collega tutto quello che sta accadendo ad una causa scatenante: una causa scatenante: le emissioni di gas serra, che contribuiscono alla creazione di tutti i problemi che stiamo vivendo, in particolare il dissesto idrogeologico.

di determinati aspetti e addirittura si chiede che la salute dei cittadini italiani venga salvaguardata dalla strumentalizzazione ideologica verso obiettivi di neutralità climatica, allora qua non ci siamo, perché, se non riconosciamo che quello che stiamo vivendo è l'effetto scatenato da una causa, cioè se non ne riconosciamo la causa, non riusciamo a pianificare e a programmare, come evidentemente bisognerebbe fare, in prevenzione anche della causa che scatena quello che accade. che ciò avvenga. Comunque, dai numeri emerge chiaro che non si sta realizzando compiutamente il PNRR. Quindi, data la considerazione che precede, mi chiedo se questo Governo non sia in grado di farlo, oppure non voglia farlo fino in fondo, perché non condivide intimamente l'obiettivo del PNRR. Peraltro, in campagna elettorale, la presidente Meloni non ha mai votato a favore; anzi, diceva che questi soldi erano sin troppi. Infatti, qua ci troviamo di fronte a un definanziamento,

la tutela e la valorizzazione del verde urbano ed extraurbano; piani urbani integrati; progetti di rigenerazione urbana. Io sono lombarda, in particolare sono di Milano e ho vissuto in diretta quello che è accaduto. Questi interventi del PNRR, su città fortemente urbanizzate come Milano, non possono aspettare anni, nel senso che quello che è accaduto, il famoso *downburst*, è stato determinato dal confliggere dell'aria fredda che proveniva dal dall'atmosfera con il suolo incandescente della città. Cosa accade nella città cementificata e asfaltata? Il calore delle altissime temperature della giornata viene assorbito dall'asfalto e ributtato fuori di notte; per assurdo, fa quasi più caldo di notte che di giorno. Quindi, se non si interviene con tempestività sui problemi delle città che questi ambiti prevedevano, non possiamo aspettare oltre il 2026. Dite che sono stati definanziati perché non si riesce ad arrivare all'obiettivo entro il 2026: accipicchia, quindi dovremo beccarci ancora più di tre anni con questo tipo di eventi.

mi chiedo dove si andranno a trovare le risorse per dare una risposta tempestiva ai problemi urgenti delle Regioni del Nord Italia. Il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico del presidente Meloni come lo finanziamo? Spero si stia pensando di spostare le risorse in base a un ordine

Quello che è importante, secondo me, è che si parli, senza peli sulla lingua, della correlazione tra i cambiamenti climatici (che finalmente questa maggioranza non può far altro che riconoscere, vista l'evidenza) e le emissioni di gas serra. e le emissioni di gas serra. Dobbiamo approfondire questo tema: magari qualcuno non ci crede, perché non è informato. Ci sono fior di scienziati che lo hanno preventivato con un certo preavviso: secondo me, è una cosa che dev'essere approfondita. Invito quindi il Governo e la maggioranza a impegnarsi seriamente a riconoscere quello che sta accadendo e a programmare e pianificare di conseguenza.

nella sua complessità e articolazione, abbia sgombrato il campo da una serie di equivoci e di titoli. Non sono qui per fare un intervento di enfasi propagandistica, a sostegno del Ministro. Tuttavia, la chiarezza con cui ha distinto i fatti da una serie di narrazioni è stata inoppugnabile. Onorevoli colleghi, potremmo anche caricare di qualche tono polemico: una delle vicende che più ha fatto discutere è stata quella delle residenze universitarie. È sembrato a un certo punto, qualche mese fa, che all'improvviso ci fosse stata una sorta di carestia edilizia nell'ambito universitario, come se, arrivato questo Governo, fossero evaporate le case degli studenti, gli studentati e tutti gli alloggi. È un problema storico del Paese, indubbiamente, di rapporto tra territorio e atenei. Dopodiché le tende, come sono spuntate, così sono scomparse. Forse adesso saranno nei *camping* estivi, giustamente, perché siamo ad agosto e anche la stagione degli esami esami conosce una sospensione. Diciamoci la verità: c'è stata una serie di proteste strumentali su questa vicenda. Non è che mi scandalizzino più di tanto, perché la dialettica politica è fatta anche di enfatizzazioni. L'alternanza democratica fa sì che i ruoli cambino nel tempo e questo è un bene, nella democrazia, però bisogna poi stare coi piedi per terra. Stiamo portando avanti un programma serio e concreto. Mi ha molto colpito, nell'intervento del ministro Fitto, ad esempio, il fatto che in materia di dissesto idrogeologico molti siano i microinterventi, addirittura sotto i 100.000 euro (ce ne sono da 1.100 euro). La documentazione e la dialettica sono quindi molto complesse nel difendere la frammentazione. È più facile difendere una grande opera pubblica, con costi magari elevati, ma comprensibili, piuttosto che una miriade di pur necessari interventi, perché vanno fatti. Pensiamo alla vicenda recente dell'Emilia-Romagna: non saranno tutti interventi giganteschi, ci saranno impianti di agricoltura da rinnovare e spese significative, ma ci saranno anche interventi di piccola portata, che sono forse quelli più difficili e complessi da gestire.

bene, anche perché, parliamoci chiaro: non voglio gettare la croce addosso ai Governi dell'epoca, i Governi Conte. Qui c'è una gara a rivendicare i meriti, ma anche noi rivendichiamo un ruolo per Forza Italia, in quella fase così difficile del Covid, quando il nostro Parlamento non aveva il voto da remoto e bisognava faticosamente riunire, anche nelle fasi più emergenziali, Commissioni e attività parlamentari, il Parlamento europeo votava da remoto

facciamo parte, che ha dato una spinta notevole alla decisione di varare il PNRR. Anzi, abbiamo rinnovato questa richiesta rispetto ad altri contesti emergenziali che si sono verificati, con i costi dell'energia e con l'aggressione all'Ucraina. Rivendichiamo quindi un percorso che oggi, in maniera analitica, il ministro Fitto ha voluto ripercorrere, con la differenza tra i fatti e le parole. Ricordo le dichiarazioni, qualche giorno fa, di alcuni esponenti dell'opposizione, quando per la terza rata sono stati erogati 18,5 miliardi di euro. La cifra differita nella quarta rata è infinitesimale rispetto ai 18,5 miliardi di euro (non ricordo se erano 500 milioni

così come sugli asili nido. Bisogna poi ascoltare e rileggere le relazioni. La discussione verteva sul fatto se la ricostruzione di edifici abbattuti e rifatti si potesse conteggiare come posti in più o in meno; in quel caso, in un'analisi molto dettagliata, immaginando la fatica di queste conversazioni in presenza, come si dice oggi,

Queste sono le discussioni e le fatiche che deve fare un Governo. Voglio quindi ringraziare l'attuale Governo e tutto il gruppo di persone che evidentemente coadiuva e supporta il ministro Fitto, che non credo possa fronteggiare tutto da con la maestria e l'esperienza che ha. È poi ovvio che tutti siamo preoccupati di tutta una serie di vicende, sui fondi di coesione o sul problema del Mezzogiorno, ad esempio. Non credo che lei, Ministro, per le sue radici, la sua esperienza e il suo ruolo

si offende, perché non competitivi rispetto alle macrocifre. Confidiamo in quello che lei ha detto per il superamento di ritardi storici; ci si lamenta, colleghi, di spese che sono state

noi teniamo al fatto che da questo dibattito emerga la concretezza dell'azione del Governo che vede lei in prima linea, ma credo che dal Presidente del Consiglio, al vice presidente del Consiglio, anche per la sua consuetudine ed esperienza europea, l'apporto sia corale.

discutendo asilo per asilo, scuola per scuola, studentato per studentato; quando torneranno dal *camping* con le tende, anche quegli studenti troveranno qualche residenza universitaria in più. Signor Presidente, ringrazio il ministro Fitto per i chiarimenti. In questi pochi minuti, vorremmo mettere ordine su tre principi che immagino ci debbano trovare tutti d'accordo e su un esempio che, analogamente, immagino ci debba trovare d'accordo. Il primo principio che la Lega da sempre ha posto con chiarezza è, che essendo la stragrande maggioranza di queste risorse a debito, quando fai un debito, devi evitare che quello che realizzi renda meno del costo degli interessi, altrimenti ci perdi, tutti i progetti devono andare in buca, altrimenti perdi le risorse. Questo è un principio cardine, che è stato finalmente accolto e ne siamo particolarmente contenti.

In buona sostanza, leggono i titoli dei giornali. Su questo tema fondamentale per la credibilità del sistema Paese abbiamo per mesi avuto titoli allarmistici che hanno minato la credibilità dall'interno del sistema Paese, che è l'esatto opposto di fare squadra. terza considerazione riguarda uno dei pilastri del PNRR, che è quello del cambiamento climatico e dell'ambiente. è ovvio che l'effetto delle emissioni sul cambiamento climatico, ma delle emissioni generali, non si ferma alle frontiere, questo mi sembra pacifico e dovrebbe trovarci tutti d'accordo. L'obiettivo, quindi, dev'essere la loro riduzione a livello globale.

Il Canada vale più o meno lo stesso in termini di PIL e fa emissioni per il 2,3 per cento. È evidente, quindi, che conviene portare la produzione laddove si fa produzione con meno emissioni, se vogliamo ridurre le emissioni a livello globale.

del PIL. Per forza: buona parte dell'energia è prodotta con il carbone, quindi è ovvio che, se vogliamo ridurre le emissioni a livello globale, dobbiamo riportare più produzioni possibili in Italia, dove la produzione è fatta con *standard* di emissioni migliori a livello mondiale. *(Applausi)*. Questo è un principio che dovrebbe trovarci tutti d'accordo, lasciamo perdere la politica. Se aumentiamo dello 0,3 per cento le emissioni in Italia, a parte che facciamo più PIL, riduciamo le emissioni a livello globale, perché riusciamo a produrre nel modo migliore possibile. faccio un esempio che va in questa direzione. Nel PNRR, giustamente, si riporta l'attenzione sulla produzione di biometano, cosa sacrosanta, perché tutto il biometano che riusciamo a produrre sostituisce il metano da fonti fossili.

(FORSU), la frazione umida dei rifiuti: 35.000 tonnellate l'anno di frazione umida dei rifiuti sono una materia prima che ci sarà in eterno e quindi è quanto di meglio si può fare per l'ambiente.

produce 4 milioni di metri cubi di metano l'anno, che sostituisce il metano fossile. Si tratta di un progetto che quindi teoricamente è esattamente in linea con l'indicazione del PNRR e del pilastro dell'Unione europea della cosiddetta economia circolare. Ci sono voluti dieci anni e tanta fatica, ma adesso da questo impianto pilota se ne faranno tanti in Italia e non solo, anche in Europa e nel resto del mondo. Ebbene, chi ha contrastato per dieci anni questo impianto? PD e 5 Stelle. Questo per dire che qui dovremmo iniziare a ragionare nell'interesse del Paese e dell'ambiente, lasciando perdere le ideologie. La Lega, poi, l'ha sempre detto: per noi ambiente e tutela ambientale non solo possono, ma devono convivere.

e ringrazio anche il Ministro per averci detto come si governa. In quest'Aula, se escludiamo Fratelli d'Italia, tutte le altre forze politiche hanno votato il PNRR nella scorsa legislatura, ma adesso scopriamo che ci sono gravi problemi anche di ammissibilità e che in qualche misura è stato approvato velocemente in Italia, ma a quanto pare anche dalla Commissione europea. Scherzi a parte, c'è un tema di cui quest'Assemblea

patriottismo italiano ed europeo, perché l'Italia è stata la prima delle Nazioni europee ad essere colpita dal Covid. Adesso lo lo abbiamo dimenticato e sul Covid facciamo le inchieste mirate, ma c'è stato un momento in cui in questo Paese c'era la solidarietà, c'erano le ragazze che giocavano a tennis sui terrazzi, le serenate sui balconi,

aggiustamenti che sono rimodulazioni, ma sostanzialmente all'interno della stessa missione e che non cambiano né gli obiettivi né i tempi; aggiustamenti che modificano alcuni tempi, ma che lasciano intatte le misure; proposte di rimodifica del Piano, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento che accompagna il PNRR europeo.

particolarissimo in cui facciamo partire questo capitolo di REPowerEU rifinanziandolo, anche aggiungendo fondi che derivano da altri interventi che cancelliamo, sui quali però diciamo che ci possono essere altri fondi comunitari. È quindi innanzitutto sul piano metodologico che noi contestiamo questo documento. Contestiamo anche il ritardo di REPowerEU, misura che si è conclusa alla fine dell'anno precedente in quest'Aula, quando abbiamo parlato del decreto-legge Quando abbiamo parlato della legge di bilancio e delle misure sulla domanda di energia, ci siamo chiesti più volte perché non attivavamo misure su REPowerEU in quella sede, liberando risorse per per altri usi, ad esempio per la sanità, per i costi che riguardavano l'inclusione sociale. In quel caso, non c'è stata risposta, ma oggi scopriamo che c'è la proposta di alcune misure che finanziano la domanda proprio nel capitolo REPowerEU. questo caso, il tema che si pone politicamente è perché è stata fatta questa commistione di situazioni così diverse e perché non c'è stata la possibilità di portare

diverse obiezioni. La prima l'ho già esplicitata: l'articolo 21, cioè quello che - lo ricordo - impone determinate condizioni per chiedere la modifica del Piano, totale o parziale, presuppone che si passi prima in Parlamento. Ora, nella parte introduttiva di questo ultimo *report* ho letto che ci sono state tantissime interlocuzioni con la Commissione.

non capiamo se l'avvio dell'articolo 21 sia stato posposto formalmente, ma c'è già stato sostanzialmente. Lei qui ci dice una cosa corretta, cioè che dev'essere avverso al rischio, per cui se ci sono dei problemi, non vuole trovarli

di una squadra che, per paura di non riuscire a portare a casa il risultato, a metà campionato si ritira, perché dice di avere troppa paura che alla fine gli diano la colpa del risultato. Nella metodologia, abbiamo trovato alcune frasi interessanti come questa, che leggo: criticità connesse all'attuazione di specifiche progettualità che potrebbero avere maggiore respiro gestionale, se incluse in programmazioni che garantiscono cronoprogrammi differenti oltre il 2026. Per queste criticità, di cui ha fatto alcuni esempi, siamo davvero convinti che non ci fossero altre soluzioni? Quando facciamo un'analisi di impatto, la facciamo anche sul famoso controfattuale. Siamo sicuri che non ci fossero altre soluzioni? Queste criticità ce le ha in qualche modo comunicate la Commissione europea o sono un'iniziativa

però voi - lei e Fratelli d'Italia - rappresentate le uniche forze politiche che non hanno mai votato a favore di questo Piano, neanche in Europa, e che in campagna elettorale, prima di entrare nel dettaglio, hanno detto che l'avrebbero modificato. Quindi noi non sappiamo se ci sono sono fatti che hanno bisogno di interventi o degli interventi che in qualche modo inventano dei fatti. *(Applausi)*. Alla fine, la misura che che ci ha lasciato più perplessi riguarda questo taglio di circa 16 miliardi. Dico perplessi per diverse ragioni: intanto, per la natura degli interventi e poi perché all'inizio, a pagina 15 del *report* (nella prima versione), si citano le raccomandazioni della Commissione europea. Ebbene, si dice che la questione del dissesto idrogeologico è una delle prime sulle quali l'Italia deve intervenire. Guarda caso però è quella sulla quale stiamo tagliando. Noi su questo ovviamente siamo contrari, ma non solo noi, come su tutta la parte che riguarda i Comuni e tutta la parte che riguarda la digitalizzazione e alcune forme di rimodulazione. Ricordiamoci che questo Piano contiene anche riforme di misure che servono a migliorare

allora realizziamo parte dei progetti con altri fondi europei e d'altra parte sappiamo dalla storia che questi fondi europei non li sappiamo spendere tutti, quindi abbiamo delle risorse. Ma se non le sappiamo spendere,

Il piano Mattei per l'Africa è qualcosa che spesso sentiamo evocare in quest'Aula, ma sinceramente non ho mai letto una riga su questo. avevamo e abbiamo il piano Mattei per l'Italia: si chiama PNRR *(Applausi)* ed è quello che può cambiare il nostro destino. C'è una responsabilità del Governo e del Parlamento e ci auguriamo che lei possa accogliere

va al ministro Fitto anche per il suo continuo confronto sulla sfida del PNRR, che sta portando avanti con il Parlamento, sia nelle Commissioni sia nelle Aule. Il Ministro è stato molto chiaro ed abbiamo sempre compreso quello che ha detto quando è venuto in Commissione e in Aula. È stato detto È stato detto tante volte, ma evidentemente ancora non è molto chiaro per alcuni: oggi il Ministro è in Parlamento per discutere le proposte di modifica complessive al Piano, qualcosa che i Governi precedenti, nonostante le sollecitazioni di Fratelli d'Italia, non hanno fatto. Se questo fosse accaduto prima, si sarebbe evitato qualsiasi problema, anche solo ipotetico. Inoltre, da quando è stata approvato il PNRR, circa tre anni fa, sono mutate radicalmente alcune situazioni oggettive oggettive di contesto: la guerra, la crisi energetica e l'aumento del costo delle materie prime. I mutamenti del contesto di riferimento e le criticità emerse nella fase di attuazione del Piano hanno reso indispensabile effettuare una ricognizione puntuale dei progetti inclusi nel Piano stesso, al fine di individuare le modifiche e le integrazioni necessarie per conseguire i traguardi e gli obiettivi previsti fino al 30 giugno 2026. Ecco perché oggi siamo qui a discutere delle modifiche al PNRR che il Ministro ci ha illustrato, insieme all'attestazione dell'avvenuto conseguimento della terza rata, che farà entrare 18,5 miliardi nelle casse dello Stato e con la possibilità di ottenere entro la fine dell'anno i 16,5 miliardi della quarta rata. Si tratta di un risultato importante, che conferma le risorse che ci erano state assegnate. In buona sostanza, la terza rata, anziché di 19, sarà di 18,5 miliardi, ma i 500 milioni mancanti non sono persi, come qualcuno vuole far credere, ma sono trasferiti come *target* nella quarta rata, che da 16 passa a 16,5 miliardi, lasciando inalterato il totale dei 35 miliardi per il 2023. È tardi? È presto? Si poteva fare prima? Non so dirlo, ma l'importante è che l'obiettivo sia stato raggiunto senza perdere i fondi. Dobbiamo anche evidenziare il rapporto proficuo con la Commissione europea, che non ha mancato di apprezzare le riforme di ampio respiro che stiamo implementando: la riforma della giustizia, che il Senato esaminerà nelle prossime settimane; quella del fisco, che affronteremo nell'Aula del Senato nelle prossime ore; la riforma della pubblica amministrazione; la riforma collegata all'istituzione di una zona economica speciale nel Mezzogiorno, una ZES unica, che permetterà investimenti agevolati con benefici fiscali e agevolazioni per le nuove imprese e per quelle già esistenti. Abbiamo quindi un giudizio largamente positivo da parte delle istituzioni europee e di questo dobbiamo essere lieti, perché l'Italia sta finalmente crescendo e acquistando un ruolo autorevole in Europa e nel mondo. La revisione del Piano è stata uno dei principali impegni che il presidente Meloni e il Governo hanno assunto ad inizio legislatura. In tale contesto, il Governo, per i progetti che non consentono la conferma del finanziamento a valere sul Piano, ha già deciso di attivare le misure necessarie per riprogrammare le risorse a favore di interventi coerenti e realizzabili nei tempi previsti. È assicurato quindi il completo finanziamento degli interventi stralciati dal PNRR. Nel complesso, le amministrazioni hanno presentato 140 proposte di modifica e di riforma. Delle riforme abbiamo già parlato. Possono essere distinte in tre categorie: vi sono quelle di natura formale; la seconda tipologia riguarda la riprogrammazione di alcune misure, come ad esempio gli interventi concernenti l'Alta velocità; l'ultima categoria riguarda invece le misure che si propone di definanziare con il PNRR e di salvaguardare attraverso la copertura con altri fondi di finanziamento, come il Piano nazionale complementare al PNRR e i fondi delle politiche di coesione (nuove misure per un ammontare di 15,9 miliardi di euro). Il Governo perciò ha proposto di definanziare alcuni investimenti del PNRR e di spostare tali risorse sul REPower EU, quindi da un punto di vista contabile il saldo è neutrale. Come detto, quindi, non c'è alcun taglio dei progetti previsti dal PNRR, ma è semplicemente una riorganizzazione volta a consentire il rispetto degli impegni presi. Nei giorni scorsi le opposizioni hanno cavalcato la polemica, diffondendo notizie non complete e artefatte circa la rimodulazione del Piano che intaccava i progetti riguardanti i beni confiscati alla mafia e le risorse di alcuni progetti per i Comuni. Le preoccupazioni relative alle misure dei beni confiscati alle mafie e alle misure che interessano specifici Comuni, che nella proposta del Governo si propone di spostare su altri fondi di finanziamento,

ipocritamente, caro Ministro, che ci sono alcuni punti che meritano di essere attentamente valutati prima di essere definitivamente eliminati. Mi riferisco alle tante misure che riguardano i Comuni, in particolare alle opere di piccola e media portata, di cui alla legge di bilancio del 2020. Per tali interventi bisogna valutare con attenzione, per esempio, se vi è qualche problema con la registrazione sulla piattaforma ReGiS di progetti già avviati dagli enti locali. È una questione che va approfondita. Ma il punto che mi preme sottolineare è che le risorse destinate ai Comuni, che vengono definanziate dal PNRR, devono essere assolutamente recuperate e sono sicuro che sarà così. Si è parlato di utilizzare il fondo per lo sviluppo e la coesione, che ha una proiezione temporale più estesa, o i fondi strutturali europei, anch'essi non ricadenti nel termine del 2026. Come tutti sanno, il nostro Governo sta lavorando per un utilizzo flessibile dei fondi strutturali europei, secondo il principio della flessibilità tra i fondi introdotto nel Consiglio europeo del febbraio 2023 su iniziativa dell'Italia e del presidente Meloni. Si continua ad attaccare il ministro Fitto, che sta facendo un lavoro encomiabile insieme a tutto il Governo. *(Applausi)*. Noi siamo stati sempre chiari: il PNRR andava attualizzato e modificato alla luce delle mutate esigenze. Nella scorsa legislatura, non a caso, eravamo gli unici all'opposizione e gli unici a dire queste cose, ma nessuno ci ascoltava, nonostante la nostra opposizione responsabile. Alla fine ci sedemmo dalla parte del torto, perché gli altri posti erano tutti occupati *(Applausi)*, aspettando che il tempo - come sta facendo - chiarisse le cose e ci desse ragione. il Piano prevede però anche il rafforzamento dei finanziamenti per gli esili nido, il REPowerEU, i fondi per la ricostruzione in Emilia-Romagna e per il finanziamento, per esempio, dei contratti di filiera in agricoltura. Per me ci sono temi che trascendono i colori politici: l'interesse nazionale e il benessere dei cittadini dovrebbero sempre prevalere sulle faziosità di parte. I fondi europei rappresentano non un'occasione per questo o quel Governo, ma un'opportunità storica per rilanciare il futuro della nostra Nazione, anche se il dibattito di questi mesi e degli ultimi giorni racconta altro. Purtroppo l'opposizione italiana, con l'atteggiamento ostativo e strumentale, sembra preferire attaccare il Governo piuttosto che volere il bene della Nazione: sarebbe felice di vedere l'Italia fallire solo per dare un briciolo di sostanza alle sue esterne critiche strumentali. Contrariamente però alla loro narrazione catastrofica, però, il presidente Meloni e il ministro Fitto stanno portando avanti con serietà e autorevolezza la questione del PNRR in Europa. La speranza La speranza delle opposizioni - e concludo, signor Presidente - di ottenere ragione attraverso il disastro dimostra la mancanza di fiducia nelle proprie capacità politiche. Non è con la speranza del fallimento che si costruisce un futuro migliore, ma con un'opposizione costruttiva orientata al bene comune. Il Governo ha rassicurato gli italiani che nessun ritardo e nessun fondo saranno perduti. Per fortuna gli italiani hanno scelto di dotarsi di un Governo serio che ha fatto ora una proposta realistica, ben più realizzabile di quell'accozzaglia di utopie messe insieme dai precedessori. Abbiamo avuto il coraggio di fare un bagno di realismo, che la Commissione europea ha apprezzato. Con questa operazione possiamo dire basta con i disfattismi interni che hanno solo carattere ideologico. La sinistra La sinistra vuole creare la società dell'ansia permanente, con un racconto che non lascia speranze per il futuro e prefigura catastrofi improbabili. Il Governo ha fatto la cosa più semplice e intelligente: spostare i progetti realizzabili entro il 2026 su altre fonti di finanziamento. tramite lei, Presidente, ai nostri dirimpettai, vorrei dire: state sereni, perché questo è un Governo che opererà sempre con la sapienza del cuore e il sentimento della ragione, perché è certo di stare dalla parte giusta, dalla parte degli italiani, guardando avanti l'orizzonte chiaro, verso un futuro prospero e florido. Grazie presidente Meloni, grazie ministro Fitto, la nostra disponibilità a lavorare con il solito massimo impegno nelle prossime settimane. Grazie a tutti e avanti così, tutti insieme, per il bene del nostro amato Paese. Signor Presidente, ringrazio il Ministro per il suo intervento e i suoi chiarimenti. Io faccio fatica ad accettare la narrazione per cui la mia parte politica sarebbe disfattista. Io ho sempre dichiarato, a nome mio e del mio Gruppo, la totale disponibilità a collaborare con il Governo e con la maggioranza per sfruttare al meglio i fondi del PNRR. Quindi, mi perdoni chi mi ha preceduto, ma non sono d'accordo con quello che è stato detto. Lei, Ministro, tra le altre cose, ha detto che va rispettata la data del 2026, anche per evitare che qualcuno possa poi rimproverare voi dell'attuale Governo se non ci si dovesse riuscire. Vorrei dire che l'autocelebrazione e il rimprovero di chi governava prima è caratteristica della vostra compagine di Governo. Dalla mia parte politica si governa, ci si rimbocca le maniche e non ci si lamenta di chi ha governato prima. Le ricordo che lei fa parte del Governo della Repubblica (articolo 92 della Costituzione). L'articolo 114 della Costituzione, inoltre, dice che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. 5 della Costituzione afferma che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali e attua, nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo. Questo vuol dire che è compito del Governo far funzionare al meglio la macchina Paese, il sistema Paese, curando che tutti gli enti territoriali che costituiscono la Repubblica siano in grado di perseguire al meglio l'interesse pubblico, ciascuno al suo livello. Invece, la revisione del PNRR che lei, Ministro, propone a quest'Assemblea va esattamente nella direzione opposta: si tolgono risorse, peraltro già accertate e in parte già impegnate, ai Comuni, soprattutto ai piccoli enti, e le si sposta nello Stato centrale. Se queste risorse - come lei dice - vengono date comunque prelevandole altrove,

che ha accentrato nei piani alti del Governo centrale la gestione del Piano, togliendo poteri e funzioni agli enti locali. Il secondo è la revisione del Piano che toglie ai territori 16 miliardi di euro per portarli in capo alla macchina centrale. Come viene fatto uno scippo vero e proprio agli enti territoriali dei fondi di sviluppo e coesione, perché, se con i fondi di sviluppo e coesione si deve pagare quello che si sarebbe pagato coi fondi del PNRR, vengono meno i fondi di sviluppo e coesione per i Comuni. si hanno il mancato rispetto del dettame costituzionale, non soltanto il danno agli enti locali e alla popolazione dei territori interessati, ma anche e soprattutto la perenne tendenza della destra ad accentrare il potere degli organi di governo dello Stato, perché per voi è il potere che conta, non l'interesse dei cittadini. Il suo è il Governo Penelope: di giorno tesse la tela dell'autonomia differenziata, di notte la disfa per dimostrare un volto ben diverso, quello di un centralismo senza precedenti, che rischia fortemente di ridurre l'impatto e la portata del PNRR.

Come ci insegnano anni di studi e convegni sulla sussidiarietà, nessuno meglio degli enti locali può sviluppare politiche che portano diretto beneficio alla vita dei cittadini. i benefici riguardavano tra l'altro un tema non da poco: la messa in sicurezza dei territori, la lotta al dissesto idrogeologico, la riqualificazione delle periferie, il contrasto al degrado e alle disuguaglianze sociali e territoriali. ministro Fitto, ancora una volta il Parlamento viene messo davanti al fatto compiuto, mentre molti amministratori locali, anche della sua parte politica, denunciano e contestano quanto sta accadendo e i danni che procurerà ai loro cittadini. Non so quale di questi due aspetti sia il più grave. Ma quello che è certo è che ancora una volta colpite le fasce più deboli e lo fate con una politica centralista che, in particolare per noi del Gruppo Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase,

la narrazione per cui da una parte c'è chi fa il tifo per l'Italia e dall'altra parte ci sono i gufatori che sperano che l'Italia vada in crisi è francamente una rappresentazione alquanto infantile. Due dei tre partiti dell'attuale Governo hanno scritto insieme all'attuale opposizione il PNRR, l'hanno presentato e votato. Quindi, continuare a dire che c'è una parte che spera che questo Piano fallisca è veramente stucchevole *(Applausi)*. E lo è non solo perché noi l'abbiamo portato a casa, ma perché - come mi era capitato di dirle in un precedente intervento il PNRR non appartiene a questo Governo, è stato scritto in una fase Conte, portato a casa da Draghi, adesso voi dovreste realizzarlo e gli effetti li vedranno anche i Governi futuri. Era un piano che si chiama Piano di ripresa e resilienza, perché dopo la pandemia, che è stata particolarmente cruenta nel nostro Paese, non soltanto per le vittime, ma perché non avevamo le infrastrutture adatte per superare una tale tragedia, doveva essere il momento della ripresa economica e e soprattutto la possibilità, per i nostri giovani, di vedere nell'Italia il Paese del futuro. Per questo non la bevo la storia che i 16 miliardi di euro non sono propriamente un taglio. In realtà abbiamo tolto i 16 miliardi di euro dal PNRR, ma c'è una corresponsabilità, una con-solidarietà di altri fondi europei. I 16 miliardi di euro del PNRR non tornano e non torneranno più *(Applausi)*. Saranno altri fondi, ma quelli non ci saranno più. Purtroppo, tra le voci mancanti - ahimè - c'è quella del dissesto idrogeologico, per cui è inutile poi fare, quando succede un'alluvione, un'informativa urgente sul fatto che bisogna intervenire, quando non si interviene. Perché fra cinque anni non avremo le opere messe a terra? Avete cambiato la *governance* nel tragitto. Noi vi dicemmo di fare attenzione, perché cambiare la *governance* una volta iniziata l'esecuzione del PNRR poteva ritardare i piani. Avete assunto giustamente la responsabilità di farlo - oneri e onori di chi governa - ma oggi non ci potete dire che, a causa del cambiamento, tra cinque anni non avremo i progetti messi a terra *(Applausi)*. Anche perché - lo dico per l'ultima volta - non è che, quando diciamo di portare a casa l'unità di missione, lo facciamo perché siamo particolarmente innamorati di quel Governo. Lo diciamo perché anche i fondi regionali prima di quell'unità di missione, non riuscivano a essere messi a terra, proprio per la complessità del nostro Paese. E l'unità di missione nacque perché tutte le istituzioni collaboravano e i tempi si riducevano. Ecco perché continuiamo a insistere. Ecco perché ci sembra assurdo che tutto questo sia stato tradotto in un ordine del giorno che fa fatica a vedere la luce.

che era una delle locomotive italiane nella produzione di PIL. Per questo abbiamo chiesto se eravate sicuri di non poter mettere altre risorse per far ripartire immediatamente quella Regione e se eravate proprio sicuri di aver fatto tutto per poterla far rinascere. Oggi

un Testo unico sulle rinnovabili che siamo pronti a discutere con l'Unione europea. Ma lei ha visto il Piano relativo alle aree idonee per la creazione delle risorse e delle energie alternative?

aver visto un po' di provvedimenti, non soltanto di sua responsabilità, ma anche dei Ministeri che gravitano in questo Governo,

derubrichiamo completamente dalla nostra e dalla vostra attività di Governo, a venir meno non sarà soltanto la ripresa e la resilienza, ma il resto delle rate del PNRR. Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, le comunicazioni del ministro Fitto confermavano purtroppo l'atteggiamento e l'azione supponente da parte dell'Esecutivo che sul Piano di ripresa e resilienza sta - ahinoi - dimostrando quanto Giorgia Meloni e i suoi sodali fossero ben lontani dall'essere pronti dall'affrontare con responsabilità e cognizione di causa la grande opportunità per l'Italia di portare a terra i 209 miliardi del Piano. Voglio ricordare, a scanso di equivoci, che il Paese intero si sta giocando l'occasione irripetibile di recuperare e colmare le distanze con investimenti in infrastrutture come asili, alloggi per studenti universitari, investimenti per telemedicina e medicina di prossimità, interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico. Per questo, responsabilmente, fin dall'inizio, come MoVimento 5 Stelle ci siamo messi a disposizione per far sì che l'Italia non perdesse neanche un centesimo di risorse assolutamente necessarie per tutto il Paese e addirittura vitali per le Regioni del Sud. del Sud. Oggi ci ritroviamo invece a constatare dei fatti che non sono relegabili - cito testualmente - a polemiche che rischiano di portarci fuori strada, come ha provato a sostenere il ministro Fitto. No: sono fatti che il Governo deve riconoscere in tutta la loro gravità, come la rimodulazione del PNRR, con cui avete escluso progetti per 16 miliardi di euro per gli interventi sul dissesto idrogeologico e contro il rischio di alluvioni dimostrando ancora una volta quanto siete totalmente distaccati dalla realtà e dalle concrete e drammatiche esigenze delle persone. Non potete rispondere a chi ve lo fa notare dicendo semplicemente che è falso. - mi perdoni Ministro, per suo tramite, Presidente - agli italiani la parola di chi dice che questi progetti saranno spostati e finanziati con i fondi di sviluppo e coesione non può bastare. E non può bastare perché il Servizio studi del Parlamento, in una dettagliata relazione sul monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rileva che non ci sono coperture alternative per i 16 miliardi definanziati. Abbiamo infatti solo un generico rinvio ad altri fondi e non una puntuale destinazione di queste risorse alternative. Facciamolo capire ai cittadini che ci stanno seguendo. È una promessa tipo ci vediamo a babbo morto? *(Applausi)*. Non può bastare soprattutto perché quello che il ministro Fitto vorrebbe far passare per un semplice spostamento è un definanziamento a tutti gli effetti e ne spiego le ragioni. Faccio un esempio pratico, perché naturalmente non posso citare la mia Sicilia o la mia Palermo, per la quale mi sono interessata in prima persona. prima persona. Ci sono dei fondi che erano destinati a Palermo e che sono stati stralciati. Si trattava di fondi che riguardavano l'intera rigenerazione urbana della costa Sud, dalla foce del fiume Oreto alla Bandita, del recupero dell'approdo della borgata di Vergine Maria e il primo lotto del Parco Villa Turrisi. E mi dica, signor Ministro, cosa succede se spostiamo l'oltre miliardo e mezzo sui fondi di sviluppo e coesione, destinando delle risorse che vengono necessariamente sottratte ad altre opere strategiche che si potrebbero realizzare con quei fondi? *(Applausi)*. Quei fondi spariscono. Anche Anche un bambino si accorgerebbe che il Governo sta facendo il gioco delle tre carte e probabilmente siamo nella stagione del mojito*.* Non mi viene in mente altro per trovare una spiegazione alle parole dell'esponente della maggioranza in quota Lega che oggi ha pensato di dare il suo contributo costruttivo al dibattito sullo stato del Piano nazionale di ripresa e resilienza cercando di giustificare i ritardi clamorosi del Governo dei pronti ricordiamolo - parlando testualmente di «pozzi avvelenati dal Governo uscente che ha volutamente creato una burocrazia parallela per mettere in difficoltà il Governo successivo». Ma volete prendere atto una volta per tutte che il Piano nazionale di ripresa e resilienza è patrimonio dell'intera Italia e non un vostro *slogan* da campagna elettorale? *(Applausi)*. La narrativa inaccettabile è quella che state facendo voi. In un altro passaggio delle comunicazioni del ministro Fitto si evidenzia tutta la supponenza con cui il Governo sta affrontando la messa a terra del Piano nazionale di ripresa e resilienza e mi riferisco a quando il Ministro dice testualmente che «il lavoro sulla terza rata ci insegna che bisogna costruire soluzioni prima che si arrivi al problema». Ministro, sempre per il tramite del Presidente, allora, perché a proposito dell'esempio dei fondi definanziati a Palermo che ho citato prima non ha ritenuto di dover tener conto delle interrogazioni parlamentari e degli emendamenti con cui più volte abbiamo sollecitato il Governo e la maggioranza sul rischio di perdere questi fondi che puntualmente sono stati persi. Perché ci avete ignorati quando abbiamo chiesto che si garantissero gli interventi strategici per la città di Palermo e si intervenisse sulle scadenze di aggiudicazioni dei lavori che di fatto erano facilmente rimodulabili, perché erano delle scadenze imposte internamente dall'Italia? E invece no: non erano delle scadenze dell'Europa, ma il Governo è rimasto sordo; quindi si è arrivati al problema senza ascoltare le soluzioni proposte. L'immobilismo del centrodestra e la noncuranza rispetto ai nostri avvertimenti istituzionali hanno causato oggi la perdita di quelle risorse e lo stralcio di questi interventi fondamentali: è questa l'idea che avete di soluzione prima che si arrivi al problema? Complimenti! Veramente non c'è che dire: efficace come sempre. Insomma, veramente pensate che queste modifiche siano utili alla soluzione dei problemi? Quello che abbiamo sentito oggi in Aula dimostra tutto il contrario. mi sembra ormai evidente che la frittata fatta di cui ha parlato tempo fa il senatore Borghi è quella che voi state servendo all'Italia, continuando a trattare il PNRR in modo totalmente inadeguato. *(Applausi)*.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatrici e senatori, ringrazio il ministro Fitto che ha documentato in modo esauriente la sua azione e quella del Governo nella trattativa con l'Europa per i tempi e la realizzazione dei progetti del PNRR. Ha presentato un'analisi dettagliata misura per misura e ha dato quella definizione che è mancata nella fase iniziale. Abbiamo letto sui giornali che il Governo definanzia. No, assolutamente il Governo non definanzia: il Governo è stato bravo a ritrattare, a fare modifiche a fronte di un aumento del costo delle materie prime, ad esempio, e anche a fronte di una reale incapacità di alcuni progetti di essere effettivamente realizzati. Come ha ricordato lei, ministro Fitto, per l'ennesima volta, il Governo è riuscito a portare a casa tanti soldi, soldi, perché l'Italia era un Paese messo peggio in Europa grazie a chi l'aveva amministrato in precedenza e che aveva sempre detto no, senza una visione di lungo termine, senza fare investimenti in infrastrutture stradali e ferroviarie; per non parlare della manutenzione - e si è visto che cosa è successo - in edilizia scolastica, in edilizia universitaria - e abbiamo visto le proteste degli studenti universitari - oppure in altri settori. La ringrazio, signor Ministro, per il continuo confronto col Parlamento che sta portando avanti sia nelle Commissioni, specialmente nella Commissione politiche dell'Unione europea - a detta di qualcuno lavora poco, ma è al quarto posto per numero di sedute - sia nelle Aule parlamentari stesse, sia alla Camera che al Senato. È una disponibilità importante, perché ci permette di avere interlocuzioni costanti e aggiornamenti sullo stato del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Da quando il Piano è stato approvato sono avvenuti fatti importanti che hanno determinato la necessità di una sua rinegoziazione (la guerra, la crisi energetica, l'aumento del costo delle materie prime, per non parlare della siccità) e che incidono non poco su un programma che complessivamente arriva a 110 miliardi di euro, in riferimento al numero delle opere pubbliche programmate. Nella relazione di bilancio dell'8 febbraio 2021 si leggeva che, nel Piano trasmesso al Parlamento, non erano indicate le informazioni di dettaglio dei singoli investimenti; in particolare non c'erano un cronoprogramma, l'indicatore sullo stato di avanzamento, nonché gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si volevano raggiungere attraverso tali interventi. Questa è la perfezione che oggi viene chiesta direttamente dall'opposizione, secondo cui tutto era perfetto e invece noi lo stiamo rovinando. Ebbene, quello che fu fatto allora avvenne in un momento di emergenza, con un'approssimazione oggettiva che, con l'avanzare del tempo, ha dimostrato tutte le sue criticità e le necessità di revisione, come il Governo ha fatto e sta facendo. quindi una ricognizione seria e capire se gli indirizzi dati erano veramente coerenti e adatti al nostro Paese non è nient'altro che guardare in faccia alla realtà, dialogare con il territorio e rendersi conto delle effettive necessità.

Questa è la risposta del Governo che denota anche la sua attenzione per risolvere i problemi della natalità in Italia. Il Ministro nel suo intervento ha fatto riferimento anche alla necessità di utilizzare altri fondi complementari al PNRR che possono e devono essere rivisti, ma anche gli altri fondi europei. Questa è una importante occasione di grande serietà proprio per utilizzare questi fondi in modo coerente, come in questi anni non era mai stato fatto. Quando si contrae un debito si deve essere consapevoli e responsabili rispetto alla capacità di restituirlo successivamente. Noi abbiamo contratto un debito e ci siamo vincolati a delle riforme e a delle modifiche strutturali nel nostro Paese. Ci siamo vincolati a seguire un piano molto severo di riforme, cui dobbiamo essere responsabili. Tuttavia, signor Ministro, questa responsabilità si deve trasferire a 360 gradi a tutti i livelli del Paese. Non mi riferisco solo direttamente al Governo e a noi parlamentari, ma anche e soprattutto ai funzionari stessi che scrivono i bandi a livello ministeriale e a livello regionale, che inseriscono criteri molto spesso assurdi. Potrei farne un elenco infinito: l'ultimo,

La Lega voterà a favore della proposta di risoluzione di maggioranza, perché rispecchia quella fatta nel 2021: prendiamo gli stessi impegni e ci impegniamo nello stesso modo per arrivare a un *target* e a una leale collaborazione tra le istituzioni, i Comuni, le Regioni e lo Stato, per arrivare direttamente al risultato di utilizzare i fondi europei per ritrasformare il nostro Paese in modo efficiente ed efficace.

facendo delle domande al ministro Fitto e sono sicura che troverà il modo di rispondermi, essendo stato presente nel dibattito parlamentare qui in Senato con una certa assiduità.

comprendere alcune cose. Innanzitutto, e lo dico da persona del Sud, quale mi ritengo, verranno rispettate le soglie degli investimenti al Sud. E lo dico visto che il PNRR era innanzitutto un grande Piano di rilancio dell'Italia, di trasformazione; un Piano di investimenti - ricordiamocelo non sulla spesa corrente, ma per la trasformazione verso la modernità e di superamento della crisi del nostro Paese. L'altro tema riguarda la parità di genere nel mondo lavorativo: noi ci eravamo molto battuti perché venisse rispettata la parità del lavoro di uomini e donne con una di uomini e donne con una mole di interventi che vale più di 200 miliardi e che significava rilancio non solo dell'occupazione femminile, ma anche del PIL e della realtà produttiva del nostro Paese.

del finanziamento previsto va bene e, quindi, è l'ultima volta che veniamo qua con un articolo 21? Queste sono piccole domande che però richiederebbero una risposta precisa, e non articolata in mezz'ora di intervento, ma precisa. Vogliamo solo sapere sì o no. Sempre oggi, perché i dubbi all'opposizione vengono e lo dico al senatore Scurria cui mi lega grande simpatia personale,

È non solo un mio diritto, ma è anche un dovere che ho come Parlamentare, che abbiamo in questo Parlamento, nel rispetto delle nostre prerogative, che troppo spesso ci sono state tolte o da cui siamo stati spogliati anche a causa degli eventi succedutisi in decenni difficili, ma di

che trasformano i processi, non basta. Le risorse servono, senza si fa poco; ma, senza riforme, non servono. Si buttano. Quindi, io sono molto preoccupata quando in Parlamento non soltanto si tolgono le risorse, ma non ci sono neanche le riforme. Non è proprio un buon viatico per il futuro. Sempre notizia di oggi - non è dell'opposizione, lo ribadisco, ma sono le notizie che ci inducono i dubbi - è una agenzia a cui è correlato il *report* del Servizio studi della Camera che dice le misure definanziate, mancano le coperture. Il rapporto del Governo sui definanziamenti di misure previste dal PNRR, complessivamente pari a 15,9 miliardi, annunciate nei giorni scorsi non specifica quali saranno gli strumenti e le modalità attraverso i quali sarà mutata la fonte di finanziamento delle risorse risorse definanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le coperture ci sono o non ci sono? Poiché sono abituata a fare una lettura complessiva delle cose, noi oggi abbiamo registrato che purtroppo - e lo dico con rammarico sincero, perché noi vogliamo che l'Italia perché se aumenta il PIL stiamo tutti bene - il PIL si è bloccato, non stiamo crescendo come era previsto e abbiamo urgenze che si infilano in tutte le parti. Siamo sicuri che la legge di bilancio che ci apprestiamo a fare a breve ci permetterà di garantire queste coperture?

molto leggero, abbiamo una fotografia del Sistema sanitario molto complessa. Pertanto, mi sento di prendere a braccio il ministro Schillaci e andare a fare la questua per trovare le risorse della legge di bilancio e garantire le riforme che dobbiamo attuare. In questo momento tali risorse non ci sono: non solo non ci sono qui, ma perdiamo anche le risorse già stanziate dal PNRR, il che non è una cosa banalissima. In che cosa si traducono questi cambiamenti?

sono le case come primo luogo di cura e telemedicina. La telemedicina è ciò di cui stiamo parlando da tre anni come panacea e soluzione per l'assistenza domiciliare dei pazienti, per la medicina del territorio. Potrei continuare con l'elenco, ma vedo già che il microfono

Devo vedere ancora realizzati gli ospedali, i centri specialistici, gli istituti di ricerca finanziati con l'articolo 20, per 11 miliardi nel 2013,

Presidente, onorevoli colleghi, è stato di grandissimo interesse per tutti noi, almeno da questa parte dell'Aula e soprattutto per me, ascoltare una relazione così puntuale, esauriente e precisa da parte del ministro Fitto, e poter apprezzare l'enorme lavoro che è stato compiuto da lui e dalla sua eccezionale struttura di missione, del gruppo di *governance* che è stato creato al momento dell'avvio di questi lavori sul PNRR. È stato anche di grande arricchimento, dal punto di vista della conoscenza di questa materia così complessa, poter ascoltare da lui ancora una volta in quest'Aula, così come altre volte in altri contesti, una spiegazione e le motivazioni di quello che ha riguardato il PNRR e che riguarderà la terza e la quarta rata. Con grande pazienza ha voluto ripetere molte cose che sono state ascoltate da tutti noi e che, per parte di alcuni, si continuano a richiedere e forse a non credere; e questo credo che debba essere sottolineato. Il netto impulso dato venerdì scorso con il via libera al pagamento della terza rata da parte della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha coinciso con la visita a Washington del Presidente del Consiglio, una visita di eccezionale rilevanza. Entrambi questi eventi - sul piano europeo il primo e su quello atlantico il secondo - dimostrano e consolidano la credibilità, la fiducia e il ruolo riconosciuti con sempre più forte evidenza all'Italia. Abbiamo detto più volte in quest'Aula - e lo abbiamo affermato ripetutamente -che la fiducia dell'Europa, dei nostri alleati atlantici e di tutti i nostri *partner* si ottiene solo e soprattutto con l'affermazione concreta dei nostri valori europei e atlantici nel rispetto della legalità internazionale, degli impegni assunti dal Governo e del Parlamento. Sappiamo che per la nostra Nazione non è sempre stato così. La storia del dopoguerra non ha sempre pagine lucide e senza ombre, ma ora con questo Governo abbiamo sentito - e lo sente la gente giorno dopo giorno - che viviamo una storia diversa nei confronti dell'Europa anzitutto. La presidente Ursula von der Leyen ha detto chiaramente che l'Italia ha compiuto progressi notevoli nell'attuazione delle riforme e degli investimenti fondamentali inclusi nel PNRR. Nella sostanza per il PNRR REPower si tratta di risultati certificati ufficialmente, non da autoproclamati esperti di cose europee o da voci di parte, ma da chi ha la responsabilità politica e legale di farlo, la Commissione dell'Unione europea. Oggi sappiamo formalmente che la terza rata sarà erogata, ben 18,5 miliardi che entrano nel bilancio dello Stato. Ci aspettiamo perciò, da qui a dicembre, 35 miliardi di fondi europei e il Ministro ha spiegato con dovizia di particolari. Tutto questo dà la misura dell'impegno del Governo, sia nel merito che nel metodo. Il Ministro ha molte volte insistito nelle sue comunicazioni al Parlamento sulle modalità e sul contesto partecipativo nelle decisioni del Governo e in questo senso si è anche espresso qui più volte il Presidente del Consiglio. Il Il metodo deve essere sempre quello del confronto costruttivo, dell'interlocuzione fattuale e della sintesi tra comuni obiettivi, un metodo che è stato e continuerà a essere la linea seguita nei confronti delle istituzioni comunitarie, di quelle nazionali, regionali e locali. Proprio con questo metodo è stato possibile nei giorni scorsi risolvere, superare o anticipare una trentina di procedure di infrazione sulle quali ugualmente il Ministero guidato dal ministro Fitto ha ottenuto dei risultati molto considerevoli, un grande lavoro. La sintonia tra Italia e Unione europea è massima e lo è anche quella transatlantica. Adesso ci sarà da compiere l'ultimo sforzo: lavorare alle modifiche al Piano, modifiche importanti che destinano risorse a infrastrutture energetiche, ai trasporti, a innovazioni, istruzione e ricerca: 19,2 miliardi, di cui 2,7 di nuove risorse per potenziare settori strategici e l'autonomia energetica del Paese. REPowerEU fissa le linee per porre fine in maniera strutturale alla dipendenza dell'Unione europea dall'importazione di combustibili fossili dalla Russia *(Applausi)* e anche solo per questo motivo la sua rapida attuazione è un'urgente necessità ed è importante per rafforzare il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, per orientarci verso le riserve di gas del Nord Africa, della Libia, dell'Algeria, del Mediterraneo orientale, del Caspio, come l'Azerbaijan. Per fare questo è anche necessario agire per ridurre le strozzature che rallentano le forniture Sud-Nord, anche attraverso una linea adriatica che garantisca maggiori flussi alla Pianura padana, lo snodo nevralgico per popolazioni, imprese e consumi. Solo così riusciremo a sostituire completamente il gas russo e al tempo stesso valorizzare il nostro ruolo nel Mediterraneo quale *hub* europeo dell'energia. *(Applausi)*. Ci attendiamo settimane di lavoro dal Governo per attuare tutti questi impegni europei, ma ma sono convinto che il Governo, il ministro Fitto e la sua struttura siano pienamente in grado di ottenere il migliore risultato, quello che attendiamo, e che il Parlamento ne sarà tempestivamente informato. Una polemica c'è stata - ne ha parlato il ministro Fitto - sul trasferimento di fondi per progetti che non possono essere completati entro il 2026: il ministro l'ha spiegato e non ci torno sopra, ma sicuramente la data del 2026 è stata intesa come elemento per evitare di perdere risorse non più utilmente spendibili per il progetto Repower EU, realizzando progetti con altre risorse disponibili. Vi è infine una seconda dimensione, certo non meno importante, che integra il quadro di credibilità e di fiducia che l'Italia riscuote con questo Governo: - lasciatemelo definire così - comunicato congiunto tra il Presidente Meloni e il presidente Biden, nel segno di una grande amicizia e di una piena intesa tra l'Italia e gli Stati Uniti. Non sono fuori tema, quando qui, discutendo di PNRR, menziono questo comunicato congiunto, perché su moltissimi punti - vorrei dire su tutti - riguarda temi di prioritaria importanza anche per il PNRR, per la crescita dell'Europa, per la sicurezza dell'economia europea, della ricerca, dello sviluppo e della sicurezza dei cittadini italiani. *(Applausi)*. Gli aspetti più rilevanti del comunicato riguardano priorità condivise dall'Italia e dall'Europa, da un lato, e dall'amministrazione americana dall'altro: brevemente, gli esiti del vertice NATO di Vilnius, la riaffermazione dell'unità e della forza del legame transatlantico, il ruolo dell'Italia nel Mediterraneo. Il presidente Meloni ha detto,

Si tratta anche della visione italiana sull'Africa, sul piano Mattei, sui rapporti con la Cina: tutti aspetti di vitale importanza per la presidenza del G7. Un'ampia visione quella del comunicato congiunto, non certo frequente nella tradizione americana delle ultime presidenze - bisogna notarlo - ed è chiarissima la netta saldatura tra la dimensione europea e la dimensione atlantica, in un'impostazione marcatamente euro-atlantica della politica estera dell'Italia di oggi e di domani con il Governo del presidente Giorgia Meloni.

Ha facoltà di intervenire il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Fitto, al quale chiedo anche di esprimere il parere sulle proposte di risoluzione presentate. Presidente, in questa replica vorrei dare alcune risposte sulle questioni che sono state sollevate, cercando però - mi scuso con qualcuno che l'ha detto - di ribadire alcuni elementi che sono di merito, perché su molte questioni continuiamo ad ascoltare considerazioni generiche, ma non elementi che vanno nel merito delle questioni di cui ci occupiamo, né risposte puntuali rispetto alle cose che devono essere fatte. Sarò preciso e puntuale: ho preso nota dei vari interventi e

sia questa mattina alla Camera dei deputati che questa sera qui al Senato, un solo intervento che, entrando nel merito delle misure alle quali abbiamo fatto riferimento, abbia detto con chiarezza che non è vero che gli interventi previsti nel dissesto idrogeologico sono del 2010, 2016 e 2018 e che quindi non sono collegabili alla possibilità di essere realizzati all'interno del PNRR o che che i sei miliardi di euro collegati agli interventi dei piccoli Comuni nulla abbiano a che fare col titolo e l'obiettivo dell'intervento e sono collegati per il 75 per cento a interventi sotto i 100.000 euro, o che non è vero che circa un miliardo di euro, essendo interventi sulla viabilità, non è rendicontabile. Potrei continuare in questa direzione per dire che non c'è stato nessun collega che ha criticato il nostro lavoro e che abbia detto che stiamo sbagliando, perché con certezza assoluta

Parliamo di tutto, diciamo, facciamo e critichiamo, ma non c'è una sola considerazione che possa partire da un dato oggettivo, che è quello della data del giugno 2026. Vorrei ricordare a tutti che non è un dettaglio marginale e non è un problema di di rimprovero personale. Qualcuno l'ha interpretato male: non sono preoccupato del rimprovero di qualcuno in quest'Aula. Sono preoccupato del fatto che il Governo si trovi, fra qualche anno, per le ragioni che ho detto e che sono oggettive, a non poter rendicontare questi interventi e a dover restituire gli interventi che sono stati coperti rispetto al PNRR e quindi a perdere queste risorse. Questa è la preoccupazione che abbiamo, non il rimprovero da parte di qualcuno in quest'Aula. Questo lo voglio dire anche in riferimento ad alcune considerazioni anche inesatte. Si è fatto riferimento, lo dico al senatore di Nicita, con una serie di riferimenti anche simpatici, che colgo positivamente nel dibattito e nel confronto, al perché non abbiamo discusso sul REPowerEU. Esso è stato approvato in via definitiva ed è entrato in vigore il 1o marzo 2023, non un anno fa, come è stato detto, ma da qualche mese. Non ci sono altri Paesi che su questo abbiano operato delle procedure differenti rispetto a quelle che abbiamo costruito noi. Non è questa l'occasione, ma potremmo discutere anche dei Paesi che, rispetto all'adeguamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non hanno in alcun modo affrontato un dibattito parlamentare. Lo sto approfondendo in modo dettagliato e ne ho già dei riscontri. Questo per dimostrare che non possiamo fare le comparazioni come piace a noi, per provare a tirare la coperta dalla parte nostra, perché il dato a cui faccio riferimento è oggettivo. Soprattutto, il termine entro il quale presentare queste riforme è quello del 31 agosto 2023. del 31 agosto 2023. Siamo nei termini o siamo fuori termine? C'è una data e la stiamo rispettando. Abbiamo costruito un meccanismo di cui mi dispiace molto: mi riferisco al REPowerEU, che è uno strumento che abbiamo messo in campo in modo serio e credibile, con una grande opportunità per il nostro Paese, sul diverso terreno degli investimenti e delle riforme. Devo dire che mi dispiace anche la banalizzazione di alcune considerazioni sulle riforme che è stata fatta, perché all'interno del REPowerEU c'è la dimensione, dal punto di vista delle riforme e degli investimenti, che dà un respiro al nostro Paese, piaccia o non piaccia, e che è in linea, esattamente e con coerenza, con le previsioni del REPowerEU. sono fatti, non sono opinioni e non sono oggetto di grandi discussioni. Nell'ambito del REPowerEU, abbiamo infatti avuto delle indicazioni precise dalla Commissione europea. Tale provvedimento è attuato esclusivamente per dare una risposta alla grave crisi energetica, che abbiamo vissuto e che ho citato prima. Perché ignorarlo e non La Commissione europea ha previsto il capitolo aggiuntivo del REPowerEU e ogni Stato membro sta predisponendo il suo capitolo aggiuntivo, che modifica, insieme all'articolo 21 - e vengo quando si valuta l'opportunità di utilizzarlo. L'abbiamo utilizzato per le modifiche della quarta rata. L'articolo 21. Lo stiamo riutilizzando adesso e lo riutilizzeremo ogni qualvolta riterremo che sia compatibile con i tempi perché se si tratta di un articolo previsto da un regolamento europeo di attuazione del REPower, è fatto per essere utilizzato e se noi abbiamo un piano, quello italiano, il più grande piano a livello europeo per dimensione, superiore a tre volte la dimensione del secondo Stato membro come beneficiario, abbiamo qualche difficoltà in più in fase di attuazione? Abbiamo qualche problema oppure è tutto semplice? Io penso e temo che si sia persa un po' la dimensione che recuperiamo quando discutiamo delle leggi ordinarie o della legge finanziaria. Oramai viaggiamo su miliardi come fosse una cosa normale, ma quando apriamo il fascicolo di un miliardo, di sei miliardi o di cinque miliardi, dentro troviamo decine e decine di migliaia di progetti con tutte le complessità che il nostro Paese conosce. Vogliamo far finta che non ci sono? Vogliamo dire, come ho ascoltato, che è colpa del Governo. Noi, in nove mesi, avremmo fatto tutto questo caos rispetto ad una situazione che era perfetta come un orologio svizzero e che funzionava sotto tutti i punti di vista. Non è corretto dire questo perché non è vero perché non è vero e soprattutto rispetto anche al concetto che voi state mettendo in campo di voler costruire una dinamica nella quale il piano sia uno strumento di tutte le forze politiche, del Parlamento e del Paese (valutazione alla quale io accedo con piacere e convinzione), vorrei sottolineare che per poter fare questo bisogna realisticamente dare le soluzioni ai problemi. Ritorno sul punto, citando

un dibattito di questo tipo. A pagina 147 della proposta di revisione c'è scritto che il processo di riprogrammazione di revisione del Piano sarà finalizzato ad assicurare l'efficace attuazione degli interventi e l'integrale utilizzo delle risorse entro il 2026, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle obbligazioni assunte nei confronti dei soggetti attuatori e degli operatori economici, anche utilizzando a tal fine spazi finanziari disponibili come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Fondi strutturali di investimento europei, il Fondo per lo sviluppo e la coesione, il Piano nazionale complementare complementare del PNRR. È il raccordo di questi fondi. Come ho detto prima infatti, siccome nessuno dà la giustificazione e la risposta sui progetti che noi indichiamo come fortemente a rischio e per i quali vi è necessità di spostarli su altri programmi di investimento, non capisco quale sarebbe la soluzione. Va tutto bene? Dobbiamo lasciare tutto così come sta? Non dovremmo modificare questo programma perché le misure che noi abbiamo indicato ed individuato come critica rispetto a tutte le cose dette vanno bene? Non ho ascoltato questo. Perché qualcuno non si alza e dice: sì, va tutto bene, state sbagliando e non dovreste toccare nulla di queste misure? *(Applausi)*. Sarebbe utile ascoltare una considerazione del genere e che essa restasse agli atti per poterla poi ritrovare nel dibattito perché anche su questa vicenda del PNRR noi dobbiamo guardare guardare non solamente alla scadenza immediata, che abbiamo da qui ai prossimi mesi. Ho fatto l'esempio della quarta rata, ma non è sufficiente. Abbiamo modificato 11 obiettivi su 28, siamo dovuti intervenire rispetto ad una serie di difficoltà oggettive. Abbiamo parlato - voglio dirlo con chiarezza - sui giornali, esattamente come in questi giorni si sta parlando della rimodulazione, di asili nido. Abbiamo ascoltato per settimane e letto titoli di giornali in cui il Governo voleva cassare gli asili nido *(Applausi)* e oggi ci ritroviamo qui con questo Governo che ha presentato una modifica che ha consentito di superare un *target* intermedio per mantenere l'obiettivo finale e noi ci presentiamo qui con 900 milioni di euro aggiuntivi per mantenere questo risultato. *(Applausi)*. Questi sono i fatti

Andava bene all'epoca? Lo chiedo ai senatori che fanno il rivendicazionismo per i dati del Mezzogiorno d'Italia. Voglio ribadire e ricordare anche il Fondo per le opere, implementato per l'aumento del costo delle materie prime, che è un fondo di 6 miliardi di euro preso per intero dal FSC e ha creato le proteste che oggi ascoltiamo su un presunto rischio che non c'è (spiegherò anche perché non c'è), che noi stiamo portando avanti. Creare avanti. Creare allarmismo rispetto alla revoca del finanziamento è totalmente sbagliato, perché i programmi e i progetti vanno avanti nel momento in cui - l'ho ribadito in più circostanze ed è scritto a caratteri cubitali anche nella proposta di revisione - si completerà la fase di revisione della programmazione del PNRR e quindi queste modifiche saranno accettate o meno, perché ci accingiamo ad avanzare una proposta nei confronti della Commissione europea. Dovete anche compiere lo sforzo di leggere quello che abbiamo inviato in Parlamento. Il titolo è «Proposta di revisione», non abbiamo presentato una proposta immodificabile, ma abbiamo aperto un dibattito rispetto a questi temi ed è una proposta di revisione che si completerà dopo il confronto confronto che ha portato in questi mesi alla soluzione di diverse questioni e di diversi problemi e lo abbiamo evidenziato anche su tutte le questioni collegate al dibattito sulla terza rata e sulla quarta rata. Quando parliamo della revisione degli altri 144 obiettivi, vogliamo vogliamo mettere in sicurezza le misure del PNRR, vogliamo avere la certezza, come ho detto prima, che non ci sia un dubbio interpretativo rispetto, ad esempio, alla demolizione e ricostruzione degli asili, perché oltre ad aver riaperto il bando più volte nel passato, si sono previste la demolizione la demolizione e la ricostruzione. Quei posti, a livello interpretativo, sono considerati non nuovi posti, piaccia o non piaccia, e abbiamo dovuto fare questa correzione. Oggi stiamo correggendo questi elementi interpretativi su una serie di altre misure per evitare che tra sei mesi, un anno o un anno e mezzo accada di nuovo questo. È una posizione caotica? È una posizione che non ha senso? Spostare le risorse su alcuni interventi della coesione? La programmazione 2021-2027 ha come scadenza il 31 dicembre 2029, che è un tempo nettamente differente rispetto al giugno 2026. È una follia ipotizzare una valutazione complessiva, visto che la stessa Commissione europea ci invita a fare questo nel raccordo tra le politiche di coesione e le politiche del PNRR. E soprattutto, guardare alla oggettiva incapacità di utilizzo delle risorse nel passato, negli anni scorsi e nelle programmazioni in corso, non è un campanello d'allarme che ci deve far comprendere, tornando, per esempio, ad alcune modifiche che proponiamo, che non si può continuare con la proliferazione e la moltiplicazione di decine di migliaia di progetti, quando è necessario, come facciamo con il REPowerEU, mettere in campo alcuni interventi strategici di cui beneficerà il nostro Paese in via definitiva e strutturale su questioni per le quali abbiamo rischiato veramente di farci male, come come la grave crisi energetica dei mesi scorsi? *(Applausi)*. Sono questi i fatti che portiamo all'attenzione e lo voglio dire anche rispetto ad alcune altre considerazioni. Ho ascoltato l'intervento del senatore Spagnolli, sollevato il tema relativo alla *governance*, che ogni tanto ritorna, anche nell'intervento della senatrice Fregolent, *governance* è un decreto-legge che è stato approvato con voto unanime in Conferenza unificata dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. Lo vogliamo ricordare? Come si può sostenere che la *governance* vada in qualche modo contro il sistema delle autorità locali, quando è stata votata dalle autonomie locali in Conferenza unificata? Così come penso che sia importante sottolineare anche il tema relativo alla suddivisione del Fondo per lo sviluppo e la coesione e delle risorse europee per la coesione, da quelle nazionali e regionali. Ho spiegato prima - e vorrei ribadirlo - che

dal punto di vista dell'imputazione e che poi determinerà, quando si completerà il lavoro di verifica dell'utilizzo delle risorse 2014-2020, l'assegnazione con dei programmi precisi: non si limiterà alla sola assegnazione delle risorse, ma la accompagnerà a un elenco di progetti precisi e a un cronoprogramma in cui si stabilisce

ma è utile se vogliamo far camminare i progetti e se vogliamo evitare che accada quello che è accaduto e che sta accadendo relativamente al dissesto idrogeologico. Ho ascoltato alcuni colleghi dire che abbiamo tolto 16 miliardi dal dissesto idrogeologico,

riferiva alle obbligazioni giuridicamente vincolanti del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Io capisco le preoccupazioni, ma la previsione dell'eventuale definanziamento è stata definita e decisa con il decreto-legge n. 50 del 2022, all'articolo 56.

comportato delle differenti valutazioni dei rischi. Dico questo anche rispetto al piano urbano integrato, perché prima ho fatto un esempio concreto dei due piani integrati che hanno avuto una criticità oggettiva (Venezia e Firenze) e oggi noi stiamo verificando nella fase attuazione. Questo non vuol dire non finanziare il piano urbano integrato, ma evitare evitare che questo finanziamento possa ricadere nella tagliola della non rendicontabilità, della non ammissibilità e dei tempi che - lo ricordo sempre - sono quelli del giugno 2026. Questo è un riferimento totalmente assente in tutti i ragionamenti che ho ascoltato, ma per quanto ci riguarda è un elemento importante. Si è parlato di ritardi clamorosi, ma non ne è stato citato uno solo. Qual è un ritardo clamoroso imputabile al nostro Governo rispetto alle questioni di cui oggi noi stiamo parlando? Ho ascoltato con attenzione anche la senatrice Lorenzin e vorrei risponderle. Mi dispiace se una mezz'ora articolata di intervento non le va bene; io ho ascoltato il suo, proverò

questi interventi, garantendone il finanziamento, ma abbiamo anche previsto 250 milioni per acquistare i macchinari diagnostici, perché le case di comunità poi vanno riempite, altrimenti realizziamo solo i muri senza dare una prospettiva. Quindi nella proposta ci sono 250 milioni di euro che vanno in questa direzione. Penso sia importante sottolineare questo aspetto, perché sinceramente il dibattito che stiamo portando avanti per quanto ci riguarda sarà sempre concentrato sul merito delle questioni. E soprattutto, rispetto alle proposte che stiamo facendo, c'è una valutazione attenta delle proiezioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza anche e soprattutto rispetto alla scadenza finale. La politica non dà certezze, ma tendenzialmente sento di poter dire che questo Governo inevitabilmente debba porsi il problema di come

qualche rimprovero, come ho detto prima, ma il rischio serio di trovarsi di fronte al mancato raggiungimento di un risultato, al taglio della rata, all'incapacità di raggiungere il risultato e ottenere le risorse e soprattutto di fronte al rischio di vedere la mancata realizzazione di una serie di interventi sui quali continueremo a lavorare. L'articolo 21 lo utilizzeremo ogni qualvolta, in corso d'opera, ci saranno le condizioni e le necessità di utilizzarlo, perché è una previsione

in cabina di regia la scorsa settimana, per evitare di trovarci di fronte a rischi e problemi di questo genere. Chiudo con un ultimo elemento: visto che è stato citato il tema della *governance*, ci tengo molto a sottolineare che il numero di riunioni della cabina di regia, la fase di costruzione del partenariato, non semplice, che stiamo mettendo in campo rappresenta un ulteriore elemento importante di novità nella costruzione dei passaggi e della gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È una novità alla quale guardiamo con molta attenzione, perché oltre a dire che il Piano nazionale di ripresa di resilienza deve essere per il Paese, dobbiamo creare le condizioni, con gradualità e anche con qualche difficoltà, per coinvolgere tutti i soggetti e gli attori del nostro Paese, dal punto di vista sociale, datoriale oltreché ai livelli istituzionali. Questo sarà il metodo che porteremo avanti è con questo metodo sono convinto che, anche alla luce dei primi risultati raggiunti, avremo la capacità e la possibilità di superare le difficoltà che non mancheranno, ma per le quali sicuramente ci siamo attrezzando per poter dare risposte serie e chiare. Questo è l'impegno del Governo e questo è il contenuto della

per le comunicazioni sulla proposta di revisione del PNRR e sull'inserimento del capitolo del REPowerEU nel Piano stesso. Prima di iniziare, vorrei esprimere il mio plauso nei confronti del Governo. Qualche giorno fa è arrivato il disco verde della Commissione europea alla terza rata e alle modifiche sulla quarta rata. Parliamo complessivamente di 35 miliardi: 18,5 della terza rata e altri 16,5 della quarta. È un grande risultato per tutta la nostra Italia. Il coinvolgimento del Parlamento in tutti i passaggi legislativi previsti è un elemento di garanzia affinché le risorse del Next generation EU siano non solo messe a terra nei tempi previsti, ma soprattutto vengano utilizzate secondo una visione d'insieme in cui i diversi livelli istituzionali coinvolti sono chiamati a collaborare per raggiungere un obiettivo che è fare il bene del Paese. Allo stesso modo, maggioranza e opposizione, sebbene nel legittimo confronto della dialettica politica, dovrebbero salvaguardare un clima di confronto costruttivo e positivo, perché il bene dell'Italia e degli italiani viene prima di qualsiasi altra cosa. Utilizzando un'espressione di stampo degasperiano, c'è la necessità di "mettersi alla stanga" e di assicurare il progresso di tutto il Paese. L'accordo raggiunto in cabina di regia sulla revisione del PNRR e sull'inserimento del nuovo capitolo del REPowerEU ha ricevuto il plauso della Commissione europea. Parto dal capitolo del REPowerEU, fondi europei che l'Italia utilizzerà contro la crisi energetica, con investimenti a favore di famiglie e imprese. L'Italia non può più ritrovarsi a fare una manovra in cui due terzi delle risorse vengono utilizzate contro il caro energia. Dobbiamo sfruttare questi fondi per promuovere un percorso che porti il Paese verso l'autonomia energetica, anche e soprattutto attraverso il sostegno alle filiere produttive produttive *green* e all'efficientamento energetico del nostro patrimonio edilizio, sia pubblico che privato. Il nostro PNRR è quello più corposo in Europa, avendo l'Italia la somma più rilevante di risorse europee: 191 miliardi. C'è la piena volontà e il forte impegno di non perdere un solo euro di questo Piano. Abbiamo davanti a noi tre binari: il primo è quello del PNRR, che ha una scadenza al 2026, come ricordava più volte lei, signor Ministro; il secondo è quello del Fondo di sviluppo e coesione, con scadenza 2029: il terzo quello del Piano nazionale complementare al PNRR, con i suoi oltre 30 miliardi che, essendo risorse nazionali, non hanno un termine di scadenza finale. La scelta del Governo è stata lungimirante e quindi ponderata. L'obiettivo di oggi è realizzare tutti tutti gli obiettivi del PNRR e dunque spendere le risorse del Piano. Faccio solo un esempio su un tema che mi sta particolarmente a cuore, gli asili nido. Sono stati individuati, come ricordava lei

il Governo garantisce, dopo una interlocuzione con la Commissione europea, il finanziamento degli interventi, anche per quelli che sono stati espunti dal PNRR e su cui si è sviluppato un dibattito politico nei giorni scorsi e anche tuttora. I progetti in questione verranno coperti, come è stato evidenziato, ma con altre fonti di finanziamento, come ricordavo prima, come il Fondo di sviluppo e coesione e il Fondo complementare al PNRR. pone dunque ora una questione importante: parlo della riprogrammazione degli interventi espunti dal PNRR. Gli enti locali legittimamente chiedono e si aspettano impegni concreti, visto che hanno sottoscritto e portato avanti contratti e gare. Da quest'Aula oggi, con la proposta di risoluzione n. 5 condivisa dalla maggioranza, il Senato impegna il Governo, assicurando il pieno coinvolgimento di Parlamento, Regioni ed enti locali, a salvaguardare gli interventi espunti dal PNRR all'esito dell'aggiornamento del Piano, individuando le giuste coperture finanziarie mediante l'utilizzo sia delle risorse (Piano nazionale complementare), sia dei fondi strutturali e del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027. Parliamo di progetti che riguardano temi e questioni importanti, chiaramente è importante poi realizzarli concretamente. È una questione che riguarda tutta l'Italia, dai territori del Nord a quelli del Sud. Sbaglia chi fa di questa battaglia una questione di colore politico. Questo è un *target* che vale più di qualsiasi altro: è una partita per l'Italia e per tutti noi. Per queste ragioni, consapevoli che la revisione del Piano è un passaggio cruciale, come Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati voteremo convintamente a favore della proposta di risoluzione condivisa da tutta la maggioranza di centrodestra.

di darsi ragione rispetto a quanto affermato nell'introduzione. Devo dire con grande franchezza che qualcosa non torna,

di fronte a una scelta avendo solo due giorni a disposizione. Comuni di tutti i colori hanno posto il problema che sono state sottratte risorse, perché stiamo parlando di 16 miliardi tolti

ad esempio, che non viene condivisa la scelta di stralciare dal PNRR fondi destinati al dissesto idrogeologico e alla rigenerazione urbana, mentre Comuni e imprese sono fortemente impegnati in tutti i territori per portare avanti questi interventi urgenti e non procrastinabili, visti anche i

sulla questione del dissesto idrogeologico e sul rischio alluvioni e li spostiamo sull'energia? Poi tornerò sul tema. Francamente

non siete in grado di centralizzarle e l'unico modo è passare queste risorse all'ENI, alla Terna, alla Snam,

affrontando il problema della rigenerazione urbana e della messa in sicurezza sismica o il fatto che potremmo produrre non comprando

non si sta facendo, diciamocelo chiaro: questo è il dato fondamentale. Quindi, il problema è molto più di scelta di indirizzo politico.

il credito di imposta, ad esempio sulla questione del superbonus. Dall'inizio di gennaio, abbiamo solo messo delle toppe su questo terreno; i crediti incagliati sono ancora tutti lì e alcune delle aziende che hanno questo problema problema sono già fallite, mentre altre rischiano di fallire. I crediti incagliati non si sono disincagliati in questa situazione, perché la piattaforma che è stata fatta, su cui dovevano poggiare questi crediti, allo stato attuale non c'è e non

Sul terreno energetico, ho letto in questi giorni che denunciate quelli che aumentano a dismisura il prezzo della benzina o del gasolio. Ebbene, ieri ho fatto benzina e devo dire che, anziché 1,7 euro, ho pagato 1,859 euro, nel giro di due giorni, al mio paesello, non sull'autostrada. Quindi, anziché affrontare questi temi,

è intervenuto in quest'Aula a rendere informative sulle attività proprie delle sue deleghe. La ringrazio di questo, per il rispetto che ha sempre dimostrato nei confronti del Senato. del Senato. Tuttavia, non mi trovo sempre d'accordo con la qualità delle informazioni che mi vengono date e che ricevo, perché non sempre posso considerarle esaustive.

di esporre anche in dichiarazione di voto. Innanzitutto, signor Ministro, per mesi abbiamo ascoltato una narrazione da parte di questo Governo, che diceva che il PNRR era qualcosa che era stato ereditato dal precedente Governo

possiamo dire, sinceramente e oggettivamente, che forse questo PNRR non era stato scritto poi tanto male. La seconda considerazione che mi viene da fare è che, da questo momento in poi, questo è il vostro PNRR. Lo avete rimodulato, ce lo state presentando un po' *ex abrupto*, senza molto margine per discuterne e per approfondirlo. Tuttavia, da questo momento in poi, va da sé che questo è il PNRR che avete impostato voi e che volete portare avanti voi. Effettivamente, ha una nota caratteristica, che contraddistingue il vostro Governo: ha un'impostazione a carattere centralista, che è poi quella che contraddistingue la vostra azione di governo che, da un lato, si fa portavoce di un disegno di legge sull'autonomia differenziata e, dall'altro, imposta azioni di governo che non esito a definire centraliste. Siete partiti con la cabina di regia, con la necessità di accentrare il controllo, di verificare la spesa, eccetera e adesso, con queste ultime rimodulazioni, sicuramente operate ancor di più in modo centralista, perché tagliate le risorse. le risorse. Anche se lei, per carità, chiarisce che le tagliate nella misura in cui si tratta di interventi di entità e di valore ridotto, le tagliate a discapito degli enti locali e di chi, con queste risorse, ha investito e ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, che per un ente locale non è una cosa da poco. Nel momento

vi impegnate a fornire queste risorse, vi impegnate a trovarle, però francamente non c'è scritto da nessuna parte dove le troverete, né quando le troverete, a fronte di gare che sono state comunque pubblicate e di impegni che sono stati assunti e che adesso vanno onorati. Ancora una volta, sento parlare dei fondi di sviluppo e coesione, come un tesoretto al quale si deve attingere, anche in questo caso, per far fronte alla necessità di reperire risorse per garantire determinati interventi. Tuttavia, francamente mi chiedo e le chiedo: quante cose vuole fare questo Governo con i fondi di sviluppo e coesione (FSC)? Quante cose volete fare? Li volete utilizzare per il Ponte sullo Stretto. Li volete utilizzare per dare le risorse alle opere che definanziate col PNRR. Li volete utilizzare anche nel disegno dell'autonomia differenziata, per le materie di cui all'articolo 119 della Costituzione. Li volete utilizzare, come ha detto prima il ministro Musumeci in Aula, anche per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di lotta agli incendi boschivi. Francamente, è evidente che tutte queste risorse non esistono, non sono illimitate - è ovvio che non lo sono, dico una cosa scontata di per sé - ma soprattutto questa scelta è essa stessa la dimostrazione di un Governo centralista. Voi sapete perfettamente infatti che alle risorse del Fondo di sviluppo e coesione attingono gli enti locali e gli enti territoriali per orientare la loro spesa, per fare quegli interventi che non hanno più possibilità di fare nel momento in cui il Governo non dà più loro le risorse. Quindi si utilizzano i fondi di sviluppo e coesione. Se però io Governo attirò a me queste risorse o le indirizzo verso spese che ho deciso io va da sé che l'autonomia è finita.

ministro Fitto, continuo a osservare, nonostante le sue repliche, e mi colpisce che siano stati definanziati progetti per la messa in sicurezza del territorio e la prevenzione delle conseguenze del cambiamento climatico.

giovedì scorso abbiamo votato il decreto-legge alluvioni. Perché li stiamo togliendo dal PNRR? Perché non erano finanziabili, perché non erano rendicontabili o perché erano in ritardo sui tempi di esecuzione? Noi questo non l'abbiamo capito e soprattutto non sappiamo come sia stata fatta questa valutazione. Ciò ci impedisce poi effettivamente di fare un controllo preciso e puntuale e di comprendere se questa scelta sia o meno condivisibile. Con

come faranno queste famiglie a goderne nel momento in cui gli sgravi per chi ha redditi bassi pongono sempre il problema della capienza fiscale. È un tema sul quale voi comunque ancora non avete dato le risposte attese. Che cosa faremo? Ricorreremo nuovamente alla cessione del credito alle banche? Lo stesso sistema per il quale ci sono milioni incagliati nelle banche e queste ultime non concedono più il credito perché non hanno neanche loro più un modo di gestire questi crediti incagliati? Tali crediti sono diventati una zavorra tanto per le banche, quanto per gli operatori. Questa è una delle tante domande alle quali non ho trovato risposta nelle sue repliche. Mi chiedo altresì cosa succederà adesso con le imprese che facevano fede sui nuovi tempi di pagamento della pubblica amministrazione e cosa si intende fare per ridurre i tempi di attesa delle cause nei tribunali civili. E ancora le chiedo, sempre in risposta alla logica centralistica, se sia possibile pensare che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome debba dare un riscontro alla rimodulazione in appena quarantott'ore. Mi sembra un tempo troppo ristretto. Insomma, in verità, ancora una volta il Parlamento viene messo davanti al fatto compiuto, con l'aggravante che non vengono fornite informazioni precise e dettagliate che almeno, stringendo i denti e lavorando, come si suol dire, a pancia bassa, ci consentano di avere una piena cognizione.

(ben 275 milioni) per la tratta ferroviaria Palermo-Catania e per quella Dittaino-Enna, che vengono stornati a favore del collegamento Napoli-Bari. Questo non può essere un *derby* tra città del Sud; non può essere un *derby* in cui Napoli-Bari si contrappone a Palermo-Catania. Non ci sta bene, non è una soluzione praticabile e io la invito nuovamente a onorare gli impegni che ha preso con noi in quest'Aula e mantenere ferme le risorse per il Sud.

dopo disfa quello che ha fatto il Governo che c'era prima, anche se alcuni partiti del Governo che arriva dopo erano anche nel Governo che c'era prima. La seconda è è che, quando si passa dalla chiacchiera all'esecuzione e all'implementazione, l'Italia si scontra con il più grande problema, anzi, forse con l'unico determinante, cioè con il fatto di non saper mai gestire, implementare, amministrare e spendere. Non è il problema di una maggioranza, come dimostra l'andamento dei fondi europei nel tempo. È ormai un problema di sistema Paese, perché sono trent'anni che stiamo a urlarci addosso «fascisti» e «comunisti», senza mai concludere niente, da un punto di vista pragmatico. Qui ho sentito anche un po' di cose surreali, come ad esempio che il PNRR di Mario Draghi era un'accozzaglia utopica. Mi permetto di suggerire un certo grado di attenzione, dato che Draghi nei primi sei mesi del 2022 ha speso esattamente dieci volte quello che avete speso voi nei primi sei mesi del 2023. Possiamo fare finta che ci siano altre ragioni, ma resta il fatto che il Governo Meloni ha fatto un'assunzione di responsabilità dicendo il PNRR così com'è non va e che la *governance* così com'è non va, pertanto vuole cambiarli: da questo momento, come diceva la collega Musolino, ve ne assumete la piena responsabilità, ma avete messo tutto sul piatto; non avete messo sul piatto la credibilità della vostra maggioranza, avete messo sul piatto la credibilità dell'Italia intera. Aggiungo due cose. Lei ci Ministro, di dimostrare che i fondi del 2019 sul dissesto idrogeologico possono essere spesi con il PNRR. No, Ministro, non funziona così.

che vi piaccia il PNRR, perché prima non vi piaceva e quindi è un fatto importante. Trovo positivo che si arrivi a conoscere un piano di modifiche, perché avete chiesto le modifiche in campagna elettorale ed è passato quasi un anno e oggi oggi finalmente le conosciamo. Trovo positivo il pagamento della terza rata e della quarta rata, che vuol dire che lei ha fatto un buon lavoro su questo, Ministro, e io ho piacere di riconoscerlo, perché non remo mai contro il Paese e contro il Governo che rappresenta non una parte degli italiani, ma anche il sottoscritto. Trovo molto positivo che il Governo abbia finalmente chiuso il REPowerEU, mettendoci quello che avevamo chiesto, cioè 4 miliardi di transizione 5.0 come crediti di imposta per far fare investimenti alle imprese su energia e ambiente. Il resto però poi è un po' deludente, non solo per le ragioni che le ho detto prima, ma anche perché il il PNRR si compone di 155.000 bandi, di cui 133.000 bandi sotto il milione di euro. Ci sta assolutamente che lei dica oggi che una parte di quei progetti non può andare a buon fine, ma manca la parte costruttiva: e quindi cosa facciamo? Qual è la vostra idea di scuola? Qual è la vostra idea di sanità? Per esempio, proprio perché vogliamo essere costruttivi, le abbiamo proposto di indirizzare sul rifinanziamento per intero di industria 4.0 tutto il pacchetto dalla formazione super e iperammortamento, con i soldi del PNRR. Ma sa perché? luogo perché, se non siamo in grado di spenderli, facciamoli investire alle imprese che hanno in questo momento margini molto elevati di profitto e possono investire; in secondo luogo, perché in questo momento abbiamo un ciclo economico che va in giù e gli investimenti li possono sostenere; perché in America c'è una cosa che si chiama Inflation reduction act, che finirà per spendere 1,3 trilioni per le imprese con crediti d'imposta. Questo perché la normativa sugli aiuti di Stato consente oggi agli altri Paesi che hanno più capacità fiscale di investire, dunque facciamolo. Ve lo abbiamo proposto e stimato, vi abbiamo dato i numeri, vi abbiamo detto tutto quello che si può fare; cerchiamo di metterceli, questi soldi, altrimenti continuiamo a dire che Draghi era inaffidabile, che quell'altro era cattivo e che mio zio era pure peggio, però poi che facciamo, dove sono le idee? Su questo punto mi faccia dire qualcos'altro rispetto al dibattito surreale che facciamo in Italia sul clima. La prossima settimana, per esempio, arriverà un'ondata di freddo, ergo potete già immaginare che i giornali dedicheranno 28 pagine al fatto che fa freddo e non fa caldo; però avete deciso che è vero che c'è il cambiamento climatico, almeno così formalmente l'avete deciso. Siete in disaccordo sulle politiche europee, anche io in parte penso che Timmermans sia stato un disastro umano, ma poi c'è un punto:

Possiamo per esempio provare a trovare una convergenza almeno su questo, cioè sul fatto che occorra una legge che può essere finanziata dal PNRR, che metta dentro tutti gli interventi che vanno fatti non solo per il dissesto idrogeologico in condizioni normali, ma per quello che si verifica in condizioni estreme? Basta infatti una piccola modifica di un grado e mezzo per moltiplicare gli eventi estremi. Possiamo farlo ricostruendo la struttura di missione che avevamo previsto e istituito con il Piano casa Italia? Possiamo farlo anche cambiando il contenuto e mettendoci nuove

non vogliamo chiudere le porte a una discussione, però le dico un punto: questa volta, ci asteniamo anche per il lavoro che lei ha fatto sulla terza e quarta rata, ma da adesso in poi la fuffa è finita e lei ci deve dire come vuole spendere i soldi ed è responsabile se questi soldi non vengono spesi. È iscritto a parlare il senatore De Poli. e possiamo certamente confermare che le intenzioni del Governo vanno esattamente nella direzione che la Lega ha sempre auspicato: non possiamo sprecare nemmeno un centesimo dei soldi che abbiamo chiesto all'Europa e che in parte dovremo ripagare. Il via libera della Commissione europea al pagamento della terza rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza e l'approvazione delle modifiche di alcune scadenze della quarta smentiscono le voci di chi avrebbe preferito un fallimento di questo Governo sui tavoli europei, anche se a pagarne le spese sarebbero stati gli italiani. Possiamo anche non condividere alcuni metodi degli uffici della Commissione; possiamo non essere d'accordo su alcune iniziative, ma c'è un dovere istituzionale di confronto e di ricerca di un'intesa al quale nessuno vuole venire meno, a Roma come a Bruxelles. La Commissione europea ha riconosciuto gli sforzi e i risultati ottenuti dall'Italia e questo patrimonio di reputazione sarà utile anche per le mediazioni che verranno. Il lavoro svolto in questi mesi conferma l'intenzione di utilizzare al meglio le opportunità offerte dal PNRR e insieme, Governo e Parlamento, Parlamento e Governo, abbiamo anche continuato ad accompagnare gli investimenti del piano con le riforme necessarie ad accelerare la realizzazione delle opere e a modernizzare il Paese: penso al codice degli appalti, ma anche alla riforma della giustizia, agli interventi sulla pubblica amministrazione e alla delega fiscale che ci apprestiamo a esaminare nei prossimi giorni. Il PNRR è un grande acceleratore, da questo punto di vista. Vogliamo rendere l'Italia un Paese con meno burocrazia, con una pubblica amministrazione più efficiente e con una giustizia rapida e certa (speriamo, almeno questo). Sono impegni che abbiamo preso con l'Europa, ma che prima di tutto abbiamo preso con i nostri elettori e noi gli impegni vogliamo mantenerli. Il Governo si è assunto anche l'onere di riorganizzare e gestire il Piano nazionale di ripresa e resilienza e di individuare i problemi che ne avrebbero potuto ostacolare la completa realizzazione. Lo Lo stesso lavoro è stato fatto per i fondi nazionali ed europei delle politiche di coesione, che ancora oggi troppo spesso non vengono spesi o, peggio, in molte parti d'Italia sono sprecati in opere e attività che non servono allo sviluppo e a migliorare la vita dei cittadini. Si è trattato di una grande responsabilità e di un notevole impegno, per il quale vogliamo ringraziare il Ministro. Ora però, Ministro, c'è bisogno di un ulteriore sforzo per rendere disponibili al più presto alle Regioni e ai Comuni tutte le risorse previste per realizzare un programma complessivo di sviluppo e di modernizzazione del Paese. Tenendo fermi i principi alla base del PNRR, che erano stati concordati con la Commissione europea, il Governo aveva il dovere di aggiornarne i contenuti, per adattarli alle diverse condizioni in cui ci troviamo oggi: la guerra in Ucraina, l'aumento dei costi delle materie prime e i primi riscontri sull'attuazione di alcune misure, a partire da quelle in essere. Da qui nasce l'esigenza di modificare il Piano, non certo da una volontà ingiustificata del Governo o di questa maggioranza: prima della volontà c'era la necessità di modificare il Piano e questo è stato fatto *(Applausi)*, anche perché, durante le durante le trasmissioni televisive, sento anche i colleghi della minoranza dire che il Piano doveva essere modificato, quindi non si possono sentire delle cose nelle trasmissioni televisive e altre cose in Aula. Per questo garantiamo al Governo il sostegno della Lega nella trattativa che si aprirà nei prossimi mesi a Bruxelles e ci auguriamo che si possa arrivare a un'approvazione rapida e senza quei preconcetti che a volte abbiamo dovuto superare tra gli uffici della Commissione europea. Ce lo auguriamo per il nostro Paese, con la P maiuscola, perché è l'Italia che ha bisogno di queste opere, non il Governo o la maggioranza; è l'Italia, e l'Italia, signor Presidente, è fatta di tante esigenze e tante potenzialità, a volte anche molto diverse tra loro. Il PNRR deve puntare a soddisfare queste esigenze e valorizzare queste potenzialità e per farlo è fondamentale il ruolo di chi conosce più di tutti il nostro territorio, in particolar modo i nostri enti locali. locali. Per questo, mentre ringraziamo il Ministro per essere qui oggi a confrontarsi con il Senato dopo essere stato alla Camera, l'invito che gli facciamo è quello di coinvolgere maggiormente e al meglio i rappresentanti delle istituzioni territoriali, perché in molti casi sono loro a dover mettere a terra le opere contenute nel PNRR e in buona parte lo stanno già facendo. Sono loro che ci mettono la faccia davanti ai cittadini. Sono questi stessi enti locali, a cominciare dai Comuni, che hanno chiesto garanzie sulla rimodulazione delle riforme che erano state assegnate e devono avere risposte puntuali in tempi brevi per garantire che i cantieri già aperti possano andare avanti e quelli programmati possano partire. Si badi bene, non stiamo discutendo di richieste astratte. Abbiamo visto nei mesi e anche nei giorni scorsi quanto il paesaggio italiano sia fragile e quanto ci sia bisogno di investire in manutenzione, in opere di protezione del territorio, come abbiamo visto prima prima con il ministro Musumeci, ma anche nella modernizzazione delle infrastrutture, nella vera transizione energetica e in quella digitale. Se i vincoli inizialmente posti dal PNRR non sono adatti alla realizzazione di queste opere, individuiamo il prima possibile le fonti di finanziamento alternative, perché stiamo parlando di interventi che non possono aspettare e per i quali i sindaci e i Presidenti di Regione hanno l'urgenza di dare risposte ai loro cittadini. Utilizziamo al meglio, quindi, tutte le risorse a disposizione, tenendo presente che a volte queste prevedono ripartizioni territoriali diverse da quelle immaginate dal PNRR, quindi, laddove i fondi per la coesione non riuscissero a coprire del tutto le esigenze di alcune Regioni, queste non potranno e non dovranno certamente essere sacrificate, ma bisognerà trovare altre fonti di finanziamento. Vogliamo essere chiari anche su una cosa e sappiamo che il Governo condivide questa considerazione: spostare le opere dal PNRR ad altri piani di intervento non vuol dire rimandarle all'oblio. Questo per noi è fondamentale, Ministro. Nessuno vuole sfuggire al bisogno di modernità del Paese; evitare la tagliola delle scadenze che l'Europa impone non significa che quelle opere non si faranno mai o che possiamo prendercela comoda e di questo devono essere consapevoli tutti, gli organi statali, gli enti territoriali e le imprese. Oggi più che mai abbiamo bisogno di uno sforzo collettivo e di remare tutti nella stessa direzione, senza inutili polemiche. Sappiamo che se qualcuno in qualche ufficio si mette di traverso, se i ricorsi bloccano per mesi i lavori, se chi ha l'opportunità e le risorse da investire non lo fa o lo fa in ritardo, a pagarne le spese sarà l'intero sistema Paese, e non possiamo permettercelo. Siamo stati tra i primi a dire che sarebbe stato giusto destinare alle imprese le risorse del PNRR che non si sarebbe riusciti a spendere, quindi siamo soddisfatti della scelta fatta dal Governo in questa direzione. Le nostre piccole e medie imprese hanno bisogno di investire nell'innovazione e nell'efficientamento energetico e molte di loro lo stanno già facendo o sono pronte a farlo. In particolare, signor Ministro, voglio sottolineare positivamente le risorse aggiuntive destinate al comparto agricolo per finanziare i contratti di filiera, migliorare l'efficientamento energetico e favorire la produzione di biocarburante da fonti agricole. Si tratta di una scelta coerente con quanto l'Italia sostiene in Europa e a proposito della necessità di introdurre anche il *biofuel* tra le fonti energetiche previste nella cosiddetta direttiva sulle auto *green*. In conclusione, abbiamo di fronte a noi un'opportunità che l'Italia non ha mai avuto prima d'ora. Mettendo insieme in un grande progetto comune il PNRR, il REPowerEU, i fondi per la coesione e gli investimenti nazionali, potremmo guidare la vera transizione ecologica e digitale, garantire crescita e lavoro, migliorare i servizi e le opportunità per le famiglie e valorizzare le potenzialità dei territori. Per riuscirci, tutti gli ingranaggi della macchina devono funzionare al meglio e a questo servono le riforme. Signor Ministro, non abbiamo possibilità di sbagliare. I cittadini ci giudicheranno sulla base dei risultati che riusciremo ad ottenere e anche la credibilità internazionale del nostro Paese uscirà ulteriormente rafforzata dal successo di questo Piano. Possiamo dimostrare a tutti, all'Europa e al mondo, che l'Italia è orgogliosamente all'altezza anche delle sfide più difficili e che questo Governo saprà guidare il Paese verso un traguardo mai raggiunto prima. Buon lavoro a tutti.

ministro Fitto, avendo ascoltato il suo intervento e avendo letto anche la relazione con le proposte di revisione del Piano, noi non possiamo che apprezzare, come già qualcun altro ha ribadito, l'approccio assolutamente pragmatico che lei ha dato al tema. Lo so, vedere alcune rimodulazioni può creare a prima vista un certo disagio, perché le misure stornate sono importantissime per il nostro Paese e perché gli enti locali forse sono la struttura principale in un ordinamento istituzionale, però lei, allo stesso tempo, ha chiarito che non ci sarà nessun definanziamento e che, anzi, si metteranno in sicurezza quegli investimenti. Sono tutte opere assolutamente prioritarie e positive in chiave ambientale per il nostro Paese (quelle sul dissesto idrogeologico, quelle che riguardano i Comuni per la rigenerazione urbana e per la resilienza e quelle sui piani urbani integrati e sull'efficientamento energetico). Per alcune di esse sono già in corso dei lavori

La revisione del Piano quindi non è certamente un vuoto e retorico esercizio di stile voluto dal Governo, come qualcuno ha detto, ma semmai dimostra questo impegno diuturno e quotidiano, direi incessante. Ricordo i quarantasette incontri anche

Ci sono correzioni tecniche e formali, modifiche necessarie, provocate dall'aumento dei prezzi, soprattutto delle materie prime nel settore delle costruzioni, opere da sostituire, perché calate da altri finanziamenti e da altri piani all'interno del PNRR e non coerenti, quindi, con i criteri di rendicontazione, il alcuni altri parametri previsti dal PNRR. Ci sono problemi con i definanziamenti che ci sarebbero per queste opere, se si portassero avanti questi progetti, e anche la scadenza temporale, come lei ha più volte ripetuto,

uno è portare a casa questi investimenti, che sono assolutamente necessari per il nostro Paese; l'altro è finanziare e rafforzare, con i finanziamenti, il REPowerEU.

Il parassita prende tutto e non dà nulla. L'ospite dà tutto e non prende nulla. E il primo dovere di un'etica del futuro è immaginare gli effetti a lungo termine delle nostre scelte e lasciarsi influenzare anche delle ipotesi più negative. La paura, per esempio, e la preoccupazione possono ispirare alcune scelte delle quali si discute in campo ambientale. Il nostro ministro Pichetto Fratin, per la sua sensibilità e per la preoccupazione che ha dimostrato anche davanti a una ragazza che aveva paura, ha tenuto un comportamento assolutamente irreprensibile, che ho molto ammirato. molto ammirato. Dall'altro lato, abbiamo gli enti locali, che sono penalizzati nel nostro Paese da un eccessiva burocrazia, che rende quasi impossibile rispettare le scadenze temporali. Lo ha detto anche lei: già con i fondi di coesione e sviluppo e con tutti gli altri finanziamenti che non

troppo eccezionali, in una Nazione che, fino a pochissimo tempo fa, aveva una pubblica amministrazione ingessata, goffa ed elefantiaca. Forse non tutti lo ricordano, ma per il primissimo slancio di modernizzazione di questo Paese c'è voluta una tragedia immane, che ancora agita le nostre coscienze, quella del ponte Morandi. Per la sua ricostruzione sono state adottate le prime deroghe al codice degli appalti, introdotte alcune semplificazioni, rivisti i classici schemi di responsabilità erariale. Grazie all'attuale Governo e al ministro Zangrillo sono state introdotte recenti riforme che mirano a una pubblica amministrazione più moderna dal lato delle risorse umane. Quindi è arrivata, signor Ministro, la proposta di rimodulazione grazie ad una visione di insieme che è resa possibile dalla sua *governance*. Ho sentito parlare della *governance* e del tempo che si è perduto. Ma proprio grazie a quello che oggi lei ha costruito, mettendo sullo stesso tavolo chi si occupa di PNRR e chi si occupa anche degli altri fondi (dai fondi di sviluppo (dai fondi di sviluppo e coesione al fondo complementare), è possibile ed è stato possibile non perdere risorse assegnate ai Comuni e realizzare complessivamente i programmi di investimento e le riforme che sono più che mai necessarie per il nostro Paese. La cabina di regia di cui lei ha parlato è stata costituita proprio per volere di questo Governo. Essa è in grado di monitorare gli atti e i fatti conseguenti, seguendo il metodo antico della concertazione. Si parla con tutti gli attori in campo, con le Regioni, con le Province, con i Comuni, con i sindacati, con le associazioni datoriali e con le associazioni di categoria; un continuo confronto anche con il Parlamento. Dopo i necessari approfondimenti, ora ci troviamo alla proposta di spostare queste risorse su alcune misure meno problematiche,

Con queste risorse si interviene concretamente con investimenti sulla rete di energia. È inutile che i privati facciano investimenti sugli impianti produttivi di fotovoltaico, di impianti solari, quando non hanno a disposizione la rete per gli allacciamenti. Si interviene sulla transizione verde, sull'efficientamento energetico, ma anche sulle filiere industriali di cui parlava prima il senatore Calenda, che sono ritenute strategiche. Accanto a questo ci sono le riforme del settore, per rendere meno conveniente l'utilizzo dei fossili e incentivare l'utilizzo del biometano e delle fonti rinnovabili. Si punta anche ad un testo unico - questo è qualcosa di straordinario - sulla legislazione delle fonti rinnovabili: questo sarà un compito anche del Parlamento. Ci aspetta un volano nella nostra economia per la creazione di posti di lavoro: l'ultima manovra di bilancio valeva 35 miliardi, di cui 21 utilizzati per affrontare il caro bollette. Adesso, con questo programma, avremo degli interventi strutturali che potranno recuperare il *gap* che il nostro Paese avrà. Questa iniezione di fondi, inoltre, darà un impulso consistente anche alla nostra economia, già da ora, già a partire dalla terza rata e poi dalla quarta; aprirà nuovi cantieri e ciò significa anche significa anche muovere settori indotti: quindi, non solo diversificazione delle fonti, ma anche efficienza energetica delle reti e aumento della produzione delle fonti rinnovabili. Poi c'è il caso del 110 per cento: abbiamo visto che così com'era non ha funzionato ed ha alimentato milioni di frodi. Oggi avremo a disposizione un meccanismo con detrazioni fiscali più limitate, ma destinate a redditi bassi e ai giovani, come lei ha sottolineato. Altri 3,6 miliardi sono per il patrimonio immobiliare pubblico e privato. Sono tanti gli interventi. Sul caso degli asili nido non mi trattengo, perché è stato più volte sottolineato. Ecco perché a noi queste queste modifiche sembrano giuste, ma anche tempestive e centrate. Chiediamo un impegno da parte del Governo a destinare maggiori risorse ai Comuni e agli enti locali rispetto a quelle che erano già complessivamente previste, da spendere anche nei prossimi anni. Alla fine il problema è quello

e le risorse che lei ha indicato nel Fondo di coesione e sviluppo per l'80 per cento devono essere destinate lì. Lei ha citato anche dei casi in cui nel passato sono state sottratte. Allora ci vuole un progetto mirato che ponga rimedio a ritardi di anni in tema di investimenti. L'idea di una ZES unica, una zona economica speciale unica, può essere di accompagnamento importante rispetto alla possibilità di accedere concretamente a questi investimenti e a realizzarli, perché con gli sgravi fiscali e le semplificazioni nel Sud potrebbero partire, questa volta concretamente, gli investimenti. stringiamoci tutti intorno a questa occasione unica di crescita del nostro Paese. Restiamo dalla stessa parte, come giustamente richiesto anche dal presidente Mattarella. È difficile forse per le parti politiche; ho sentito molti proclami, mentre dalla parte del Governo e del Ministro delle osservazioni nel merito molto precise. Noi vogliamo sostenere il Governo e per questi motivi Forza Italia valuta positivamente la comunicazione del ministro Fitto e le proposte di revisione del Piano italiano presentate dal Governo Meloni. signor Ministro, colleghi, stavo iniziando dicendo che era bellissima l'immagine che arrivava dai banchi del Governo, anche se ora vedo il ministro Calderoli andar via. Sembra un quadro di Escher, di quelli impossibili: da un lato il centralismo sovranista, dall'altro l'autonomia secessionista. *(Applausi)*; quindi l'impossibile che sta vicino. Presidente, mi associo alle parole di vicinanza e solidarietà che in quest'Aula sono state espresse più volte, nelle dichiarazioni rispetto ai ai Gruppi Civici d'Italia-Noi moderati-MAIE, Forza Italia e Lega, per le parole stranamente sopra le righe di un senatore molto mite che apprezzo molto, il senatore Matera, quando ha detto che il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un'accozzaglia ereditata dai nostri predecessori: ecco, quindi anche da voi. Non posso che rinnovare un moto solidaristico verso chi ha scritto il Piano e oggi una parte della maggioranza dice che è un'accozzaglia di progetti vuoti. Così come, rivolgendomi al ministro Fitto, che ha anche dispensato consigli alle opposizioni - ma su questo tornerò - dico: sia più ottimista rispetto alla capacità del Governo e della maggioranza di semplificare il Paese e di migliorarlo. Dire oggi che, certamente, blocchi interi di misure e di progetti del PNRR non si riusciranno a fare - ma qui tornerò, perché lei ha chiesto delle risposte e sarò molto puntuale nel dargliele - esprime anche un po' di sfiducia verso questa maggioranza e questo Governo. Forse da parte vostra non lo meritano, anche se da parte nostra certamente sì.

anche altre volte in quest'Aula. Do atto della sua presenza costante: anche oggi, nemmeno per una pausa di qualche minuto si è allontanato dall'Aula, né questa mattina, né questo pomeriggio; quindi cercheremo di liberarla presto, anche per questioni organiche. però, ad esempio, rivendichiamo con forza uno di quelli che ritengo sia tra i più grandi successi del Governo di centrosinistra, cioè del Conte II della scorsa legislatura, ossia l'aver ottenuto i fondi del Piano non può essere derubricato a un fatto tecnico rispetto ai parametri. Lei ha ragione: i parametri erano quelli e, quindi, le cifre che abbiamo potuto ottenere, in parte a fondo perduto e in parte a prestito, sono legate a quei parametri che lei ha citato.

contro il Governo italiano *(Applausi)* quando in Europa cercava di battersi contro la Francia, la Germania, i Paesi del Nord e quelli di Visegrad, che non volevano il debito comune europeo Il successo e la credibilità di quel Presidente del Consiglio e di quella maggioranza stanno non nei parametri di riferimento, ma nel fatto che ha convinto, grazie anche al lavoro fatto con la Spagna e con il Portogallo in particolare, che c'era la necessità di un cambio di paradigma nell'atteggiamento europeo nei confronti della pandemia e di una crisi simmetrica, che andava colpendo tutti i Paesi in modo più o meno profondo. Quella è stata la vittoria e quei parametri sono stati frutto del negoziato, perché c'erano *n* parametri utilizzabili, ma guarda caso sono stati presi i tre parametri che più hanno favorito il nostro Paese. Lei ha citato spesso l'esigenza di entrare in profondità e nel merito. Avevamo chiesto che questo momento molto importante, le sue comunicazioni, le dichiarazioni di voto, la discussione generale e le risoluzioni, fossero accompagnati da una procedura più ampia nelle Commissioni quindi con l'affidamento alla 5a Commissione in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva - per approfondire ancora di più le modifiche, che in parte, peraltro, possiamo dire di condividere per alcuni aspetti, soprattutto per quanto riguarda la parte di REPowerEU. Non ho capito perché non c'è stata questa possibilità e mi auguro, siccome dalle sue parole traspare l'evidenza che c'è ancora una fase di concertazione con la Commissione rispetto a tali modifiche, che questa possibilità ci venga data o prima del 31 agosto, o prima delle decisioni finali sull'approvazione delle modifiche al Piano. La questione di metodo non è indifferente, anche per entrare nel dettaglio di alcune cose. Lei ha detto non c'è un rischio di definanziamento, ma ci sono misure e progetti puntuali che nulla c'entrano con gli obiettivi del Piano. Non siete però entrati in questo dettaglio, perché avete tagliato le misure con l'accetta. Sul tema della rigenerazione urbana, sul tema dei piani urbani, sul tema del dissesto idrogeologico non avete differenziato i progetti che stanno iniziando da quelli che probabilmente non si riusciranno a portare a termine entro il 30 giugno 2026.

Questi, al momento, sono in quel pacchetto che viene stralciato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché fanno parte dei 3 miliardi di euro che sono stralciati integralmente. Lei ci dice che saranno rifinanziati con i fondi FSC, che però ad oggi non sono ancora approvati con delibera del CIPES.

Lei potrà darci tutte le garanzie, ma forse una fase di condivisione preliminare rispetto a questo documento era necessaria con gli enti locali, i Comuni e le amministrazioni locali. sono state espresse pure dal Centro studi del Senato che, nonostante in poco tempo abbia fatto un *dossier* molto preciso, dice che non c'è certezza rispetto a quelle fonti di finanziamento. Veniamo ad alcuni aspetti sul REPowerEU. Intanto io non posso che ringraziare il Governo che anche nella relazione dice con forza che il superbonus non è stata la più grande truffa della storia del Paese.

Vengono finanziati interventi di efficientamento energetico sul modello del superbonus, e ciò è positivo. Sono altresì molto felice che anche il senatore Calenda dia atto che il il piano Industria 4.0 che funzionava aveva però il limite sugli ammortamenti e che, grazie al piano Transizione 4.0, che è passato ai crediti di imposta, si è consentito al mondo industriale di investire in modo profondo in innovazione, nuove tecnologie e tecnologie *green*.

del nostro Paese di addivenire a una indipendenza energetica. Io vedo un progetto per trasformare questo Paese in un *hub* energetico che è una cosa ben diversa, perché significa che il nostro Paese diventa il punto di collegamento tra dove si produce energia (probabilmente Nord Africa) e dove si consuma (cioè al Nord e verso gli altri Paesi).

La parte che consente al nostro Paese di produrre energia da fonte rinnovabile è troppo debole nel REPowerEU e in questo senso va anche la nostra risoluzione.

il Piano che voi criticate tanto, ma che modificate per il 6,76 per cento complessivo, diventa il vostro Piano. Noi non facciamo il tifo perché fallisca. Noi facciamo il tifo veramente per il nostro Paese e facciamo il tifo perché queste misure, che sono in gran parte figlie del nostro Piano nazionale di ripresa e resilienza, arrivino fino in fondo e migliorino l'Italia.

favorevole del Partito Democratico alle risoluzioni delle opposizioni e contrarietà alla risoluzione della maggioranza di centrodestra. Il nostro è un voto politico per la contrarietà alla gestione che avete messo in campo da quando avete vinto le elezioni ad oggi ed è una critica nel metodo e nel merito. Lo è nel merito perché i primi mesi solo e unicamente su chi dovesse gestire i progetti, ossessionati da chi dovesse avere il controllo delle risorse - come abbiamo visto anche sulla gestione dei fondi dell'Emilia-Romagna - perdendo intanto l'attenzione all'attuazione dei progetti del Oggi noi non dovremmo essere qui a discutere di quello che non ha funzionato nella terza rata, in quegli obiettivi che dovevano essere chiusi entro dicembre 2022, e neanche degli obiettivi che dovevano essere chiusi entro giugno e che non avete ancora chiuso. Noi oggi dovremmo essere qui a discutere degli obiettivi della quinta rata del secondo semestre del 2023, 18 miliardi. Vi siete però dimenticati della *governance* nell'articolo più importante, il 9-*bis* del decreto-legge n. 152 del 2021, che dice che tutte le riforme e le proposte di modifica, ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento (UE) 2021/241, devono essere tempestivamente mandate alle Camere in modo tale che si possa utilmente discutere, approfondire e dare degli indirizzi chiari a questo Governo. tre giorni a cavallo di luglio e agosto per discutere delle proposte e delle modifiche che incidono così pesantemente sul futuro del PNRR? *(Applausi)*. lei ci ha elencato, nella proposta di modifica, ben 13 incontri della cabina di regia, una decina di incontri del gruppo tecnico del REPowerEU, un numero enorme di riunioni preparatorie agli incontri culminati nella visita della Commissione europea a giugno, in cui dice di aver fatto 35 riunioni tecniche: perché non ha trovato il tempo di venire una volta in Parlamento a raccontarci nel dettaglio i progetti, a vedere le schede dei progetti singolarmente? È questo il rispetto per il Parlamento? Mi sembra che non stiano meglio le Regioni e i Comuni (citofonare a Fedriga e a Decaro).

Posso anche capire il ragionamento che ha fatto, perché non diciamo che tutto va bene. Sappiamo che è un'opera complessa, che è un Piano maledettamente complicato e non la invidiamo per il lavoro che sta facendo, siamo persone responsabili, ci siamo passati prima di lei con il lavoro che abbiamo fatto, magari coinvolgendo un po' di più il Parlamento.

delle grandi città, ma anche i progetti di rigenerazione urbana, per i quali i Comuni hanno già aggiudicato i lavori e sono stati firmati i contratti, è stata fatta la revisione dei prezzi, per cui sono pronti ad aprire i cantieri. A queste comunità cosa diciamo?

le Vele di Scampia. Sappiamo come per quella città, e non solo, sia un intervento simbolico: 70 milioni, la riqualificazione di un'area, l'abbattimento delle ultime vele, 500 nuovi alloggi. Un segno di riscatto per quella città. secondo è il Parco della rinascita a Bari: 13 milioni, dove prima c'era la fabbrica della morte, la Fibronit, e c'era amianto; un segnale di riscatto delle periferie che metto in connessione, da questo punto di vista, anche con il messaggio cinico che avete mandato con gli SMS per la fine del reddito di cittadinanza. Dovevate mettere in grado i Comuni e le amministrazioni locali di affrontarlo perché, poi quando ci sono queste misure, le persone vanno dai sindaci, perché la disperazione le porta lì, Da questo punto di vista, la nostra proposta, ministro Fitto, è molto semplice: ripristinate quei progetti degli enti locali; ragionateci con l'ANCI e con le Regioni; tenete fuori solo quei progetti per cui avete l'assoluta certezza che non si arriverà a fine 2026. Mi rifiuto di pensare che progetti già avviati, per cui sono pronti ad aprire i cantieri, non possano essere portati a termine entro il 2026. Ripensateci. Inoltre, su quelli che spostate, entro il 31 agosto e comunque entro la fine del negoziato con la Commissione, indicate quali sono le fonti alternative, concertandole con Comuni e Regioni. Lei, infatti, ha citato - glielo voglio dire - il caso dei 15 miliardi che, prima con il Governo Conte II e poi con il Governo Draghi, abbiamo inserito

fare alcune considerazioni più generali che allungano e aggiornano l'elenco dei nostri dubbi. Più in generale noi percepiamo da parte di molti nella maggioranza (non tutti) una sensazione di fastidio nei confronti del PNRR, perché è stato costruito da noi, dal centrosinistra. Lo dico in riferimento a due casi rispetto ai quali dovete stare attenti anche nella narrazione e nei messaggi che passano: mi

venga attaccato da un membro autorevole di questo Governo solo perché osa a dire che ha dei dubbi sulla valorizzazione dei beni confiscati. *(Applausi)*. Sulla lotta all'evasione fiscale,

la delega fiscale con i concordati preventivi e le sanatorie, ma ci volete dire qual è il nuovo obiettivo? Su quello, infatti, ci giochiamo la credibilità nei confronti dell'Europa, che vuole capire se la lotta all'evasione rimane una priorità di questo Governo. È su questo che ci giochiamo la credibilità. con un tema su cui noi abbiamo costruito il PNRR che - come diceva prima il collega Patuanelli - è un patrimonio di tutti. Se vince l'Italia, vinciamo tutti. Se questo Governo porta a casa dei risultati, vinciamo tutti.

mancare uno dei punti fondamentali del PNRR, che noi avevamo pensato sì per uscire dalla crisi pandemica, ma per affrontare i nodi di competitività del nostro Paese, per legare un modello di sviluppo sostenibile alla crescita. Questa è la scommessa che abbiamo fatto e non vogliamo certamente perderla.

gli antichi romani erano maestri di saggezza e affidavano al tempo dei ruoli molto importanti, uno dei quali era quello di smascherare le menzogne e far trionfare

abbiamo assistito al peggiore circo della iattura da parte di una opposizione che ha preferito tifare contro il pagamento della terza rata, non comprendendo che un fallimento da lei mai manifestato equivaleva a un fallimento per la Nazione. dicevo, ogni cosa a suo tempo. All'indomani del nostro trionfo elettorale, il Governo ha dovuto farsi carico di portare a terra le risorse del PNRR;

il *post* pandemia, la guerra, il rincaro delle materie prime e dei costi dell'energia. Non considerare l'attualità, la situazione internazionale, i cambiamenti dell'economia mondiale è da irresponsabili, è un atto da persone in malafede. Credo che i colleghi, pur nella differenza di opinioni, non possano essere così in malafede da non riconoscere le tante congiunture che sono intercorse negli ultimi mesi e che hanno portato alla revisione del Piano. Ebbene, al di là dei gufi, mi consenta, Ministro, lasciamoli pure gufare questi colleghi dell'opposizione. Se i risultati sono questi, vuol dire che il Governo è su un'ottima strada, da oggi agli anni a venire. Siamo riusciti a ottenere il pagamento della terza rata ed è singolare come l'opposizione, offuscata dalla rabbia, non abbia notato come in questi mesi lei, ministro Fitto, sia stato uno dei Ministri più presenti in quest'Aula, trasmettendo sicurezza e serenità sul lavoro del Governo. Oggi votiamo favorevolmente plaudendo al lavoro immane che è stato svolto in operoso silenzio da parte sua, lontano dalle prime pagine dei giornali, lontano dalla propaganda ma attento ai fatti. Lei, Ministro, sta portando avanti un lavoro encomiabile, riconosciuto anche dalla Commissione europea per consentire il rispetto degli impegni presi e l'attuazione del Piano stesso. Lo abbiamo già detto e lo ribadisco: nessun taglio al PNRR, ma semplicemente una riorganizzazione dei progetti perché Fratelli d'Italia aveva detto in campagna elettorale che avremmo utilizzato le risorse del PNRR ma senza sprechi. *(Applausi)*. Questo è il concetto primario: senza sprechi. Le opposizioni quindi la smettano con la propaganda, una propaganda che fa male al Paese. Chiedete a piè sospinto le dimissioni di qualsiasi membro orbiti attorno al Governo. Sventolate bandiere intrise di demagogia. Ci accusate di tutti i mali del mondo, come se governassimo da dieci anni e non da soli dieci mesi. *(Applausi)*. Vi ricordo una cosa, cari colleghi: molti di voi, se non la maggior parte, hanno governato questa Nazione negli ultimi anni. Molti di voi hanno governato per dieci anni spesso senza legittimazione ma per inciuci e accordi indicibili che dicevate di non voler mai fare *(Applausi)* e che invece avete fatto. E questo è un dato politico. Pertanto, è il momento di parlare con il linguaggio della verità. È il momento di dire le cose come stanno, perché è facile giocare con i travisamenti. Ci sono 191 miliardi di euro del PNRR da spendere entro il 2026. Cosa fa un Governo serio? Cosa fa un Governo che, per dirla come la nostra Costituzione, si comporta come un buon padre di famiglia? Fa i conti con la realtà; individua quali sono le opere che si possono portare a compimento entro il 2026 e quali no. Sapete cosa succede se noi queste opere entro il 2026 non le portiamo a completamento? Dobbiamo restituire i soldi indietro. Bisogna essere quindi chiari e seri. Quindi questo Governo, che è appunto serio, rappresentato egregiamente dal ministro Fitto, rimodula, si confronta con la Commissione europea, individua le opere più urgenti per il Paese, realizzabili in tempi congrui e per quelle precedentemente inserite appronta la soluzione utilizzando altre fonti di Infatti - e qui il ministro Fitto è stato oltremodo chiaro - i fondi di coesione che hanno scadenze più lunghe, come il 2029, potranno finanziare le altre opere; quindi nessuno stralcio, nessuna cancellazione, ma una rimodulazione dettata dai tempi di realizzazione. E qui potremmo aprire un capitolo infinito, colleghi, che riguarda tutti. Il tempo di realizzazione in Italia di un'opera pubblica è un capitolo amaro; un capitolo, caro Presidente, su cui è necessario e urgente intervenire perché decisivo in questo caso per l'acquisizione delle risorse del PNRR, ma anche fondamentale per lo sviluppo della Nazione. Le stime più recenti ci dicono che gli investimenti per inferiori ai 100 milioni di euro sono infatti completati mediamente in 2,9 anni, mentre per le opere di importo superiore ai 100 milioni di euro sono necessari oltre anni per un'opera pubblica, e ancora c'è qualcuno che ha governato per dieci anni senza intervenire per invertire questa tendenza che sbraita sui giornali *(Applausi)* e accusa il ministro Fitto di rimodulare il Piano proprio in base ai tempi. Ritengo peraltro che la rimodulazione raggiunga obiettivi sinergici tra sostegno ai ceti con redditi bassi e tutela dell'ambiente. Infatti, un punto lodevole e degno di nota è quello della transizione *green* e dall'autonomia energetica, con l'innalzamento del REPowerEU che ha una dotazione di 19 miliardi, destinando circa 4 miliardi all'avvio di un ecobonus per le famiglie meno abbienti che in passato sono state escluse dagli interventi di efficientamento energetico delle abitazioni private, con un meccanismo di detrazione che va a sostenere chi davvero ha bisogno e in maniera sostenibile con i conti pubblici. La rimodulazione accolta dalla Commissione premia l'intendimento del Governo Meloni di puntare sulla crescita e sull'occupazione. Abbiamo messo nel motore propulsione del Paese le aziende piccole e medie, puntando sull'ecologia e sul digitale. In questi giorni di polemiche strumentali, di polemiche che soffiano sul fuoco gettando benzina sul malessere sociale relative al reddito di cittadinanza, la migliore risposta la diamo con i fatti: non con gli *slogan* di chi diceva che aveva abolito la povertà, ma con sostegno a chi

energetica (MASE) per la realizzazione dei progetti Snam, terna ed Enel per le reti energetiche ed elettriche. Attraverso il piano Transizione 5.0, con una dotazione di 4 miliardi di euro, sarà possibile sostenere le imprese negli investimenti necessari a realizzare progetti e al perseguimento di obiettivi di transizione ecologica e digitale. Restiamo sempre sul fuoco alimentato da voi, colleghi dell'opposizione, con le polemiche becere sul reddito e sul Sud. Il Sud è al centro dell'agenda di questo Governo, ma negli ultimi dieci anni è stato abbandonato da chi fino a qualche tempo fa

ma anche ad incentivi e crediti di imposta alle imprese che decidono di investire nel Sud. Inoltre, altrettanto positivo è il lavoro sull'energia. Il Sud può e deve essere un grande *hub* energetico: lo testimoniano i 500 milioni per il cavidotto sottomarino di Terna,

chi come me cittadino del Sud - è un settore cruciale, c'è un pacchetto di 14,8 miliardi sulla sostenibilità e sul fronte del *welfare.* Positivo il rafforzamento della misura sugli asili nido, con 900 milioni di euro per consentire un nuovo bando, visti i rincari delle materie prime, per raggiungere l'obiettivo dell'incremento sostanziale dei posti disponibili, ove, specie al Sud, si è in forte sofferenza. Complessivamente, l'aumento è pari a 2,5 miliardi di euro dei fondi del PNRR per le filiere agricole approvato dal Governo è fondamentale per il sostegno dell'intero settore agricolo. Mi accingo alla conclusione, signor Presidente. Ministro Fitto, l'*okay* alla rimodulazione del PNRR è un risultato straordinario, importante e atteso, ed è stato reso possibile grazie all'intenso lavoro di squadra che lei ha compiuto, da abile regista, con tutti i Ministri coinvolti. Ancora una volta abbiamo smentito i profeti di sventura che da settembre non fanno altro che sperare nel peggio per l'Italia. Questa volta le critiche infondate delle opposizioni vengono demolite dai complimenti arrivati dalla presidente della Commissione europea von der Leyen sui progressi e l'attuazione delle riforme e degli investimenti cruciali inclusi nel PNRR. Andiamo avanti con serietà, fermezza e passione. Andiamo avanti per l'Italia pensando non al domani e al rapido tornaconto elettorale, ma alle prossime generazioni: questo è, per noi, fare

ha accettato la proposta di risoluzione n. 5 dei senatori Malan, Romeo, Ronzulli e Biancofiore, che pertanto sarà votata per prima ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Regolamento,

trasporti Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica